sulle dimissioni reiterate da parte di alcuni senatori, sulle quali abbiamo già votato una prima volta. volta. Vi comunico che, per ragioni di funzionalità, bisognerebbe anticipare il voto sulle dimissioni dei senatori alla relazione della Commissione giustizia sul disegno di legge Mastella. C'è una ragione, perché

non si potevano lasciare inevase le speranze e le aspettative dei detenuti, al di là delle opinioni che ciascuno di noi ha sul provvedimento.

in tempi rapidi, proprio per evitare che le aspettative, così forti e drammatiche, nate all'interno dei penitenziari, andassero nuovamente deluse.

emendamenti, presentati però soltanto da tre Gruppi (questo, almeno, è accaduto in Commissione, e credo che lo stesso accadrà in Aula: non ho ancora avuto il tempo materiale di valutarlo, ma ritengo che sia così).

dell'ordine del giorno, nei termini in cui le ho riferito.

coerente la sua scelta, seppur nella discrezionalità della Presidenza. Non voglio entrare in polemica con quanto affermato dal collega Boccia, ma vi è una coerenza d'insieme da rispettare, e noi la apprezziamo.

Pur trovandomi d'accordo con la decisione assunta dai Capigruppo e nell'autonomia dell'Aula, chiedo dunque che anche l'Italia dei Valori, sottogruppo del Gruppo Misto, possa essere messa in condizione di sviluppare le sue argomentazioni tese al miglioramento del testo oggi al nostro

nell'assurda ristrettezza dei tempi così come imposti dalla calendarizzazione voluta all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo, che si ultimasse il lavoro in Commissione per fare in modo che vi fosse la possibilità in Aula di portare avanti un dibattito che fosse compiuto, magari aspro ma comunque fattivo. L'*iter* della proposta di legge in esame ha avuto inizio alla Camera dei deputati, dove sono state presentate numerose proposte di legge. Ad eccezione dell'Atto Camera n. 372, presentato il 3 maggio 2006, prima firma onorevole Iannone, tutte le proposte in questione - nove in totale - prevedevano la concessione sia dell'amnistia, sia dell'indulto. In data 18 luglio 2006, su richiesta della Commissione giustizia, l'Assemblea della Camera dei deputati deliberava lo stralcio delle disposizioni in materia di amnistia, ed infatti le disposizioni in materia di amnistia sono rimaste alla Commissione Giustizia della Camera in sede referente. Occorre subito considerare come l'ultimo provvedimento di clemenza approvato prima di quello che stiamo discutendo risalga al 1990 e che da allora per 16 anni - nessun provvedimento di amnistia o di indulto è stato approvato in conseguenza della nuova formulazione dell'articolo 79 della Costituzione.

nel trasferire esclusivamente in capo al Parlamento la procedura di adozione dei provvedimenti di amnistia e di indulto, mentre prima dell'approvazione della modifica la competenza ad adottare tali provvedimenti era assegnata al Capo dello Stato sulla base di una legge di delegazione approvata dal Parlamento; la seconda, La seconda modifica - individuazione di una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei componenti di di ciascuna Camera per ogni suo articolo e nella votazione finale - è stata prevista, probabilmente, dal legislatore per autolimitarsi e per non incorrere in un uso distorto degli strumenti di clemenza generale previsti dall'ordinamento costituzionale. Ed infatti i 21 provvedimenti di clemenza che si sono succeduti tra l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e la revisione dell'articolo 79 del 1992, in gran parte, rispondevano ancora alla tradizionale concezione indulgenziale degli istituti che, provenienti dallo strumentario della *indulgentia principis*, si prestavano al libero arbitrio di un sovrano *legibus* *solutus*. Dal punto di vista dell'efficacia deflazionante, va detto che la legge costituzionale del 1992 ha raggiunto il suo scopo, non essendo stato approvato da allora alcun provvedimento di amnistia o di indulto e su tale tematica vi è stato un dibattito profondo, anche ad esempio nella XIII legislatura, ponendosi il problema se un *quorum* così elevato non finisse poi per determinare una sorta di paralisi di quello che può essere considerato anche come uno strumento di politica criminale. A mio avviso, ragionando sull'articolo 79, è giusto mantenere all'amnistia e all'indulto il carattere della eccezionalità, per lunghi anni obiettivamente disattesa, e quindi è necessario mantenere la previsione di un *quorum* qualificato più rigoroso rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie, anche se però un *quorum* dei due terzi appare in questo momento anacronistico. appare anacronistico, se consideriamo, ad esempio, che è un *quorum* molto più alto di quello previsto per le leggi di revisione costituzionale. Nel merito del provvedimento, il punto di partenza è sicuramente rappresentato dall'indiscusso sovraffollamento delle carceri e dalle connesse e disagiate condizioni in cui versano le persone ristrette. Le carceri italiane ospitano circa 16.000 detenuti in più rispetto ai posti disponibili: a maggio di quest'anno i detenuti erano 61.353 a fronte di una ricettività regolamentare di 45.490 posti. Su questi dati poi, in ogni caso, il Governo, che dovrebbe aver operato un aggiornamento, potrà fornire ulteriori precisazioni. Le esigenze sottese all'adozione del provvedimento di clemenza attengono tutte ai principi in materia di esecuzione della pena. Innanzitutto, vi è l'esigenza di salvaguardare il rispetto del divieto costituzionalizzato di trattamenti contrari al senso di umanità e ad essa, strettamente correlato, si affianca il doveroso rispetto del principio di rieducazione della pena, principio destinato a non trovare attuazione concreta, attesa l'assenza di condizioni ambientali dignitose: non è possibile che un detenuto che si trovi e vivere in condizioni disumane possa davvero portare a compimento un percorso rieducativo. La pena deve essere sicuramente anche afflittiva, ma quando è disumana non può garantire alcun reinserimento sociale. In sostanza, l'adozione del provvedimento, lungi dall'essere un mero atto di indulgenza, risponde all'improcrastinabile necessità di ripristinare una situazione di vivibilità e quindi di legalità delle carceri: nessuno può concedersi l'ipocrita lusso di far finta di non sapere o di non vedere quel che sta accadendo nel nostro sistema carcerario. Il disegno di legge al nostro esame dispone, al comma 1, la concessione dell'indulto, causa estintiva della pena che presuppone l'accertamento della colpevolezza dell'imputato, per tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006. La fissazione del limite temporale - 2 maggio 2006 - risponde astrattamente al parametro costituzionale del terzo comma dell'articolo 79, in forza del quale amnistia ed indulto non possono applicarsi a reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge all'evidente fine di evitare che si possa delinquere nelle more della presentazione del disegno di legge, confidando appunto sulla impunità futura. Tuttavia, appare corretto sottolineare - ed è il primo elemento che il relatore sottopone all'Assemblea - come la data del 2 maggio 2006 appaia troppo vicina a quella di presentazione della prima proposta - Atto Camera n. 372 del 3 maggio 2006 - e quindi sostanzialmente inadeguata. Sarebbe stato più corretto far riferimento ai reati commessi almeno prima delle consultazioni politiche, essendo questo un tema del quale si parla da tempo e di cui si è parlato anche in campagna elettorale. Questa, ad avviso del relatore, è una prima concreta inadeguatezza di un termine di riferimento essenziale della normativa. Il primo comma continua prevedendo che l'indulto è concesso nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive, e non superiore a 10.000 euro per le pene pecuniarie sole o congiunte a pena detentiva. Quanto all'individuazione in tre anni della misura dell'indulto, si è ritenuto che una misura più ridotta non avrebbe consentito il conseguimento di apprezzabili risultati in termini deflattivi, anche se (ed è il secondo dato che il relatore sottolinea con forza all'Assemblea) i precedenti specifici di provvedimenti di indulto non prevedevano mai pene superiori ai due anni. In sostanza, abbiamo un'innovazione rispetto al limite quantitativo che viene previsto. Sul punto occorre considerare tutti gli effetti che un tale provvedimento di clemenza comporta. che secondo i dati che il Governo ci ha fornito dovrebbero interessare 12.700 persone circa (anche su questo il Governo che interverrà dopo potrà precisare sicuramente meglio), dobbiamo considerare gli effetti successivi, gli effetti differiti, dell'indulto per l'intero sistema penale, effetti che dureranno svariati anni con riferimento ai processi che dovranno comunque celebrarsi per tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006. La terza anomalia che il relatore sottopone alla valutazione dell'Aula è quella relativa alla previsione dell'indulto per le pene pecuniarie fino a 10.000 euro, giacché non si comprende quale rapporto possa mai avere tale previsione con la problematica correlata al sovraffollamento delle carceri.

ad altre fattispecie di reati (mi riferisco per esempio alle contravvenzioni per le violazioni sulle leggi che regolano la sicurezza nel mondo del lavoro) che stranamente vengono in questo modo assolutamente depotenziate. Nel prevedere che non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale, la disposizione che stiamo per approvare comporta l'applicazione dell'indulto anche nei casi di recidiva di cui all'articolo 99 del codice penale per i delinquenti abituali o professionali o per tendenza. Questo, è evidente, risente dell'approvazione nella scorsa legislatura

prevedeva anche la possibilità di estinzione delle pene accessorie, ma tale disposizione è stata soppressa dall'esame dell'Aula. Il comma 3 è stato oggetto di un'ampia discussione nell'altro ramo del Parlamento, sia in Commissione sia in Aula. Esso attiene all'individuazione tassativa delle fattispecie penali escluse La predetta individuazione è stata operata, nel rispetto del principio di parità di trattamento e oltre i limiti di pena astrattamente fissati dal legislatore, sulla base del particolare e maggiore allarme sociale di alcune fattispecie criminose e quindi sulla scorta di un criterio oggettivo di ragionevolezza. Ma se questo è il parametro, se questa è la stella polare che ha guidato il legislatore che ha già provveduto all'approvazione del disegno di legge che viene sottoposto oggi all'esame del Senato, non appare assolutamente tranquillizzante, in questa logica, la mancata esclusione dall'applicazione dell'indulto che viene deciso della fattispecie relativa all'articolo 416-*ter* del codice penale, relativo al reato cosiddetto di voto di scambio mafioso, assolutamente non riconducibile, ad avviso del relatore, nell'altra autonoma fattispecie prevista dall'articolo 416-*bis*. Il ragionamento è sostanzialmente il seguente: è evidente che nel ragionare della capacità di individuare quali sono i reati che provocano un maggiore allarme sociale ogni interprete mette in campo le proprie esperienze, la propria cultura, la propria sensibilità, e quindi utilizza criteri abbastanza soggettivi. Quando però un'intera categoria di reati viene comunque ricompresa, e mi riferisco al fatto che il disegno di legge al nostro esame preveda già espressamente l'esclusione dall'applicazione dell'indulto delle misure previste dall'articolo 416, comma

in quella valutazione astratta, cercando di ripercorrere, come dire, i confini esterni della scelta, una discrasia appare evidente ed è un'anomalia che il relatore sottopone alla valutazione dell'Assemblea. Degna di rilievo appare, infine, la previsione della revocabilità del beneficio in questione nell'ipotesi di ricaduta nel delitto nei cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento: essa sicuramente rappresenta uno strumento preventivo per il corretto funzionamento dell'istituto. Consentitemi adesso di svolgere una brevissima considerazione politica di natura finale. Non possiamo non considerare che qualunque misura di clemenza, proprio per la sua eccezionalità, andrebbe preceduta - o almeno accompagnata - da una serie di riforme che servissero a rimuovere le cause che hanno determinato l'emergenza. Nel caso di specie, una riforma del codice penale, accompagnata magari da una robusta depenalizzazione e da una rivisitazione dei criteri generali di politica carceraria con la previsione di misure alternative alla detenzione inframuraria, avrebbero contribuito a rendere più giustificabile un provvedimento di indulto che, invece, rimuove un effetto negativo (il sovraffollamento delle carceri) senza intervenire minimamente sulla patologia esistente. Speriamo che l'Aula abbia la forza di affrontare i nodi critici di questo provvedimento che - come ho detto - attengono alla quantificazione della misura, alla incomprensibile previsione delle pene pecuniarie e all'esclusione arbitraria di alcune figure di reato, ma, come sempre, saremo pronti a confrontarci liberamente, sperando che alla fine possa prevalere la ragionevolezza ed il buon senso, consapevoli delle aspettative che ormai si sono create, in un mondo come quello carcerario che si alimenta con la sofferenza e la disperazione. Non è giusto semplificare chiedendoci di scegliere fra Caino ed Abele, signor Presidente, perché in un Paese civile bisogna sempre farsi carico delle ingiuste sofferenze di tutti, anche di quelli che hanno sbagliato.

Onorevole Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, è il primo intervento in materia giudiziaria del nuovo Parlamento e di questo Senato. si faceva e si fa sì riferimento ad atti di clemenza (amnistia e indulto previsti dall'articolo 79 della Costituzione), ma in esso si legge chiaramente da adottare però dopo, o contemporaneamente, comunque in coerenza con una organica riforma del codice penale e del relativo codice processuale. Siamo invece in presenza di una proposta di indulto senza amnistia e senza riforme, anzi di una proposta di indulto in contrasto con la riforma che l'Unione, negli ultimi cinque anni, ha invocato contro il lassismo fatto di depenalizzazioni di reati societari e di conflitto di interessi. L'indulto, per il quale è richiesta la maggioranza dei due terzi, è atto parlamentare, è atto di grande delicatezza perché incide sulla divisione dei poteri: consente al legislativo di annullare in tutto o in parte una formale sentenza giudiziaria. Sostenere la necessità di un atto di indulto anche per ridurre il sovraffollamento delle carceri, invocando un sistema carcerario civile, ricordare l'esigenza di umanizzare la pena è parte del programma di Italia dei Valori, è parte del programma dell'Unione, è parte del programma di gruppi ed esponenti politici di entrambi gli schieramenti. Ma che rapporto ha con tali esigenze? Italia dei Valori non è contraria all'indulto, è contraria a questo indulto. Si escludono dall'indulto, nella proposta oggi al nostro esame, alcuni reati ritenuti di particolare allarme sociale. Non si escludono (rivelando un'inaccettabile mistificazione) reati ritenuti di non particolare allarme sociale. Non è di particolare allarme sociale l'estorsione? Non sono di particolare allarme sociale i reati contro la pubblica amministrazione? E ancora: peculato, concussione, corruzione in atti d'ufficio non sono reati di particolare allarme sociale? Un corruttore di magistrati e magistrati corrotti non determinano un clima e un particolare allarme sociale? Avvelenare le acque e adulterare alimenti non produce particolare allarme sociale?

non produce particolare allarme sociale applicare questo indulto a questi reati? E ancora, non produce particolare allarme sociale applicare questo indulto a questi reati commessi sino al 2 maggio 2006, reati commessi, ancorché non contestati, per i quali ancora non è stata avviata alcuna azione penale? Non produce particolare allarme sociale tale termine finale del 2 maggio 2006, con un termine iniziale che risale all'ultimo provvedimento di indulto, ad oltre sedici anni fa? Si propone uno scandaloso colpo di spugna per i reati sino al 2 maggio 2006, cui si aggiunge un incredibile *bonus* per reati che verranno contestati e magari accertati fra quattro o cinque anni? Il messaggio è chiaro: chi sbaglia non paga. Un indulto che diventa un insulto per magistrati, poliziotti, carabinieri e finanzieri, ai quali questo Parlamento si accinge a mandare un messaggio devastante: lavorate, indagate, rischiate rappresaglie e conflitti a fuoco, ma ai criminali che riuscirete a individuare e condannare viene dato un *bonus* di impunità. Un insulto, una derisione. Un insulto, una derisione per quella cultura della legalità che avrebbe dovuto marcare la differenza tra una maggioranza e un Governo nato anche sull'onda dell'indignazione per la questione morale e il precedente Governo. Questa legislatura, che avrebbe dovuto essere la primavera dopo l'inverno appena trascorso, rischia di consolidare sfiducia nella giustizia e di passare alla storia del nostro Paese come la legislatura della cultura dell'illegalità. Italia dei Valori vuole impedire che questa legislatura, in materia giudiziaria, si apra con un vero e proprio sequestro: il sequestro della speranza di legalità e trasparenza; il sequestro da parte di criminali dal colletto bianco; il sequestro di migliaia e migliaia di disperati, in carcere per reati che potrebbero essere depenalizzati, i quali potrebbero essere scarcerati con legge ordinaria (a maggioranza semplice e senza nessun accordo).

Signor Presidente, signori del Governo, colleghi senatori, il tema dell'indulto non merita gli allarmismi ai quali ha fatto ora riferimento il collega che mi ha preceduto. Si tratta di un tema che presuppone ed esige riflessione, ponderazione, ragionamento e forse sarebbe stato utile non relegarlo in un ritaglio di tempo, in un sabato. Solo su questo punto condivido le anomalie etiche ed estetiche alle quali ha dato luogo l'onorevole Di Pietro nei giorni scorsi. Stiamo assistendo effettivamente ad una gravissima anomalia. Di Pietro ha messo in atto una contrapposizione barbarica ed offensiva nei confronti di deputati e senatori. La *criminal* *list*, alla quale ha dato luogo con la visualizzazione fuori del Senato, costituisce una ulteriore lacerazione etica ed estetica; non è una novità, per chi disistima Di Pietro da tempo. E Di Pietro non può né deve invocare la categoria della moralità e della immoralità, perché non può dividersi il Paese fra persone che sono dotate di moralità, se sono contro l'indulto, e di immoralità, se sono a favore dell'indulto L'onorevole Di Pietro la deve smettere di guaire. E se il collega senatore Calvi gli ha risposto riesumando una sofisticata categoria giuridica, quale quella della irricevibilità, se, ancora, il Capogruppo dell'Ulivo, senatrice Finocchiaro, gli ha risposto evocando un famoso testo di Molière (ma credo che non lo abbia capito io voglio qui affermare in maniera solenne e forte che Di Pietro, con questi toni falsamente ed ipocritamente moralistici, non può continuare ad eccitare i bassi istinti della popolazione, mescolando ad un basso populismo una grande dose di opportunismo, perché continua a non dimettersi da ministro della Repubblica Colleghi senatori, tutti avremmo preferito discutere in altri termini di questo indulto. Avremmo preferito parlare di concomitanti e contestuali riforme strutturali; avremmo preferito discutere di programmi seri e concreti di edilizia carceraria differenziata; avremmo preferito parlare della organicità del lavoro previsto dalla Costituzione ai fini rieducativi di cui all'articolo 27; avremmo voluto parlare della necessità di un rinnovamento normativo, di un codice penale minimo che inseguiamo da anni,

Avremmo potuto e voluto collegare l'adempimento delle riparazioni civili, anche se ci rendiamo conto che si tratta di un terreno impervio e difficoltoso che potrebbe discriminare il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Io condivido perfettamente questo catalogo di richieste e proposte che Alleanza Nazionale ha portato avanti anche nel corso di questo dibattito. E apprezzo ancora di più il mio partito perché rispetta la diversità delle opinioni, e rispetta, in particolare, la diversità del mio dissenso: abito, questo, di Alleanza Nazionale ispirato a democrazia e a libertà. Dobbiamo porci velocemente alcune domande. La prima: cosa prevale nella valutazione e nello stimolo a votare a favore, come farò, dell'indulto? al tono estremistico, allarmistico che ho oggi letto in una intervista rilasciata da un autorevole senatore della Repubblica a «la Repubblica»? Gli assassini in libertà? 60.000 detenuti fuori delle carceri? Sono numeri che non esistono. La impunità alla quale fa riferimento continuamente in maniera distorta l'onorevole Di Pietro?

uscire, i detenuti per omicidio nelle carceri italiane, non superano, o superano di poco, le 2.000 unità. Se dovessero uscire in virtù di questo indulto, essi avrebbero già certamente espiato la maggior parte della pena, quindi avrebbero pagato il debito nei confronti della società. Per gli altri si tratta di una rimessione in libertà assai differenziata nel tempo, quando avranno scontato gran parte della pena. Non dobbiamo dunque introdurre false ed inutili suggestioni. Certamente nessuno di noi è contento del catalogo di esclusioni oggettive, anche se questo catalogo è molto più ampio di quello dei precedenti condoni. Per esempio, noi abbiamo cercato di introdurre l'omicidio aggravato dalle sevizie, ma i tempi della discussione in seno alla Commissione non hanno consentito l'approvazione di questo emendamento, che ripresenteremo in Aula. Vi sono però altri motivi che debbono essere considerati e che, in una gerarchia di prevalenza e in uno stimolo valutativo, mi inducono a votare a favore dell'indulto:

il numero di sieropositivi crescente; il numero di coloro che sono affetti da altre grave malattie, anch'esso crescente; le difficoltà per l'avviamento al lavoro. Un amico e un grande penalista del nostro Paese, Tullio Padovani, ha scritto che nelle carceri italiane si è al confine fra la legalità e la illegalità istituzionale. Si tratta di una situazione non più sostenibile, di una situazione sulla quale bisogna intervenire in maniera strutturale, ma anche in maniera immediata, topica, urgente. Questa misura può premiare le possibilità di intervento, domani in maniera strutturale, se vi sarà la volontà del Parlamento, la convergenza delle forze di maggioranza e di opposizione. Si tratta di una precondizione assolutamente importante per poter avviare il grande processo di ristrutturazione riformatrice del sistema penitenziario italiano. Ma l'indulto porta con sé un altro effetto non secondario, quello che i giuristi chiamano l'indulto improprio, cioè la deflazione giudiziaria. E, in un momento come quello attuale, questi due elementi si sommano l'uno all'altro per determinare condizioni che possono domani farci discutere con maggiore tranquillità, con maggiore lucidità, senza l'urgenza dei bassi istinti ai quali fa riferimento l'Italia dei Valori inseguendo qualche briciolo di voto. è però un altro motivo, signor Presidente e colleghi senatori, che non possiamo dimenticare: l'indulto è normato nel codice penale del nostro Paese; l'indulto è previsto nella Costituzione del nostro Paese.

L'indulto ha una sua ispirazione umanitaria di carattere giusnaturalistico e di carattere costituzionale. L'indulto appartiene alla storia del nostro Paese e, se nel passato si è fatto abuso dell'indulto, non possiamo dire che se ne sia fatto abuso dal 1990 ad oggi. E, se oggi siamo costretti, anche in maniera indiretta, ad intervenire con questo strumento, è perché la situazione è divenuta veramente intollerabile. Questi motivi, anche di carattere umanitario, non falsamente, stupidamente e ipocritamente umanitario, mi spingono a scegliere questa posizione. Voglio ancora in chiusura ricordare, colleghi senatori, che, quando la casa brucia, certamente bisogna progettare un nuovo edificio, ma la prima cosa da fare è spegnere l'incendio. Voglio contribuire con il mio voto favorevole a spegnere questo incendio.

personalmente ritengo che la legge sull'indulto sia una legge, oltre che necessaria, sostanzialmente giusta, e ciò perché è mia ferma convinzione che il grado di evoluzione e civiltà di uno Stato lo si valuti anche dal modo in cui esso attua la pena. In tale ottica è intollerabile che strutture carcerarie con una capienza di 40.000 detenuti, come le nostre, ne ospitino attualmente 62.000. È pacifico, almeno credo lo dovrebbe essere tra di noi, che il vertiginoso aumento della popolazione carceraria non vede certamente come suoi protagonisti soggetti appartenenti alle classi dirigenti (i cosiddetti colletti bianchi), essendo al contrario alimentato prevalentemente da tossicodipendenti, extracomunitari - qui la legge cosiddetta Bossi-Fini ha dato il suo contributo in maniera rilevante - e soggetti ai margini della società. Tutti elementi che gravitano nell'ambiente carcerario senza alcuna prospettiva - ripeto, senza alcuna prospettiva - di reinserimento sociale. Su questi soggetti si è abbattuta la scure della tolleranza zero, veicolata dalla legge ex Cirielli, destinata ad aumentare continuamente il numero dei detenuti se non prendiamo provvedimento e sono anche l'effetto delle scelte politiche operate dal precedente Governo di essere molto forte con i deboli e molto, molto debole con i forti. È evidente che l'approvazione del solo indulto non sarà sufficiente a riportare la popolazione carceraria entro i limiti di capienza, non essendo un atto di clemenza idoneo ad azzerare gli effetti di una cattiva legislazione che ha puntato, negli ultimi anni, esclusivamente all'inasprimento delle pene, senza curarsi minimamente della funzione

che vi sia urgenza di pianificare un programma di recupero e di reinserimento sociale dei detenuti, implementando l'organico delle carceri, mediante la presenza non solo di personale cosiddetto normale, che è sotto organico, ma anche di personale medico e di assistenti sociali, attuando ed attivando istituti di pena alternativi che consentano il reale reinserimento del detenuto. Tutto ciò non senza aver rivisto prima le leggi che hanno portato nelle carceri un'imponente quantità di soggetti emarginati, per i quali dovrebbero e potrebbero essere previsti sistemi di pena alternativi alla detenzione in carcere e per i quali in precedenza la detenzione non era affatto prevista. Ciò detto, posto che è prevista una maggioranza qualificata per

Però tale principio di ragionevolezza e buonsenso politico non può, ripeto, non può travalicare dei limiti, come quello dell'inclusione del provvedimento di condono dei delitti di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, cioè il voto di scambio mafioso, che non ha nulla a che fare con

che nella norma siano inclusi i reati societari, i reati fiscali, i reati contro la pubblica amministrazione. Per queste motivazioni, insieme ad altri colleghi

Va da sé che riteniamo che una norma di clemenza sia giusta e che quindi sia necessario che anche questo ramo del Parlamento

essi vengano condonati attraverso l'indulto. Per questo chiedo all'Assemblea di approvare questi emendamenti. Infine, anche se mi è stato mi è stato spiegato da autorevoli rappresentanti di quest'Aula, che sino ad oggi, nessun provvedimento di indulto ha escluso dal proprio ambito di operatività i reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ritengo che l'odierna inclusione che l'odierna inclusione nel provvedimento di indulto sia un segnale particolarmente negativo e grave e, soprattutto, molto contraddittorio rispetto allo stato attuale del dibattito socio - politico che si è svolto in questa materia. Infatti, uno dei primi interventi del Capo dello Stato ha avuto ad oggetto proprio la stigmatizzazione del fenomeno delle morti bianche, e ripeto, bianche,

la Commissione parlamentare d'inchiesta speciale sull'argomento degli infortuni e delle morti bianche sul lavoro. Una delle prime norme poste all'ordine del giorno è quella relativa ad una parte di questo fenomeno che riguarda la questione dell'amianto. Anche per queste motivazioni annuncio che ho presentato un emendamento in questa direzione. Ritengo sia utile e necessario che l'Assemblea escluda i reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro. Tra l'altro in carcere non vi è mai stato, nella storia della nostra Repubblica, un datore di lavoro che ha coscientemente provocato la morte di lavoratori,

*ad horas* non sono nelle condizioni di dare assicurazione che il mio voto sarà favorevole. Deciderò nel corso del dibattito e alla fine della discussione.

fondamentalmente contrari a questo provvedimento. Abbiamo, tuttavia, deciso di assumere un atteggiamento responsabile e rispettoso verso questo provvedimento, sul quale non siamo - ripeto - assolutamente d'accordo. è stato un ramo del Parlamento che ha votato; non possiamo far altro che prendere atto di questo voto, lo rispettiamo. Il prosieguo del dibattito, quindi, per noi sarà improntato a non tanto di ostacolare l'approvazione di questo provvedimento, quanto piuttosto di migliorarlo. Infatti, colleghi, vi invito tutti a leggere esattamente cosa c'è scritto nel provvedimento dal punto di vista tecnico. tecnico. Esso non ha mai avuto eguali in tutta la storia della Repubblica. In tutta la storia della Repubblica non vi è un provvedimento di questa natura che di fatto - ed è vero, lo confermo, posso portare i conti - libererà

luogo, per rivendicare il ruolo fondamentale del Senato: non possiamo essere, su una questione così importante, la mosca cocchiera della Camera. In secondo luogo, vi sono alcune correzioni che vanno apportate per forza, che bisogna assolutamente

approfondire un'altra questione fondamentale. Si dice: intanto liberiamo tutti; intanto diamo questo segnale di resa; intanto tutti i delinquenti e i criminali andranno in giro nel mese di agosto, quando la gente è in vacanza (pensate quali problemi di ordine pubblico!); poi faremo le riforme, poi vareremo i piani. vareremo i piani. I piani per costruire nuovi penitenziari e per far fronte al sovraffollamento ci sono già, sono al Ministero della giustizia, alcuni anche innovativi. Io ho presentato l'ordine del giorno

che consentirà di costruire a costo zero e rapidamente nuovi penitenziari. Credo che questa sia l'unica via civile, rispettosa della volontà di giustizia e sicurezza dei nostri cittadini, per rispondere al problema effettivamente esistente di garantire la dignità ai detenuti.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatrici e senatori, l'indulto, come previsto dall'articolo 79 della nostra Costituzione, è un provvedimento di clemenza che condona totalmente o parzialmente la pena, e la proposta di legge di concessione dell'indulto, che qui oggi si discute, rappresenta lo strumento da adottare d'urgenza per migliorare, almeno in parte, le condizioni delle carceri, il cui sovraffollamento fa sì che l'esecuzione della pena assuma forme disumane, violando non solo la dignità dell'uomo, ma anche il principio rieducativo della sanzione penale stessa. Sovraffollamento, dicevo: infatti, basti pensare che nei 200 penitenziari italiani, che hanno una capienza massima di 42.959 unità, sono detenute 61.392 persone, di cui la prevalenza risulta composta da migranti e tossicodipendenti. L'indulto che si discute costituisce un provvedimento essenziale per contenere la profonda crisi delle strutture penitenziarie. Mai, come negli ultimi anni, si sono intensificate le proteste, le richieste di interventi, finanche i suicidi di detenuti, costretti a scontare pene, a subire la custodia cautelare in condizioni di disagio che violano il diritto fondamentale ad un vivere dignitoso, stipati per lo più fino ad un numero di otto per ogni cella, condizioni, queste, che determinano paradossalmente effetti criminogeni, in netta contraddizione con la finalità risocializzante della pena. Ma il testo in discussione non è soltanto un provvedimento ispirato al solo «clemenzialismo», ma spinge verso un sacrosanto riordino complessivo del sistema penale italiano, che necessita della depenalizzazione di numerosi reati sociali e legati all'emarginazione. Per il prossimo anno si prevede che più di ventimila persone rischino il carcere con le migliaia di procedimenti contro i movimenti sociali e grazie a leggi proibizioniste e razziste come la Fini-Giovanardi sulle tossicodipendenze, la ex Cirielli, che esclude i recidivi da molti benefici penitenziari, e la Bossi-Fini sui migranti. Il carcere, credetemi, non può e non deve permanere nella sua condizione di discarica sociale. Occorre che la società, il mondo della politica, le istituzioni si facciano carico, carico vero, partecipato, della rimozione delle condizioni socio-ambientali ormai croniche che stanno all'origine dei reati e della disuguaglianza dei cittadini, rispondendo in tal modo anche al dettato costituzionale dell'articolo 3. Vorrei però tornare al carattere riabilitativo del sistema reclusivo che dovrebbe e deve prevalere su quello giustizialista. La rieducazione e la reintegrazione sociale sono diritti da garantire, attraverso il detenuto che lo esercita, alla società, ad una società che si dà delle regole che aprono le porte alla civiltà, all'evoluzione del pensiero sociale, piuttosto che precluderne l'ingresso fortificando il muro del «vendettismo» e dell'intolleranza. Inoltre, ci sono diritti violati, come quello alla salute, alla *privacy*, al rispetto e alla considerazione, su cui non si può tacere. La tutela dei diritti non può discriminare tra i soggetti che li detengono. È dalla loro violazione che prende corpo una cultura ed un *modus operandi* che genera violenza. C'è solo l'imbarazzo della scelta. In Italia la violenza nelle carceri ha fatto ritenere indispensabile alla magistratura l'apertura di numerose inchieste. Dal 1991 al 1997, infatti, sono stati firmati dai giudici 237 rinvii a giudizio a carico di agenti di custodia per lesioni, percosse, minacce e ingiurie, 129 per violazione della legge sugli stupefacenti, 66 per abuso d'ufficio, 24 per omicidio volontario e colposo e 13 per atti di libidine. Nel carcere di Secondigliano sono alla sbarra in questi giorni venti agenti penitenziari accusati dai giudici di Napoli di violenze a danno dei detenuti, alcuni dei quali avevano anche modi «ricercati» per le punizioni, come, ad esempio, «costringerli in tempi diversi a rimanere rinchiusi in un montacarichi in piedi con la faccia al muro» e tutto per futili motivi. Nel carcere di Nuoro, Luigi Acquaviva, un detenuto, che aveva partecipato ad una protesta, viene trovato morto alcuni giorni dopo quell'episodio: suicidio? Ma successivamente tre agenti vengono indagati per lesioni ed un quarto per omissione di soccorso. Le carceri, con le loro diverse problematiche ambientali, sono deleterie non soltanto per la vita dei detenuti ma anche per coloro che vi lavorano. Lo Stato, con le sue risposte, i suoi provvedimenti, le sue disposizioni, si riflette negli occhi di quelle persone, perché i detenuti sono persone, e la luce che ne traspare non è lusinghiera - credetemi - e neanche il silenzio di chi ha smesso di chiedere alle istituzioni e credere nell'equità sociale e nella giustizia. Io le ho incontrate quelle persone

«Mi chiamo Enrico e sono detenuto presso la Casa circondariale di Fuorni. Santo Iddio, siamo emarginati dal mondo qui. Qui è pieno di ragazzi che per uno spinello finiscono in carcere, mentre i potenti che hanno forse commesso reati molto più gravi, magari rovinando migliaia di persone, stanno fuori e dopo alcuni anni te li ritrovi nelle liste elettorali». «Anch'io mi chiamo Enrico, sono mesi che aspetto una visita medica perché affetto da fistole coccigea con pus senza che venga disinfettato. Mi lavo con acqua corrente e basta». «Mi chiamo Michele (II sezione) ho un figlio di quindici anni invalido al cento per cento con un problema al cervello ed anche mia moglie è ammalata, ma non mi danno gli arresti domiciliari». «Io sono Domenico, qui le lenzuola le cambiano ogni 4-5 mesi. Non ci sono neanche libri da leggere ed il tavolo è rotto. C'è stata un'epidemia di scabbia e abbiamo dovuto comprarci la crema da soli perché nessuno ce la dava». «Io mi chiamo Michele. Ho una gamba con un tutore perché è stata operata ed è più corta, ma il tutore si è rotto, nessuno mi accompagna e sono venti giorni che non scendo a fare la passeggiata, sto sempre qua, come un topo». «Sono Antonio. Io quando sono venuto non facevo le mie cose al bagno, perché mi si poteva vedere, sta nella stessa stanza la tazza e ha una piccola porta e si vedono la testa e le gambe con i pantaloni abbassati, mi vergognavo, ma poi...». «Io sono Daniela dicono che sono mezza pazza, perché pulisco sempre, ma qui cade l'intonaco e perde il bagno di sopra, che devo fare? E poi il caldo. Si fa l'ultima doccia di venerdì, e poi si riprende il martedì. E, quindi, noi siamo in una condizione di precarietà igienica: abbiamo, oltre alla tazza, un lavandino, dove laviamo i piatti e ci laviamo anche noi». Credetemi, non è certamente solo con l'indulto che potremo fornire risposte e dignità a tali voci; è certo un atto di clemenza che dà inizio ad un percorso che ci vuole tutti impegnati nella costruzione di un progetto detentivo coerente con lo spirito della nostra Costituzione.

ha consentito ad alcuni di noi di assecondare le proprie pulsioni culturali rispetto a questa vicenda, che è una vicenda tutta particolare. Signor Presidente,

Non posso non evocare un paragone rispetto ad altre aree politiche di questo Parlamento che hanno manifestato la propria opposizione sbracciandosi, urlando, offendendo, non apportando alcun costrutto al dibattito, rivelando un atteggiamento con il quale si deve assolutamente dissentire. L'onorevole Di Pietro si è autosospeso dalle proprie funzioni ...

coalizione e imponendo repliche che rivelano tensioni e malumori che vanno al di là del fatto specifico, signor Presidente. Sono momenti che rivelano atteggiamenti in conflitto, con i quali non credo che i nostri contraddittori politici, l'attuale maggioranza, possano andare avanti per molto tempo. invece, l'atteggiamento all'interno di Alleanza Nazionale: molti voteranno contro l'indulto, la più parte. La maggior parte assumerà un atteggiamento critico che rispettiamo, e rispettiamo profondamente, perché cogliamo appieno come esso sia interprete di un malcontento diffuso; questa mancanza di regole che nel Paese si vive e che determina fatalmente esigenze che debbono essere comprese. Mancanza di regole: detenzione; mancanza di regole: carcere, forme di appagamento da parte di un'opinione pubblica che per queste cose è tormentata e che forse non riesce ad intendere, e non a torto, le ragioni per le quali si può essere favorevoli ad un atto clemenziale. Ma c'è un argomento, signor Presidente, onorevoli colleghi, che intendo sottoporre alla vostra attenzione, come argomento determinante, a mio avviso, perché si possa considerare con occhio diverso questa vicenda che involve emozioni, culture e sentimenti. Non solo 61.000 detenuti vivono in una condizione che è già stata ampiamente

che la pena sia scontata per intero. Ma la pena del reo, la pena di chi ha commesso il reato, la pena di chi suscita l'indignazione si traduce anche nella pena dell'innocente, signor Presidente. Gli imputati, i detenuti passano, la gente che serve lo Stato, che tutela lo Stato, che assume dei rischi resta in galera.

lo sottolineo, perché lo spirito costituzionale questo impone: non soltanto di custodirli, ma di educarli. Mettiamoli in condizione di fare il loro lavoro. Bisogna avere rispetto di costoro, e rispetto grande. Ecco, signor Presidente, la ragione prevalente per la quale io mi accosterò a questo provvedimento con un atteggiamento differente rispetto alla maggioranza dei miei compagni di partito, con un atteggiamento che è tollerato, con un atteggiamento che forse da molti non è compreso, ma questa è la vera ragione. Lo studio fatto da un insigne studioso dell'università di Messina, signor Presidente, ha rivelato che il 90 per cento dei detenuti è affetto da patologie, il 90 È con costoro - in numero sempre crescente - che coloro che servono lo Stato devono vivere. Aiutiamoli a vivere meglio, anche se il provvedimento è traumatico, anche se la scelta è traumatica, anche se la scelta mortifica attenzioni, attenzioni, aspirazioni, esigenze di larga parte della pubblica opinione. Credo che questo dovere il Parlamento ce l'abbia. Io, perlomeno, credo di averlo. *(Applausi

il clima che dovrebbe improntare i lavori del Senato. Ho, invece, ascoltato interventi che prescindevano dalle battaglie fatte da partiti o movimenti per attagliarsi a contestazioni su singole persone.

di amnistia o di indulto, comunque un provvedimento di clemenza, non potesse non essere inserito in una serie di provvedimenti che tenessero conto e mettessero in piedi una vera politica delle carceri, una vera politica per i detenuti. Chi vi parla, a differenza di tanti altri colleghi, è stato ad ascoltare le parole di Giovanni Paolo II quando al Parlamento in seduta comune ha chiesto alcune cose. Quindi, il mio approccio al problema è fatto tenendo conto di ciò

Anche accedendo al problema che abbiamo davanti tuttavia, da questo punto di vista vi sono però delle incongruenze sulle quali, signor Presidente, onorevoli colleghi e signor Ministro, bisogna fare chiarezza prima che il Senato si pronunci, essendo importante quello che il Senato farà oggi. Ho a mente l'intervista del senatore D'Ambrosio pubblicata questa mattina su "la Repubblica", che invito tutti i colleghi a leggere perché ancora sui numeri parlo di numeri - derivanti dall'adozione di questo importante provvedimento non c'è chiarezza. Come fa allora il legislatore ad intervenire se non vi è chiarezza sui numeri che derivano dal suo intervento? È un modo scorretto di porre i problemi, questo, o è un modo serio dire a tutti: pensiamo bene a quello che stiamo facendo?

tutti i procedimenti penali o c'è ancora spazio per aprirne altri? E se c'è ancora spazio per aprirne altri, non è ipotizzabile che, una volta approvato l'indulto, verremo probabilmente

InCommissione giustizia, ieri sera, mi è stato risposto che non c'è nessuno in carcere in conseguenza di questo reato. Ma allora, a maggior ragione, per dare completezza sistematica, se dobbiamo escludere i reati

nella democrazia piena la nostra battaglia, anche nelle fasi successive del dibattito. Senza enfatizzare, così come è stato fatto, abbiamo lasciato libertà di coscienza ai senatori dell'Italia dei Valori, perché quando parliamo di questo tipo di provvedimenti è naturale che ognuno

prima di adottare questo provvedimento. Come ho detto, vorremmo un altro tipo di indulto, non perché pensiamo che l'indulto risolva i problemi, ma perché pensiamo, avendo a mente quel che disse Giovanni Paolo II qualche tempo fa, che possa dare una mano, però - lo ribadisco - chiediamo al Senato di valutare bene, fino in fondo. Devo solo chiarire che, in Conferenza dei Capigruppo, ho acceduto a questi tempi perché ho un ruolo che va oltre l'Italia dei Valori: in Conferenza dei Capigruppo rappresentavo anche i senatori del Gruppo del ministro Mastella Mastella e i senatori a vita, e di fronte a nove senatori Capigruppo che chiedevano di avere questi tempi, sarebbe stato inelegante che mi fossi dissociato. Credo di avere agito secondo scienza e coscienza.

siamo chiamati ad approvare o respingere una proposta di indulto, cioè un provvedimento generale di clemenza, di fatto prevalentemente destinato ad operare, come tutti ben sappiamo, per lo sfoltimento della popolazione carceraria. Non siamo pregiudizialmente contrari all'indulto. Saremmo molto più convinti se le sue motivazioni fossero effettivamente riconducibili a solide ragioni di opportunità politica o di pacificazione sociale; meno entusiasmo nutriamo, invece, per l'uso strumentale, seppure ben comprensibile nel momento attuale, di questa leva quando è utilizzata al solo scopo di risolvere il problema del sovraffollamento dei nostri istituti penitenziari. E innegabile, invece, che questo provvedimento si renda oggi ineludibile e indifferibile per il fallimento del sistema di repressione del crimine, per la durata eccessiva dei processi, e ancor più per la tormentata esecuzione del giudicato penale. Lo Stato sembra quasi gettare la spugna, incapace a rendere giustizia in modo certo e soprattutto in tempi accettabili. Il processo dei benestanti è diventato supergarantito, mentre quello riservato ai non abbienti diventa spesso processo sommario, generando un'intollerabile discriminazione e una pesante emarginazione sociale. Ciò che turba particolarmente, poi, sono naturalmente i trattamenti non rispettosi della dignità umana e in aperto contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento, come quello dello scopo rieducativo della pena sancito dall'articolo 27 della Costituzione, in forza del quale «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». In un carcere in cui si vive in troppi, dove non si può lavorare, dove ci si ammala spesso e dove si diffondono le peggiori propensioni, la pena si trasforma e diventa ingiustamente afflittiva. Di fronte al collasso della giustizia penale abbiamo, però, il dovere di affrontare l'argomento in modo responsabile e trasparente, uscendo da logiche di scambio fra le forze politiche e soprattutto evitando un ulteriore premio per la criminalità politico-amministrativa già beneficiata da tante prescrizioni. L'estensione dell'indulto ai reati commessi fino al 2 maggio 2006 e l'innalzamento dello «sconto» di pena a tre anni, rispetto ai due originariamente stabiliti, rende a nostro modo di vedere discutibile la chiave di lettura di questa proposta: essa porterebbe alla scarcerazione di moltissimi detenuti, con un colpo di spugna di cui potrebbero beneficiare anche categorie di persone il cui operato ha rappresentato in questi ultimi anni un modello pesantemente negativo per la comunità. Mentre opportunamente rimangono esclusi dal provvedimento reati come associazione sovversiva, terrorismo, strage, associazione mafiosa, delitti contro i minori, violenza sessuale, tratta di persone, sequestro di persona, traffico e grande spaccio di stupefacenti, usura, avvertiamo preoccupazione nel vedervi ricompresi i reati finanziari e soprattutto quelli contro la pubblica amministrazione, come corruzione e concussione. A noi non interessano le situazioni personali di questo o di quel potenziale beneficiario. Questa proposta ci pare però essere un ulteriore differimento della soluzione reale dei problemi della giustizia: è tempo invece di porre mano ai problemi strutturali. La nostra coscienza, più che ragioni di calcolo politico, ci induce perciò a dare ascolto a chi, anche in Senato, portando esperienza professionale e indiscussa saggezza, propende per riforme più durature e radicali nel settore della giustizia, che non vanifichino *sic et simpliciter* anni di lavoro nell'accertamento della verità. Guardiamo perciò piuttosto con favore alla depenalizzazione di certi reati e a soluzioni stabili per i problemi della giustizia piuttosto che un indulto che non fa che rimandare in questo momento i problemi di fondo del settore e ci farebbe ritrovare daccapo fra pochi mesi. II dovere di ricreare oggi certezza nel diritto e nella giustizia ci impone di cercare vie diverse da quella oggi proposta. Per questi motivi, senza falsi moralismi e con meditata convinzione, esprimiamo la nostra preoccupazione per l'adozione del provvedimento in discussione e ci riserviamo di esprimere il nostro consenso dopo aver seguito il dibattito, sentite le considerazioni dei rappresentanti del Governo e anche a seguito dell'eventuale presentazione e accoglimento di ordini del giorno

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la situazione delle carceri è drammatica; drammaticamente note sono le cifre: 40.000 la capienza, 62.000 la presenza. Le carceri scoppiano e nelle condizioni materiali in cui vivono i detenuti svanisce la funzione rieducativa che la Costituzione assegna alla pena. All'affollamento delle carceri e al carattere della composizione sociale dei detenuti, per tanta parte imputati e condannati per reati di droga e per reati legati all'immigrazione clandestina, per tanta parte appartenenti ai settori più marginali della nostra società, hanno contribuito in questi anni leggi sbagliate, che hanno puntato essenzialmente ad un pesante inasprimento delle pene, senza accompagnarle ad un vero programma di recupero e al reinserimento sociale dei detenuti. È necessario, indispensabile, quindi, un atto di clemenza. Ma quando si affronta un tema così delicato come quello in discussione oggi, occorre capire anche quali sono gli argini, argini etici, innanzitutto, entro cui tale atto di clemenza debba essere collocato, perché dei tanti provvedimenti che vengono discussi in quest'Aula pochi interrogano, come quello in esame, l'idea del bene e del male, l'idea dell'etica. Portiamo in questa Aula tutte le nostre preoccupazioni; di due voglio dar conto nei pochi minuti che mi sono assegnati. La prima è la centralità della lotta alla mafia, è l'urgenza, l'impellenza di fare della lotta alla mafia una vera e propria priorità nazionale, di non dare nessun segnale di tolleranza, indulgenza, impunità per la mafia a quelle donne e quegli uomini che nel Mezzogiorno del nostro Paese lottano quotidianamente, senza clamore, con piccoli gesti, contro l'invadenza mafiosa e contro la paura. Penso ai sindaci coraggiosi che fanno saltare certe regole del gioco, penso a chi fa impresa senza piegarsi alle logiche del ricatto, penso a chi non accetta di scambiare la dignità della politica per un pugno di voti comprati alla mafia. La seconda è il rapporto tra etica e politica, un tema che ha cambiato il volto del nostro Paese. Sarebbe drammatico se il messaggio al Paese fosse che la classe politica compie quel che ci accingiamo a compiere, che dovrebbe essere un gesto di grande equilibrio e di grande responsabilità, per togliere dagli impicci qualche amico o amico degli amici. Se è vero che questo provvedimento, per quanto attiene alla corruzione, non libererebbe che poche decine di persone, ma aiuterebbe i colletti bianchi che già in carcere non sarebbero andati, ciò sarebbe gravissimo: significherebbe l'assunzione di quel modello di uso personale del potere politico che abbiamo tanto, fortemente combattuto. Noi rifiutiamo, per storia, cultura e impegno, l'idea che la politica possa essere occasione di vantaggio personale e rifiutiamo qualunque messaggio che tale idea possa avallare. Ci guida l'idea che la giustizia sociale non possa essere vera senza una giustizia giusta. Il duplice senso della parola "diritti" non si è costruito per caso: «diritti» come diritto di ciascuno; «diritti» come regole che governano un valore impalpabile, ma fondamentale, come quello della giustizia.

io abbia tentato di uccidere una persona. Ho preso un arma, l'ho caricata e ho sparato. La Provvidenza ci ha messo la mano e non ho raggiunto il risultato, ma ho sparato. La vittima ha subito delle lesioni. Ho commesso un reato grave: tentato omicidio con arma. Un reato per il quale i tribunali italiani, in media, danno sui nove anni di reclusione. Bene, se io fossi processato il giorno cui l'indulto, qualora venisse approvato - spero di no - dal Senato, entrerà in vigore, chiederei anzitutto di essere giudicato con il rito abbreviato: meno tre anni; siamo a sei anni di reclusione. Aggiungiamoci i tre anni dell'indulto e la mia pena effettiva scende a tre anni di reclusione; entro, cioè, non in carcere, ma nell'area dell'affidamento in prova al servizio sociale. Chiedo all'Assemblea, signor Presidente: tutto questo corrisponde a giustizia? Il problema non è solo l'indulto, ma è l'indulto inserito nel quadro dei benefici del codice penale, del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, la cui somma rende la sanzione penale qualcosa di virtuale. Noi non ignoriamo - e, anzi, siamo fortemente preoccupati - la situazione di congestionamento degli istituti di pena, ma siamo convinti che una situazione così problematica vada fronteggiata con interventi di carattere strutturale, non con misure di respiro cortissimo: potenziando l'edilizia penitenziaria, in linea con il lavoro svolto negli ultimi cinque anni; razionalizzando e rafforzando l'impiego della polizia penitenziaria e del personale di sostegno ai detenuti; aumentando i magistrati di sorveglianza; lavorando per un raccordo più efficace con la polizia giudiziaria, quando devono essere fornite le informazioni per le misure alternative alla detenzione; incrementando gli accordi con gli Stati di provenienza dei detenuti extracomunitari, al fine di far espiare la sanzione detentiva nei Paesi di origine. Se ci fosse stato tutto questo - lo dico in modo particolare al Ministro della giustizia - accompagnato dalla quantificazione, ad esempio nel Documento di programmazione economico-finanziaria, delle risorse da investire su tali fronti, avremmo anche potuto prendere in considerazione, ma a condizioni diverse da quelle di questo testo, un'ipotesi di respiro temporaneo per il mondo penitenziario. Ma queste condizioni non ci sono. Non le avete prospettate. C'è invece un provvedimento inaccettabile, che, per come è stato congegnato, avrà un solo effetto: elevare la soglia di criminosità. Non guardo nella sfera di cristallo; guardo all'esperienza maturata. L'ultimo indulto in Italia - è stato prima ricordato - risale al dicembre 1990 e condonava non tre, ma due anni di reclusione. Bene, nel 1989, un anno prima, i reati commessi in Italia ammontavano complessivamente a 1.348.333. Nel 1990, in aprile, c'è l'amnistia, e si crea una fortissima aspettativa per l'indulto, che arriverà a dicembre. Già questo fa balzare i reati complessivamente commessi a 1.642.159: 300.000 in più. Nel 1991, quando i beneficiati dall'indulto tornano in libertà, si sale a 1.741.280. Abbiamo la prova *a* *contrario* dell'effetto negativo dell'indulto. Negli anni successivi, infatti, quando l'effetto delle scarcerazioni si esaurisce e i recidivi che erano stati liberati con l'indulto tornano in carcere, il numero dei reati progressivamente decresce, fino ad arrivare, nel 1993, a 1.363.070, esattamente il punto di partenza del 1989. Ma in mezzo ci sono stati migliaia, migliaia e migliaia di reati

di cui pure avevamo richiesto la presenza - che valuti l'impatto del provvedimento in termini di sicurezza. Io rinnovo alla Presidenza del Senato la richiesta - siamo in tempo della presenza di un rappresentante del Viminale e di una relazione che ci dia la sua valutazione sul punto. Il ministro Amato non vuole venire adesso? Da qui dovrà passare, fra qualche mese, per rendere conto dei delitti che a seguito della messa in libertà torneranno a commettere ladri, rapinatori, estortori, omicidi e truffatori. *(Applausi dal Gruppo* *AN)*. In quel momento il problema sarà suo, non dei suoi colleghi Mastella o Di Pietro, anche perché, secondo elemento di oscurità, si è parlato di 12.000 detenuti in libertà. Dai dati del DAP, risalenti al 22 giugno 2006, coloro che hanno condanne residue fino a tre anni di reclusione risultano 24.001, e tralascio il dettaglio anno per anno. Su questa cifra complessiva va fatta la tara delle esclusioni che però non possono arrivare alla metà perché non riesco ad immaginare che ci siano 12.000 violentatori o terroristi nelle carceri italiane in questo momento. E tutto questo in cambio di quale vantaggio per la popolazione penitenziaria? Torno all'indulto del 1990:

Un anno dopo, nel dicembre 1991, 35.469. Questa è una ulteriore conferma dell'incremento della criminosità a seguito di provvedimenti di questo tipo. L'indulto che si vuole approvare è inaccettabile nella sua articolazione: lo ricordava prima l'ex guardasigilli Castelli. Tre anni è un dato senza precedenti,

con indagati in custodia cautelare che verranno immediatamente rimessi in libertà anche se il provvedimento non li riguarda direttamente. Quindi, esso avrà effetti ancor più gravi.

la modalità attraverso la quale l'usuraio direttamente o per interposta persona consegue i proventi della sua attività illecita. Per quale motivo non vi è nessuna eccezione nell'applicazione dell'indulto ai plurirecidivi?

Abbiamo presentato degli emendamenti in questo senso mi auguro che saranno presi in considerazione. Signor Presidente, è un provvedimento profondamente ingiusto. La sanzione penale è la componente più dolorosa del sistema giustizia, ma è garanzia di libertà. Io ho il diritto di comportarmi verso di te come tu hai il diritto di comportarti verso di me. Se questa simmetria nei comportamenti tra gli esseri umani viene rotta, l'assenza di giustizia non ha effetti soltanto nei confronti delle vittime, ma ha conseguenze sociali devastanti. Proprio perché la sanzione penale non è la ritorsione della vittima nei confronti del reo (era così in alcune società tribali dell'antichità), la sua assenza fomenta istinti di vendetta e di giustizia personale. Di più: aumenta la schizofrenia del nostro ordinamento penale, che si avvicina sempre più al mitico Saturno che si autoalimentava e divorava sé stesso. La fuga dalla sanzione definitiva, di cui questo indulto è un esempio, porta a cercare rimedi empirici estendendo in modo abnorme la carcerazione preventiva, spesso la sola effettivamente espiata. Ma ciò conduce fatalmente al sovraffollamento e alla tensione in carcere, cui si cerca di rimediare con l'indulgenza legislativa, che a sua volta porta ad un ulteriore aumento della carcerazione preventiva. La politica criminale, da pacata politica della ragione, diventa in questo modo agitata politica dell'espediente, della sopravvivenza giorno per giorno, quel tirare a campare che - chissà - ministro Mastella, forse, farà saldare a qualcuno qualche cambiale elettorale, ma non farà campare bene la gente. *(Applausi dal Gruppo AN).* Signor Presidente, queste sono le ragioni di contrarietà all'indulto e sono ragioni obiettive, non folcloristiche né strumentali. E vorrei tanto che almeno in questa Aula fosse risparmiato un argomento, tra i molti ascoltati in questi giorni, quello secondo cui con questo provvedimento si darebbe seguito all'esortazione del Santo Padre nell'Aula di Montecitorio nel novembre 2002. Colleghi e colleghe, non cerchiamo coperture pie ad un atto che di pio ha molto poco e che avrà certamente effetti empi, sia perché la risposta il Parlamento l'ha data con il cosiddetto indultino dell'estate 2003, sia perché, ogniqualvolta che la Chiesa è intervenuta sul tema, ha avuto cura di affiancare alla richiesta di clemenza la richiesta di garanzia della sicurezza pubblica (e questo indulto è la garanzia del contrario), sia perché è veramente singolare

il diritto alla vita all'essere umano innocente, una sanzione proporzionata al colpevole di gravi reati. Per questo, con le motivazioni fondate delle eccezioni che prima sono state illustrate, Alleanza nazionale voterà contro l'indulto.

Comunico che, per accordi intercorsi, la 10ª Commissione permanente è autorizzata sin d'ora a convocarsi per l'esame della richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di un componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. **Ripresa della discussione dei

Giovanni Paolo II, in un supremo atto di cristiana umiltà, si inginocchiò innanzi al Parlamento della Repubblica italiana e chiese un atto di clemenza, un segnale forte e deciso a favore di una comunità di sofferenti, uomini e donne, che hanno sbagliato ma che chiedono, in molti casi, la possibilità di redimersi e ai quali il Paese spesso ha dato il segnale di una punizione che a volte è contro perfino le norme che regolano il rispetto dei più elementari diritti umani. Il sovraffollamento delle carceri italiane ha ormai raggiunto un livello insostenibile: ogni 100 posti carcere vi sono 139 detenuti, il che rende irrealistico parlare di riabilitazione e perfino assolutamente impossibile parlare di recupero dei condannati a pene detentive. Al contrario, la condizione inumana e degradante della detenzione cozza con le Convenzioni internazionali e pesa sulla nostra coscienza come un macigno insostenibile. Signor Presidente, comprendo le ragioni dell'onorevole Di Pietro, *leader* di Italia dei Valori, che proviene da una cultura che non gli consente di guardare alle ragioni della coscienza contro quelle del mondo e delle radici da cui proviene. Ho un personale problema di coscienza, lo ammetto. Guardo alle ragioni di Giovanni Paolo II, guardo a quel supremo atto di umiltà dinanzi al Parlamento della Repubblica italiana, eppure comprendo Di Pietro che, dal mondo dal quale proviene, dalla cultura specifica dalla quale ha tratto fonte vitale per la sua azione politica, riceve sollecitazioni forti perché questo atto di clemenza, seppur perfino insufficiente provvedimento di indulto, non passi. Eppure io conosco le carceri, come le conoscono molti parlamentari che nell'ambito delle proprie funzioni le hanno girate; conosco il problema delle donne che hanno figli al di sotto dei tre anni, costrette a tenerli in quella umanità degradata, in quelle condizioni disumane; conosco le lettere, gli appelli dei detenuti, cui faceva riferimento la collega di Rifondazione Comunista che parlava addirittura di impossibilità di curarsi, di impossibilità di guardare alle minime condizioni di igiene, parlava, insomma, di uno scandalo che è sotto gli occhi di tutti. Che facciamo: consentiamo a qualche decina di migliaia di detenuti di ritornare in libertà, decongestionando le carceri italiane, oppure non diamo loro questa suprema possibilità di guardare al futuro con un minimo di speranza? Privilegiamo le ragioni dei corrotti, dei corruttori, degli imputati di voto di scambio, che pure rappresentano un problema serio e che usufruirebbero di questo provvedimento di indulto, oppure, per non fare, ci assumiamo la suprema responsabilità di dire di no? Onorevoli colleghi,

ma non dimentico, ad esempio, che un'intera classe politica è stata cancellata da quel voto di scambio che spesso poi, nelle aule di giustizia, ha trovato le corti indisponibili a proclamare sentenze di condanna. Mi regolerò con un atto di personale codardia politica, probabilmente, ma che guarda alle ragioni della mia coscienza più che a quelle della politica: mi asterrò, onorevoli colleghi,

Signor Presidente, onorevoli colleghi e amici di Topolinia e Paperopoli, come direbbe il commissario Basettoni, *alias* Di Pietro, parlando alla banda Bassotti, nell'immaginario collettivo, amnistia ed indulto risultano ancorati ad un atto di clemenza che il sovrano concedeva per ragioni particolari; spesso si riferivano ad eventi personali suoi e della sua famiglia. Addirittura, la fantasia popolare ritiene che l'elezione di un Pontefice o del Presidente della Repubblica rechi con sé, automaticamente, un provvedimento di amnistia o di indulto. In realtà, la cosa è assai diversa ed amnistia ed indulto sono diventati momenti di politica giudiziaria; hanno perso, cioè, la connotazione premiale, per diventare qualcosa di ontologicamente diverso. Dal 1989, cioè dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, i provvedimenti di amnistia e di indulto si sono riproposti con cadenza frequente in relazione al sovraffollamento delle carceri, destando, ovviamente, clamorose polemiche e nonostante le statistiche disastrose, qui ricordate proficuamente dal collega Mantovano. Quando le carceri esplodono, arriva con cronometrica puntualità la proposta di indulto ed amnistia, con un duplice obiettivo: svuotare le carceri, con tutto ciò che ne consegue (e parlo anche dell'emergenza sociale che si registrerà nel mese di agosto), e di mandare al macero quintali di fascicoli di procedimenti penali chiusi negli armadi impolverati delle procure, in attesa della prescrizione. Pochi si sono soffermati sul significato di redenzione, su quello di rieducazione e di reinserimento sociale del detenuto. Credo davvero che tutti possano sbagliare e che, commisurata allo sbaglio, ci debba stare una pena che va espiata con il preciso obiettivo della rieducazione. Non mi scandalizza uno Stato che costruisce un carcere in più, magari più accogliente, ma certamente non un albergo; non mi scandalizza affatto il detenuto che lavora, anzi, un po' per sé, per mantenersi e per non gravare sulle tasche dei cittadini, ma anche di questo non si è parlato. Mi scandalizza quello Stato che rinuncia alle proprie prerogative, ai propri poteri, quello Stato che, per un malinteso senso della pietà, rimette in circolazione, indistintamente, criminali incalliti insieme a poveri cristi, per i quali il recupero sociale non è solo un auspicio, ma è anche un dovere. Mi scandalizza quello Stato che tratta gli agenti della polizia penitenziaria quasi fossero dei reclusi e che non incentiva il lavoro dei volontari; uno Stato che applica uniformemente una misura di clemenza a prescindere dalla gravità del reato, arrivando a premiare anche l'omicida, perché nella trentina dei reati che avete escluso da questo indulto non vi è l'omicidio. Mi scandalizza un Governo che sostiene l'indulto senza presentare, parallelamente, provvedimenti utili a rimuovere le cause che determinano il sovraffollamento delle carceri. Con l'entrata in vigore del nuovo codice, che proponeva il rito accusatorio in luogo di quello inquisitorio del codice Rocco, si era detto, forse un po' affrettatamente, che mai più si sarebbe dovuto ricorrere a provvedimenti di amnistia e di indulto e invece, pur di arrivare a questo, qualche forza politica non ha esitato a strumentalizzare le parole di Giovanni Paolo II. Alleanza Nazionale crede che l'indulto rappresenti una sconfitta per lo Stato, che rinuncia a far scontare la pena che esso stesso ha inflitto a chi ha sbagliato. Crede anche che con una giustizia efficiente il problema non dovrebbe nemmeno porsi. Pensare di intervenire per legge su sentenze e condanne è un pericoloso atto di cannibalismo tra i poteri dello Stato: il potere politico e legislativo che va a fagocitare quello giudiziario.

mi rendevo conto che per ogni Caino difeso a spada tratta c'è un numero imprecisato di Abele che non chiede molto, ma solo giustizia e garanzia di una civile convivenza. La filosofia che caratterizza il vostro intervento è sostanzialmente la stessa che ispira il condono fiscale. Comodo, ma sostanzialmente immorale. Da uomo di destra, credo che amnistia e indulto rappresentino la spia di un malessere che colpisce la nostra giustizia e quindi lo Stato. Si sceglie la scorciatoia, piuttosto che affrontare organicamente i problemi della giustizia penale, con la riforma del processo penale, con le carceri nuove, con l'implementazione degli organici delle procure, della polizia penitenziaria, dei tribunali e così via. Dite che l'indulto sia la soluzione per i detenuti reclusi per questioni di droga. Certo, semmai per gli spacciatori che dal primo di agosto saranno liberi grazie a questo vostro indulto. La legge Fini sulle tossicodipendenze, infatti, non solo non prevede il carcere per chi assume sostanze, ma addirittura prevede percorsi terapeutici alternativi alternativi al carcere, in comunità di recupero, siano esse pubbliche o private, con il solo requisito dell'accreditamento. Cosa succederà ai detenuti extracomunitari che beneficeranno del provvedimento? Lo dico senza demagogia: saranno rimpatriati immediatamente? Resteranno in Italia con lo *status* di clandestini e con buone probabilità di tornare a delinquere? Cosa accadrà quando, tra qualche mese, la maggioranza dei detenuti graziati tornerà scientificamente (perché queste sono le statistiche) in carcere? Se i processi fossero più rapidi e non vi fosse la macchia vergognosa della carcerazione preventiva, se la giustizia fosse stata riformata, se tutti i magistrati lavorassero più serenamente, se l'edilizia carceraria si fosse evoluta diversamente e se lo Stato avesse lavorato ad un progetto rieducativo del detenuto, oggi non saremmo qui, nelle condizioni di dover difendere non solo la rispettabilità dello Stato, ma anche il diritto alla sicurezza della gente per bene

Se manteniamo un clima di maggiore silenzio questo ci permetterà di andare avanti anche più speditamente, oltre che di ascoltare gli oratori. Desidero rispondere ad un'affermazione che ha fatto il collega che mi ha preceduto e che peraltro stimo: stimo: difendere Caino non è contro Abele e probabilmente Abele avrebbe difeso Caino. Caino. È un ragionamento più complesso, che comunque spinge noi, democratici cristiani, a dare una valutazione

preminente), di quella popolazione carceraria a cui tutti hanno fatto riferimento. L'indulto costituisce una causa di estinzione della pena, secondo quanto previsto dall'articolo 174 del codice penale. codice penale. È un provvedimento di vera e propria clemenza dettato da ragioni tanto di opportunità politica quanto di pacificazione sociale. Lungo è stato il dibattito fin qui svolto, il quale tuttavia si è sempre concentrato su aspetti prettamente giuridici anche in ossequio al dettato della nostra Carta costituzionale e ai principi dell'ordinamento giudiziario. L'adozione di un provvedimento di clemenza costituisce oggi una necessità imposta dalla situazione in cui versano, da un lato, gli uffici giudiziari e, dall'altro, le carceri del nostro Paese, ma lo stesso costituisce non solo una misura giuridica amministrativa per tamponare delle emergenze generate dall'inefficienza della macchina giudiziario-processuale o dalle inimmaginabili carenze dell'edilizia penitenziaria, ma soprattutto un gesto di civiltà in un Paese con una profonda coscienza morale e religiosa come il nostro. il nostro. Come è possibile non ricordare il ruolo di primo piano svolto in questo contesto da Giovanni Paolo II durante il Giubileo, prima con quattro appelli rivolti al Governo, ai giudici, ai detenuti e al personale di polizia e successivamente con un discorso pronunciato in Parlamento, riunito in seduta comune durante la sua visita a Montecitorio? Da allora la situazione non ha potuto che peggiorare giungendo ai livelli critici attuali. È nota ormai ai più l'insostenibilità delle condizioni di detenzione e i ritardi della giustizia. Quello che i detenuti - ed ormai una gran parte della società civile -chiedono è un vero e e proprio atto di giustizia, che verrebbe a riparare parzialmente i delitti commessi dalle istituzioni che costringono degli esseri umani a vivere in una sorta di *lager*. Questo è purtroppo vero e dunque invito i parlamentari che ne hanno il diritto e l'opportunità a visitare

ma la tortura no. Questo provvedimento legislativo, pur essendo causa di forti e comprensibili divisioni nella società e tra le forze politiche, tuttavia costituisce un'importantissima occasione di cultura e civiltà. Per accrescere la sensibilità della società civile verso le problematiche legate al mondo carcerario, appartenenti a diversi orientamenti culturali, politici ed etici, laici, credenti e non credenti si trovano però uniti nel ritenere necessario ed urgente l'adozione di questo provvedimento in nome della giustizia e della ragionevolezza e nell'ottica di riforme di ampio respiro, soprattutto alla luce della notizia che l'Italia è il quintoStato per il numero di ricorsi

gridano vendetta per un Paese civile come riteniamo sia l'Italia. Sono dieci milioni i processi in attesa di giudizio, la cui durata media è di otto anni per i civili e di cinque per quelli penali, un numero che aumenta di anno in anno. Dal 2000 al 2005 più di un milione di processi sono stati annullati per prescrizione a causa della loro eccessiva durata, una vera e propria amnistia ufficiosa destinata alla fine ad ampliarsi. Molti di più sono tuttavia i reati che neanche vengono perseguiti. Giustamente i cittadini richiedono che colui che si macchia di un reato sconti la propria pena secondo le norme previste dal nostro ordinamento giudiziario, anche se non hanno una precisa consapevolezza delle condizioni in cui versano i detenuti nel nostro Paese nel 2006. La maggior parte delle strutture carcerarie attualmente presenti nel nostro territorio risale all'ottocento e non risulta assolutamente predisposta ad ospitare una tale mole di popolazione carceraria. Infatti, a fronte di una capacità di accoglienza di circa 43.000 unità, l'istituzione carceraria si trova a contenerne oltre 60.000 attualmente. È evidente poi una situazione di fatiscenza e di inadeguatezza degli istituti stessi, spesso ancora oggi privi di un semplice impianto di riscaldamento, come dicevo prima. Non è possibile, inoltre, ignorare che il sovrappopolamento e la promiscuità che ne deriva è anche causa di forme gravi di violenze personali tra i detenuti, che nulla hanno che fare con le pene previste dal codice penale. La coscienza civile del popolo italiano ha già da tempo compreso che la pena non deve costituire una vendetta, ma un percorso necessario di riabilitazione, da perseguire al fine di poter recuperare e restituire alla società coloro che hanno in qualche modo commesso un atto illegale, in modo particolare quando a delinquere sono dei giovani o dei giovanissimi. Ma com'è possibile seguire questo processo di riabilitazione, quando la stessa deve svolgersi in una situazione cronicamente sovraffollata e priva di strutture idonee? In una tale situazione, l'adozione di un provvedimento d'indulto non è in contraddizione con il reale significato della certezza della pena, soprattutto se, contestualmente, si manifestasse alla reale volontà di operare un'incisiva riforma che porti ad uno snellimento veloce delle procedure processuali, ad una seria programmazione in materia di edilizia penitenziaria e ad una seria ottimizzazione delle strutture attualmente esistenti. Queste misure così necessarie potrebbero essere avviate anche in collaborazione con il mondo privato, operando contestualmente un piano di recupero per gli edifici penitenziari posti nei centri delle grandi città, che tra l'altro traggono notevoli benefici economici dall'intero sistema che ruota intorno a queste realtà. Una società civile e forte come la nostra non deve temere il perdono, perché oramai è giunta ad un grado di maturità adeguata. La crisi della giustizia e del sistema penitenziario, così delineata, è una delle giù gravi questioni sociali del nostro Paese che colpisce direttamente milioni di persone e mina, essa stessa, il principio di legalità e certezza del diritto. È per tali ragioni che noi del Gruppo Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia riteniamo opportuno, per il bene dell'intero Paese, appoggiare il disegno di legge oggi in discussione.

sono d'accordo sulla necessità e l'urgenza di un provvedimento di clemenza che allevi la disumanità della condizione delle carceri. Sono tra quanti, nell'Aula di Montecitorio, all'invito pressante rivoltoci in tal senso, da Giovanni Paolo II. Considero, non le parole del Papa, senatore Mantovano (e mi fa piacere incontrarla per un volta sul terreno della laicità e della distinzione, che non è separazione, tra fede e politica), ma quel nostro applauso, un applauso corale e convinto di tutta l'Aula di Montecitorio, un impegno d'onore che certo non coinvolge il Parlamento nel suo complesso, ma coinvolge, sicuramente, la mia persona. Del resto, per quanto mi riguarda, l'applauso all'invito del Papa non fu motivato da una generica sensibilità umanitaria, ma da una precisa ragione costituzionale: la nostra Costituzione vieta pene contrarie al senso di umanità e prescrive che la pena debba essere finalizzata al recupero sociale del reo. Il nostro sistema penitenziario, che pure ha interiorizzato nel suo personale questa cultura nuova, questa cultura della Costituzione, non è oggettivamente in grado di corrispondere al vincolo che la Costituzione pone. Non è in grado di farlo per la scarsità delle risorse, in particolare quelle destinate a finanziare il lavoro in carcere, e non è in grado di farlo anche per il sovraffollamento, che ha raggiunto livelli insopportabili, come chiunque di noi abbia visitato un carcere ha potuto constatare di persona. Tuttavia, colleghi senatori, noi non possiamo ignorare o anche solo sottovalutare l'impatto che un provvedimento necessario e difficile come questo avrà sull'opinione pubblica. Un'opinione pubblica che appare oggi frastornata e inquieta, preoccupata per l'impatto di questo atto di clemenza sulla sicurezza pubblica e sulla questione morale. Abbiamo il dovere di considerare con attenzione tale inquietudine, se non vogliamo che i timori diffusi nella nostra società siano cavalcati in modo inaccettabile - perché strumentale e demagogico - da esponenti sia della maggioranza, sia dell'opposizione. Chiedo a quest'Aula, quindi, un supplemento di lavoro, per migliorare il provvedimento nella direzione auspicata, con argomentazioni pacate e ragionevoli, da molti nostri autorevoli colleghi. È dall'esito di questa verifica e da quello della valutazione di gruppo sui suoi risultati che farò dipendere il segno del mio voto. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, l'Italia dei Valori è sempre stata favorevole ad un provvedimento di clemenza, ma ad un provvedimento di clemenza che, di pari passo, affrontasse anche la riforma del sistema giudiziario. Sappiamo bene che esiste il problema contingente dello svuotamento delle strutture carcerarie, ma sappiamo anche che nel giro di cinque o sei mesi il problema si ripresenterà. Si è voluta, invece, percorrere la via dell'urgenza perché, evidentemente, si ha più facilità a coprire accordi che poco hanno a che vedere con quell'atto di clemenza che non solo noi dell'Italia dei Valori vogliamo. Si rischia di dare ragione a quel proverbio che ci ricorda che la gatta frettolosa fece i gattini ciechi. I nostri colleghi deputati ci hanno inviato un indulto che è un insulto: un insulto alla gente onesta; un insulto ai piccoli risparmiatori; un insulto ai taglieggiati; un insulto che non riesco ad avallare e, soprattutto, a giustificare presso i miei elettori (sì, colleghi, a chi mi ha espresso il proprio consenso a rappresentarlo nella massima istituzione dello Stato e, quindi, mi permette di parlarvi in questo momento). Comprendo che, grazie a quella scellerata legge elettorale, gran parte di noi debba rendere conto soltanto ai capi che li hanno nominati e non ai cittadini elettori, ma dovremmo farne un problema di coscienza. Spero vivamente che le coscienze di tutti noi si ribellino a questo scandaloso accordo, che ha incluso nel provvedimento di indulto reati come il voto di scambio mafioso, i reati finanziari e contro la pubblica amministrazione, gli estortori, i delinquenti abituali. Il Presidente del Consiglio del precedente Governo e i suoi alleati per ben cinque anni hanno tentato di dare un colpo di spugna come questo, ma non vi sono riusciti: mi sembra veramente singolare che l'Unione stia proseguendo con quella politica dei provvedimenti legislativi personalizzati. Voglio, quindi, concludere il mio intervento affinché in questo ramo del Parlamento vi si metta riparo, approvando quegli emendamenti tesi ad escludere dall'indulto i reati che certamente non contribuiscono allo svuotamento delle carceri, ma rispetto ai quali sarà estremamente difficile giustificarsi con la stragrande maggioranza del popolo italiano.

Lega Nord Padania è contrario a qualunque provvedimento di clemenza generalizzata, perché ritiene che ciò contrasti con i sacrosanti principi dello Stato di diritto. Nel caso dell'indulto, ad esempio, viene violato il principio della certezza della pena, senza contare, poi, che la liberazione di certi criminali mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini. La sinistra sostiene che l'indulto serve ad abbattere il sovraffollamento carcerario, ma non si può scaricare tale problema sui cittadini onesti e sulle vittime dei reati.

luogo, facendo in modo che i detenuti extracomunitari - popolazione ormai maggioritaria in queste strutture - scontino la pena nei propri Paesi di origine. Apro e chiudo una parentesi, signor Presidente: con tutti i delinquenti che già vi sono in Italia, non vedo perché se ne debba importare un numero ancora maggiore e gratuitamente. L'indulto è solo un colpo di spugna che offende le vittime dei reati per la seconda volta. contrariamente a quanto affermato da qualche collega, non è certamente un partito che non si interessa delle condizioni di vita dei carcerati. Se dobbiamo scegliere, però, stiamo dalla parte di Abele, non dalla parte di Caino. A questo proposito, vorrei stigmatizzare l'atteggiamento del ministro Di Pietro *(Applausi del senatore Amato)*, che sta portando avanti la battaglia per escludere corruttori e responsabili di reati finanziari dall'indulto, ma solo per una sua visibilità personale. Anche la Lega Nord la pensa come il ministro Di Pietro sui reati finanziari, ma ovviamente ci preoccupa di più il fatto che questo provvedimento possa rimettere in libertà anche degli assassini e dei rapinatori. Questi sono i reati che destano il maggiore allarme sociale. Infatti, se per i reati finanziarsi si parla di un numero di detenuti che può variare dai 70 ai 300, i condannati per omicidio che usufruirebbero dello sconto di pena sono ben 6.952, mentre i condannati per furto a cui si applicherebbe l'indulto sono invece 2.148; sono dati ufficiali. Senz'altro fa pensare questa sinistra con un Bertinotti presidente della Camera dei deputati che fa di tutto per calendarizzare l'indulto in Aula. Mi chiedo: ma Rifondazione Comunista non poteva pensare a qualcos'altro? Fa certamente sorridere vedere come quelli che si sono posti come i principali sostenitori delle battaglie morali adesso facciano melina e se ne stiano zitti per fare passare il provvedimento. Sulla coerenza dei partiti dell'Unione potremmo scrivere pagine e pagine di storia politica. Ormai, sono un'armata Brancaleone allo sbando in cui ognuno, per giunta, è alla ricerca del suo momento di visibilità. Altro che Ministro che attenta alle istituzioni, collega Salvi; questo è un Governo non credibile. Che dire dell'attuale opposizione? L'opposizione è divisa su questo argomento specifico, ma non c'è niente di nuovo. Anche in passato, infatti, Forza Italia e UDC erano state più possibiliste, mentre la Lega Nord e Alleanza Nazionale sono sempre state fermamente contrarie. In Parlamento è stato trovato un accordo trasversale che, però, non ha cambiato di una virgola la posizione della Lega Nord. Noi vogliamo che chi commette dei reati espii la sua colpa fino in fondo e risarcisca il suo debito con la società. Ribadisco che questo non significa essere disumani; significa semplicemente assicurare il rispetto del principio fondamentale del diritto per cui chiunque viene condannato deve sopportare una pena. Se così non fosse, signor Presidente, l'effetto di deterrenza della sanzione

Governo. Lo ripresentiamo in questo ramo del Parlamento perché pensiamo, in questo modo, di rafforzare ulteriormente l'azione del Governo. riguarda quelle persone che hanno scontato la pena per provvedimenti di condanna per corruzione o speculazione finanziaria e che potrebbero tornare a godere dei grandi patrimoni e delle ingenti ricchezze accumulate illegalmente. Riteniamo si debba intervenire perché i beni confiscati ai colpevoli dei reati di corruzione seguano la normativa oggi in vigore per i beni confiscati agli appartenenti alle organizzazioni mafiose. il dispositivo che proponiamo prevede la necessità di approvare entro settembre un adeguato provvedimento di sequestro e confisca dei beni per coloro che abbiano subito provvedimenti di condanna per corruzione o per reati finanziari e che questi stessi beni siano destinati ad un uso collettivo e sociale. Questo è il dispositivo che proponiamo

Signor Presidente, sono grata - e credo che tutti, in quest'Aula, dovremmo esserlo - alla collega Olimpia Vano che ha voluto dar voce qui a chi vive il carcere: uomini e donne che perdono identità, la cui storia e le cui vicende sono dimenticate e annullate perché diventano numeri, tipologie di reati. Noi ne parliamo troppo spesso in questi termini astratti, dimenticando che, con in particolare riguardo a una decisione come quella dell'indulto, essa ha effetti sulle vite concrete di donne e uomini, di cui noi - intendo proprio noi istituzioni - siamo responsabili in modo del tutto particolare, perché decidiamo direttamente delle condizioni in cui vivono. Se il carcere è degrado, afflizione, negazione nei fatti di diritti e dignità dell'essere umano e delle persone, se queste sono pene aggiuntive che infliggiamo perché le carceri strutturalmente non sono in grado di garantire la dignità e il rispetto dei diritti di chi è detenuto, noi ne siamo responsabili direttamente, per scelta o per omissione,

Tengo conto - ma non è su questo che mi voglio soffermare - che questa campagna è stata alimentata dalla disinformazione e da falsità volute e precise

tale campagna è stata favorita dalla condizione di lungo periodo, che si è resa più acuta in anni recenti, in cui la giustizia ha vissuto nel nostro Paese: troppe e troppo diffuse le condizioni di illegalità per alcuni reati, troppa e troppo diffusa è l'impunità, specialmente per quelli che vengono definiti i «soggetti forti». Penso ai reati contro la pubblica amministrazione e a tutto l'intreccio tra politica e affari. Ciò ha fatto dimenticare che in questi anni abbiamo vissuto anche un'altra vicenda, un'altra tendenza che è decisiva per la giustizia,

di ricorso forte al penale. Si sono citate molto spesso in questi giorni, in quest'Aula e anche alla Camera dei deputati, l'immigrazione e la tossicodipendenza. Più in generale, penso che vi sia vasta area di soggetti sociali, di conflitti, condizioni e bisogni che vengono stigmatizzati come devianti, come incapaci e impossibili di inserimento nella società e che quindi devono essere tenuti sotto controllo È una tendenza che scarica sui più deboli, sugli emarginati, spesso sui giovani, più sui giovani, anche un problema che che qui è stato più volte richiamato, quello del modo in cui una società riesce a coniugare giustizia, sicurezza e riconoscimento reciproco, nell'ordine delle norme, nel rispetto delle norme. C'è una paura e una insicurezza diffusa che non ha origine da una diffusione del crimine, ma dalla crisi del legame sociale, dalla difficoltà sempre maggiore a riconoscersi nelle differenze e quindi stimola ad una difesa della della propria condizione di presunta normalità e a ricacciare tutti coloro che non corrispondono a questo carattere, a questa fisionomia, emarginandoli e criminalizzandoli. Io sono tra coloro che pensano non soltanto che il carcere non è la risposta, ma che il penale non ha le risposte ai problemi sociali, alle condizioni e ai bisogni di larga parte della popolazione. Penso che questa risposta produca soltanto esasperazione; non soltanto sofferenza, ma esasperazione dei problemi della società. Penso, certo, che l'indulto non è la risposta a questi problemi, che le risposte sono altre, come molti hanno detto, sono quelle strutturali. Sono tuttavia convinta che l'indulto sia un primo passo indispensabile per affrontare una politica di riforme strutturali, di cambiamento delle leggi, come di cambiamento degli indirizzi dell'amministrazione della giustizia, nella direzione giusta. In questo senso, certo, l'indulto è un intervento, una risposta di emergenza ad una condizione di emergenza. Condivido, però, quanto ha detto il sottosegretario Manconi ieri in Commissione giustizia: questo provvedimento è il primo passo indispensabile senza il quale la politica delle riforme non può decollare. Sono convinta, cioè, che il richiamo alle riforme strutturali, che molti che sono contrari a questo provvedimento fanno, vada assolutamente rovesciato. Mi ha confortato, leggere un intervento del magistrato Caselli, che non mi pare sia imputabile di lassismo, di tolleranza rispetto ai reati, ai crimini, che considera l'indulto il motore di avviamento per questa politica di Teniamo conto - altri lo hanno detto - che è dal 1990 che un provvedimento di questo tipo non viene adottato e che quindi non siamo certo di fronte ad un regime di ricorso facile, inflazionato, all'indulto. Si è anche detto, nel corso della campagna sui giornali e nell'opinione pubblica, che la motivazione di questo indulto non è la clemenza e nemmeno lo sfollamento delle carceri, ma piuttosto la ricerca di un accordo sottobanco. Si è parlato di

ha imposto proprio per limitare il ricorso all'indulto. Infatti, perché il Parlamento adotti questo provvedimento è richiesta una maggioranza ampia, un accordo ampio e quindi una convergenza tra forze politiche differenti, tra forze politiche della maggioranza e dell'opposizione. Un accordo, una convergenza, tesi a sottrarre la decisione di questa scelta e la modalità concreta con cui è adottata a ragioni di opportunità, sia nel merito specifico che nella decisione stessa, che possono dipendere da valutazioni politiche, da convenienze politiche della collocazione di maggioranza e di opposizione. Penso che questo accordo sia stato trasparente, politico e abbia prodotto un equilibrio proprio nei punti che più vengono discussi, cioè quello della definizione dei tre anni

devono essere inevitabilmente eccezionali; l'esclusione è una scelta delicata, rischia di minare il principio costituzionale della parità di trattamento. le esclusioni devono essere eccezionali. Mafia, terrorismo, reati sessuali, reati contro i minori, reati di traffico della droga: queste sono le esclusioni che il provvedimento prevede.

possibilità di applicazione, nella sua stessa natura non affronta minimamente il vero cuore del rapporto tra mafia e politica, che non sono i soldi dati al mafioso, ma lo scambio di favori che il politico può avere con il mafioso. Così come per i reati

con una formula di chiusura: esso produrrà notti meno sicure per moltissimi cittadini italiani. Veniamo allora ad analizzare i benefici che produrrebbe. primo luogo, le indagini in corso in ogni caso si dovrebbero condurre e i processi in corso si dovrebbero in ogni caso celebrare. Sembrerebbe, ministro Mastella, un gioco virtuale, nel senso che nelle aule e nei tribunali bisognerà continuare a lavorare pur sapendo che alla fine quelle pene non verranno scontate.

demotivati, demoralizzati, mortificati? Non c'è dubbio che sapere di lavorare a vuoto non è una grande soddisfazione. Ministro, illustri dottrinari si sono spinti fino a elaborare quella che viene definita la teoria economica del reato, ossia il calcolo che compie un reo, o potenziale reo, prima di commettere un reato. Egli fa un calcolo anche di convenienza economica: mi conviene comportarmi in modo lecito o illecito? Si opta per la seconda scelta quando una serie di requisiti danno un segnale positivo. Quali possibilità ho di essere preso nel momento in cui commetto un reato? E questo è un problema di polizia, di organizzazione del sistema di sicurezza. Quali possibilità, in seconda battuta, ho di essere portato a giudizio, cioè di essere assicurato e di avere poi un giusto processo? Terzo, quali possibilità ho di essere condannato? E questo tocca il sistema della giustizia: l'elaborazione delle prove, il confezionamento di un castello accusatorio sufficiente per arrivare ad una condanna. abbiamo letto delle statistiche, in base alle quali 96 reati su 100, nella fattispecie il furto, non vengono nemmeno assicurati alla giustizia; cioè, il sistema

è un incentivo, sostanzialmente, a comportarsi in modo non lecito. Se andiamo poi a verificare le possibilità di avere un giudizio e un sistema di elaborazione di prove non sufficienti per condannarlo, capite che da quel 96 passeremo ad un 97-98 per cento;

daremo anche la possibilità - nonostante essere stati presi, assicurati alla giustizia e aver subito una condanna - di non scontare la pena. Di questo trattasi nel provvedimento

Allora, questo provvedimento dovrebbe interessare circa 10.000 detenuti, o comunque processandi, dei quali 5.000 o più, sembrano essere extracomunitari. Ministro di "grazia" Mastella, vi siete preoccupati di capire dove andranno, se li rilasciate, questi 5.000 extracomunitari? Finiranno tutti per strada, non v'è dubbio. Non hanno una lira in tasca, non v'è dubbio. Non hanno una casa, non v'è dubbio. In quanti giorni, settimane o mesi questi ritorneranno nelle carceri che avete aperto? E alle vittime? Nessuno si è preoccupato di spendere mezza parola per chi tutti questi delitti li ha dovuti subire. Penso alle vittime passate, ma anche a quelle future, perché, con questa gente in strada, ci saranno vittime potenziali da calcolare. Per questi motivi, che a noi sembrano non ideologici, politici o partigiani, ma estremamente razionali, non potremmo dire che questa che la resa dello Stato di fronte ai pochi che riesce a pizzicare e a condannare può andare bene. Dovendo scegliere tra Caino e Abele, noi sceglieremo sempre Abele. Ministro Di Pietro, assente, noi chiediamo alle persone adulte, o ci è richiesto dalla nostra società, di decidere e di non stare nel vago. Non si può si può approvare, stando al Governo, un provvedimento e mandare i propri sostenitori in piazza a manifestare contro il provvedimento che lei stesso propugna, in quanto facente parte del Governo. Bisogna decidere da quale parte stare; gli uomini adulti e grandi sanno prendere delle decisioni adeguate.

Alleanza Nazionale non è contraria per principio ad un atto di clemenza, non è contraria per principio all'indulto. Alleanza Nazionale è contraria a questo provvedimento, perché esso non è accompagnato da quelle misure strutturali che soltanto sarebbero in grado di poterlo giustificare agli occhi

questo provvedimento non ha il consenso della stragrande maggioranza dei cittadini italiani. Di quelle persone che vivono, lavorano tutti i giorni, faticano a guadagnarsi da vivere e che chiedono che chi sbaglia, chi viene processato, chi viene condannato debba espiare la propria pena. Noi siamo certamente favorevoli a che la pena abbia anche una funzione rieducativa, ma siamo anche convinti che non c'è rieducazione se prima non c'è l'espiazione della condanna che ci si è meritati con il proprio comportamento illecito.

di dare il loro voto favorevole a questo provvedimento e ringrazio l'onorevole Mantovano di avere chiarito, senza ombra di dubbio, che la posizione di AN è contraria e che coloro che voteranno a favore lo faranno esclusivamente a titolo personale. Come dicevo, molti di coloro che voteranno a favore di questo provvedimento lo faranno in nome di un certo umanitarismo. Cari colleghi, dopo le false liberalizzazioni dopo la falsa fiducia che si è votata l'altro giorno in questa Aula, siamo arrivati al falso umanitarismo. Sapete tutti benissimo che dopo pochi mesi queste migliaia di disperati, che voi liberate sì dal carcere oggi, ma di cui vi dimenticate da domani, torneranno a delinquere e quindi in carcere. Nei loro confronti, tra tra l'altro, questo indulto sarà revocato perché è previsto che chi commette altri reati nei prossimi cinque anni subirà la revoca del

tutto il rispetto nei confronti dei carcerati che soffrono nella loro condizione; tutto il rispetto per chi deve vivere una condizione umana certamente difficile; tutto il rispetto per coloro fra voi che hanno voluto dare voce a chi vive questa condizione difficile nel carcere. Ma non si può abdicare al principio della certezza della pena in nome di queste considerazioni. Soprattutto, non si può accettare che per liberare alcune migliaia di detenuti

Questo è un dato di fatto che non può essere dimenticato. Se esistono ragioni umanitarie nei confronti dei detenuti, devono esistere altrettante e più valide ragioni umanitarie nei confronti delle centinaia di migliaia di vittime dei reati, alle quali in questa Aula nessuno ha rivolto un solo pensiero. Dunque, non c'è nulla di più politico di un provvedimento come questo e non capisco come si possa invocare

fra due situazioni che vedono, da un lato, i delinquenti in condizioni umane difficili ma che sono in carcere e, dall'altro, il popolo italiano che nei prossimi mesi, a causa di questo provvedimento, subirà certamente

e noi questo non lo possiamo consentire rimanendo in silenzio. Un indulto di tre anni, come mai era stato votato nell'intera storia della Repubblica italiana. Già altri lo hanno fatto, ma anche io voglio sottolineare questo aspetto: mai prima nella storia della Repubblica si era votato un indulto di queste dimensioni sproporzionate anche rispetto ai numeri precedenti legislativi. Una sproporzione di cui vi siete resi conto anche voi perché, da un lato, si concede un indulto di tre anni, ma, dall'altro, si prevede una serie infinita di esclusioni e di eccezioni che fa capire come

Non si riesce a capire in base a quale logica si arriva a questa esclusione, ma, guarda caso, il delitto che colpisce la vita umana, l'omicidio volontario, non è escluso L'indulto si applicherà dunque anche agli assassini e, facendo un rapido conto tra rito abbreviato, attenuanti generiche, affidamento in prova al servizio sociale e sconti

sentiamo il peso della responsabilità del dover rendere conto ad un Paese che ci guarda e nello stesso tempo ci rendiamo conto che, qualunque sia la nostra decisione, chiaramente

un problema per i cittadini comuni che non hanno garanzia del rispetto dei loro diritti nei nostri Tribunali in tempi ragionevoli e non hanno garanzia del risarcimento, di quei comportamenti che colpiscono i loro interessi, la loro persona e il loro patrimonio. Abbiamo procedimenti lunghi per i quali siamo sottoposti a sanzioni di condanna anche in sede europea. Nonostante le nostre carceri siano affollate a dismisura i nostri cittadini non hanno il senso della certezza del diritto e della certezza della pena. Dobbiamo incidere in modo efficace nella struttura del nostro sistema giudiziario, oppure questo Stato abdica ad un suo dovere fondamentale. Passatemi il paragone: si può anche delegare ad altri, al privato, la gestione della sanità - questa parte politica non lo condivide, però in teoria e in astratto si può fare ma uno Stato non può delegare ad altri la certezza del diritto e la realizzazione della giustizia. Quando uno Stato non dà certezza del diritto e non dà giustizia non è più riconosciuto come tale dal cittadino. allora che questo Parlamento ed il Governo si occupino di giustizia, ma della giustizia che interessa ai cittadini, e quanto prima,

Abbiamo bisogno di ripristinare la legalità costituzionale: lo Stato devo essere il primo a rispettare la Costituzione: la deve rispettare nel garantire la certezza del diritto e dare sicurezza ai cittadini, la deve rispettare nel rendere umana l'espiazione delle pene. quello di oggi non è neppure un provvedimento di clemenza: viene anzi visto come un provvedimento necessario anche da chi ne usufruirà, un provvedimento necessario per uno Stato che non sa fare la sua parte. I provvedimenti di clemenza hanno altra *ratio*: hanno la *ratio* di recuperare alla vita sociale, con un atto umanitario e di clemenza, chi in questa società ha sbagliato. Noi oggi invece, molto probabilmente, adotteremo un provvedimento

come una sorta di avallo morale alla scelta difficile che oggi ci apprestiamo a compiere. C'è chi in quest'Aula c'era e lo ha applaudito: per questo si senta investito della responsabilità di essere coerente con quell'applauso. Io non c'ero, però c'è chi c'era ed ha applaudito. Ebbene, il Pontefice ha chiesto la clemenza, ma ha anche chiesto che ciò avvenga senza compromettere la necessaria tutela della sicurezza dei cittadini. Abbiamo presentato quindi un ordine del giorno aver riassunto quanto ho appena detto, cioè quale sia il gravissimo stato della crisi strutturale della nostra giustizia, al punto che i cittadini, nonostante le nostre carceri siano piene, non percepiscono la certezza del diritto e della pena, diritto e della pena, impegniamo il Governo: «in sede di attuazione del provvedimento di indulto, ad impartire tempestivamente le opportune direttive alle Prefetture, al fine di garantire il mantenimento della sicurezza sul territorio e di realizzare il necessario coordinamento con gli enti locali, volto a monitorare l'effetto creato dall'indulto sul territorio, ad accogliere nel sociale pubblico e privato chi ne manifesta la necessità, assistendo i singoli detenuti in un percorso di recupero attraverso la formazione e l'avvio al lavoro; a reperire fondi straordinari per far fronte alle necessità sopraindicate e ad utilizzare l'occasione straordinaria ed eccezionale dell'indulto per riorganizzare effettivamente il sistema penitenziario, ampliando e migliorando l'edilizia carceraria e dando nuova funzionalità all'organizzazione complessiva del sistema penitenziario, dotandola delle risorse finanziarie ed umane necessarie».

e, soprattutto, perché esso sia l'inizio di un coraggioso impegno del Governo e del Parlamento ad affrontare il nodo della giustizia, nodo che io ritengo cruciale per la credibilità dello Stato nei confronti dei cittadini che ci hanno votato.

tutti, avvertiamo il senso della responsabilità che assumiamo in nome dei cittadini, ai quali dobbiamo rispondere. Ma quando lo Stato non è in grado di garantire ai cittadini, a tutti cittadini, dunque anche a quelli che vivono il dramma della privazione della libertà, condizioni di vita decorose e rispondenti ai principi di umanità, ebbene lo Stato ha l'obbligo di intervenire con l'adozione di misure eccezionali. L'eccezionalità della situazione carceraria nel nostro Paese è fatto ineludibile. Basta considerare i dati numerici per avere la cifra del disagio profondo, delle condizioni spaventose in cui si dibatte la popolazione carceraria. Il Gruppo di Forza Italia voterà a favore del provvedimento d'indulto, ma ciò non significa che Forza Italia sia dalla parte dei delinquenti. Significa sicuramente che noi riconosciamo anche a costoro i diritti che competono a ciascun componente del genere umano. Su una materia così importante sarebbe opportuno non lasciare spazio alla demagogia e alle divisioni ideologiche, spesso pretestuose. Siamo dinanzi ad un evidente stato di necessità, che impone decisioni immediate, non procrastinabili all'esito di un dibattito più articolato, anche a costo di mortificare le prerogative dei due rami del Parlamento. Qualcuno, onorevoli colleghi, dica finalmente al ministro «congelato» che la campagna elettorale è finita. Ormai anch'egli è solo, visto che l'onorevole Gasparrini voterà a favore del provvedimento d'indulto e che il senatore De Gregorio provvederà ad astenersi sullo stesso. Qualcuno gli dica che la campagna elettorale è finita e che le battaglie demagogiche non si conducono sulla pelle dei cittadini, anche di quelli che soffrono comunque a cagione delle loro condotte antigiuridiche. Qualcuno dica al dioscuro del giustizialismo più becero che è ora di chiudere con un passato difficile da sradicare, quel passato che ha prodotto lacerazioni profonde tra gli opposti schieramenti. Il provvedimento che oggi ci accingiamo ad approvare probabilmente - me lo auguro - consentirà la ripresa del libero e democratico confronto politico, ricondotto nelle Aule del Parlamento e nei luoghi della politica, finalmente sottratto all'innaturale luogo delle aule giudiziarie, dove per anni è stato strumentalmente trascinato. Nel nostro Paese, colleghi, assistiamo alla violazione costante del principio costituzionale dell'articolo 27, che reca in maniera inequivoca le finalità della sanzione penale. La Costituzione ci indica una pena che tenda alla rieducazione e al recupero del condannato. Afferma, nel contempo, che occorrono strutture, spazi, luoghi; occorre il lavoro, l'istruzione, le attività fisiche: tutto ciò di cui un uomo libero o in ceppi ha bisogno per condurre una vita dignitosa. Occorrono le strutture che dopo l'espiazione restituiscano alla società un uomo migliore. Oggi i nostri istituti carcerari non rispondono ad alcuna delle esigenze indicate e offendono profondamente il concetto di umanità della pena. Il senso di umanità può acquietarsi soltanto nell'acquisita certezza del rispetto di cui ogni uomo gode anche nel momento in cui è nella polvere. Il sovraffollamento è un dato allarmante. Certo, sarebbe stato meglio affrontare per tempo il problema, ma oggi non abbiamo più il tempo per costruire nuove carceri, per ristrutturare quelle esistenti, per operare una forte depenalizzazione, affinché non tutte le controversie sociali siano devolute alla magistratura penale. Non si può far tutto in tempi rapidi. Allora l'emergenza va affrontata con decisione e coraggio, anche a rischio di quella impopolarità che un provvedimento del genere può evocare. Nessuno è esente da responsabilità. Si tratta di una situazione che l'Italia vive da sempre. Approvando l'indulto consentiamo e diamo attuazione a un principio costituzionale, poiché esso è lo strumento che la Costituzione ha preso in considerazione per una finalità precisa, quale momento di riequilibrio dei valori in discussione, laddove si versi in una situazione d'emergenza. Non è solo strumento di deflazione carceraria, di sfollamento di un sistema al collasso: sarebbe troppo semplice questa visione dell'istituto. È un provvedimento che serve ad uniformare il tempo della detenzione e a renderlo accettabile. Il tempo - voi sapete - è diverso se il trattamento carcerario risponde ai principi di umanità della pena. Tutto ciò non significa che siamo solo dalla parte dei delinquenti. Siamo per una pena che non sia solo sinonimo di vendetta, nell'ovvia necessità di bilanciamento degli interessi in gioco. Certamente, colleghi, il provvedimento non è immune da difetti evidenti. Il primo per la prima volta questo provvedimento non è accompagnato da un provvedimento di amnistia, nonostante tutte le proposte di legge recassero la previsione dell'amnistia. soltanto al sovraffollamento carcerario, senza tenere in debito conto il carico di processi pendenti (dieci milioni), che costituisce forse il problema principale. Non si è avuto il coraggio di prevedere l'amnistia, lasciando l'estinzione del reato nel demanio delle procure, le quali, nella previsione della pseudo-obbligatorietà dell'azione penale, decidono quali sono i processi ai quali dare priorità e quali quelli da lasciare su un binario morto perché vi provveda la prescrizione. E ancora, il secondo motivo di doglianza da parte nostra. Si opera l'esclusione delle pene accessorie dimenticando che per legge molte delle pene accessorie seguono la pena principale. Quindi, è un fatto assolutamente specioso e privo di alcun fondamento serio, indice di fortissima confusione. Avremmo comunque preferito votare un provvedimento complessivo più giusto e più completo. Allora chiediamo che la maggioranza si ponga subito il problema dell'amnistia e, a seguire, la questione della risoluzione dei problemi strutturali e di quelli attinenti alla necessità di adeguamento dei principi di diritto sostanziale e processuale alle nuove e mutate esigenze della collettività. Il sistema penale è la cartina di tornasole della civiltà di un popolo. Non penso che oggi il nostro Paese sia in condizione di rivendicare il ruolo di culla del diritto e di corretto interprete dei principi universali in materia di espiazione della pena. Signor Presidente, chiedendo che si torni al filo dei discorsi sereni e alla ragione. Non è il momento della propaganda sulla sofferenza, ma quello della necessità di condivisione, che suoni anche come segnale alla Nazione mediante il quale, superando gli interessi di parte, i consociati siano rassicurati sulla capacità del Parlamento di guardare con serietà ai diritti fondamentali dei cittadini, cosa che rappresenta certamente il fine vero,

causato dalla consapevolezza di dover trattare di un questione molto delicata, forse complessa, sicuramente contraddittoria, che pone in forte contrasto tra di loro alcuni tra i principi e gli interessi fondamentali che regolamentano la nostra società e le nostre stesse leggi. Da una parte, l'interesse alla sicurezza e alla tranquillità per tutti i cittadini, l'esigenza della certezza della pena; dall'altra, i principi del rispetto umano, della dignità umana, della considerazione e del tentativo di recupero sociali anche nei confronti di chi ha sbagliato, di chi ha violato le norme penali del nostro Stato. Possono sembrare interessi e principi in insanabile contrasto tra di loro, ma è la nostra coscienza, la nostra storia, la nostra cultura, le nostre leggi che ci dicono che questo contrasto non è insuperabile. L'articolo 27 della nostra Costituzione sta lì a dimostrarcelo, l'articolo 27 di una Costituzione tanto esaltata ma alle volte disattesa, che ci richiama ad un concetto civile ed umanitario della responsabilità penale e della pena, un significato profondo, non di afflizione, ma di recupero morale e civile del reo attraverso la privazione della libertà personale. Ci sono dei momenti in cui questo contrasto appare più acuto e questa è la situazione attuale delle nostre carceri, della popolazione carceraria italiana giunta a livelli di vera emergenza, con punte di vera drammaticità non solo per i detenuti ma anche per gli agenti stessi della polizia penitenziaria. Tutti lo sappiamo, è così, ed è colpa della politica che per tanti anni non è stata in grado di intervenire e di risolvere in modo adeguato ed efficiente la situazione. Ed ora, qui, cosa facciamo? Questo è l'interrogativo cui rispondere ricorrendo ai poteridel Parlamento e alle nostre leggi. Nessuno di noi si sogna nemmeno lontanamente di infrangere la legalità e principi ed esigenze di legalità perché vogliamo ricorrere ad un istituto giuridico previsto dalla nostra Carta costituzionale e dalle leggi ordinarie. Si tratta di un intervento urgente, emergenziale,

e tutto ciò viola pesantemente il dettato costituzionale di cui ho parlato poco fa. Non è un colpo di spugna perché si tratta di un provvedimento di indulto e non di amnistia. Riconosciamo con questo provvedimento la necessità di non cancellare i reati, di non cancellare i processi, di non cancellare le dichiarazioni di responsabilità e quindi di non cancellare i legittimi risarcimenti dei danni e i diritti delle persone offese da reato. Nei giorni scorsi, sono state fornite pubblicamente notizie sbagliate sul fatto che questo condono negherebbe la possibilità a centinaia e centinaia di operai colpiti da patologie tumorali letali, a causa dell'amianto, Non è vero: pena condonata non significa annullamento della responsabilità penale. Se c'è pena condonata, vuol dire che una pena è stata inflitta e che vi è stato un regolare processo. Non vengono cancellati con l'indulto né il processo, né le responsabilità penali, né le pene accessorie e neppure il risarcimento dei danni. A questo proposito, mi sia consentito intervenire su un altro punto interpretativo controverso, sollevato anche stamattina dal senatore Formisano,

È quindi inutile questo inserimento. Ne comprendo il significato pubblicitario e propagandistico, ma è inutile. Il programma politico che ha accompagnato le forze dell'Unione durante la campagna elettorale della scorsa primavera già prevedeva quest'intervento di clemenza - non lo possiamo dimenticare - ma lo coordinava con tutta una serie di altri interventi più specifici, proprio nell'ottica di una nuova politica della giustizia e della sicurezza: interventi strutturali ben noti a tutti, a cominciare da quelli nel settore edilizio, e interventi sulle norme, norme sostanziali penali, norme di rito penale, norme sull'ordinamento penitenziario, sulle misure alternative al carcere, sulla depenalizzazione, sulla legge Bossi-Fini, norme in materia di sostanze stupefacenti, norme a tutela delle persone offese da reato e abrogazione delle leggi vergogna della passata legislatura. Su alcune (poche peraltro) di queste materie, in Senato, come Gruppo dell'Ulivo, abbiamo già presentato e stiamo presentando alcuni disegni di legge: per l'abrogazione delle leggi Cirami e ex Cirielli, per una modifica della legge n. 689 del 1981, per una modifica dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, al fine d'inserire in Costituzione una specifica previsione di tutela e garanzia dei diritti delle persone offese da reato. Va, però, rilevato che, in materia di giustizia e sicurezza, sono ancora carenti l'intervento e l'iniziativa dell'Esecutivo. Questo è il vero problema che dovrà essere affrontato e risolto a breve. Ma nel frattempo che si fa? Come risolviamo la drammaticità di certe situazioni del carcere, dove ogni anno si verificano decine e decine di suicidi? L'intervento di indulto è reso urgente e necessario da concrete esigenze di umanità, di civiltà e anche di buonsenso, alle quali non ci possiamo - credo nessuno - sottrarre, anche se, sicuramente, esistono possibilità di interventi integrativi e migliorativi. Il fatto è che la norma costituzionale per l'approvazione dell'indulto impone una maggioranza particolarmente qualificata, a seguito della modifica costituzionale intervenuta nel 1992. Appare quindi necessario giungere ad un ampio consenso parlamentare. Questo è il motivo per cui vi sono state numerose discussioni sul numero e la qualità dei delitti da escludere dal beneficio dell'indulto. Non va sottovalutato il risultato finale: ieri sera, in Commissione giustizia, il sottosegretario Manconi e il Governo hanno ricordato come queste esclusioni dal beneficio riguardino qualche migliaio di detenuti,

Certo si poteva fare di più e si poteva fare meglio, come sempre. Ma questa non è una resa dello Stato, come ha sostenuto questa mattina il senatore Castelli; è, invece, un'assunzione di responsabilità da parte nostra e da parte dello Stato, per affrontare un problema delicato e scottante, che esiste, è sul tappeto e non può essere rinviato. Nessuno si può nascondere: è una decisione impopolare, difficile da far comprendere; forse per qualcuno è anche un rospo da ingoiare. Bisogna decidere: è un problema, sì, di coscienza, ma soprattutto politico e sociale, al quale va data una risposta politica e sociale. Per questo, pur conscio dell'esistenza di tante questioni e nodi ancora da affrontare e sciogliere, il mio voto non potrà che essere favorevole.*(Applausi

ha chiesto che venisse in Parlamento, in particolare al Senato, il Ministro dell'interno, per esprimere la propria valutazione sugli effetti, in termini di sicurezza pubblica, derivanti dall'applicazione delle norme che stiamo esaminando: finora non vi è stata nessuna risposta. Allora, se un cittadino qualsiasi intende affiggere un cartello di divieto di sosta davanti a casa sua deve chiedere il permesso a mezzo mondo e ne viene valutato anche l'impatto ambientale; 20.000 criminali - più sì, meno no - vengono messi in libertà non riusciamo a capire, da parte del titolare del Viminale o di un suo delegato, se ciò abbia o meno effetti sulla sicurezza di ciascuno di noi? Il Ministro dell'interno affermi in modo chiaro che non vi sarà nessuna lesione. Ma lo dica! Non ci può essere tale disinteresse nei confronti di ciò che il Parlamento sta esaminando in questo momento e che ha, comunque, quindi, una risposta: ovviamente, se sarà negativa, la valuteremo per la sua negatività; ma una risposta ci deve essere e, possibilmente, ci deve essere la presenza

e che, in qualche modo, è la cartina di tornasole di un dibattito che è stato vero, appassionato, convinto, con varie sottolineature ed approfondimenti significativi, che offrono la chiave di lettura di una sensazione che qualche collega ha voluto definire di disagio. Molti colleghi, infatti, hanno parlato di un profondo disagio nell'approcciarsi ad un provvedimento che, obiettivamente, non è ordinario. Proprio per questo, dobbiamo riscontrare che, accanto ai prevedibili strumentali atteggiamenti ostruzionistici di alcuni, che non sono riusciti - e mi scuseranno i colleghi del Gruppo dell'Italia dei Valori - ad offrire un grande contributo al dibattito in Aula,

nobile e alta partecipazione ai lavori dell'Assemblea. Posizioni pregne di considerazioni importanti, di perplessità molto spesso condivisibili, di proposte migliorative apprezzabili, di una convinta condivisione del provvedimento da parte di alcuni, pochi, o

e poi delle aree estreme che, in qualche modo, o lo sposano totalmente o lo contestano totalmente. Ciò rende ancora più improbo il compito di un relatore che non è relatore di maggioranza o di opposizione, visto che,

una serie di aggregazioni che servono a predeterminare una condivisione. Questo è un tema che è stato toccato nel momento in cui operava delle valutazioni complessive circa il percorso che si è materializzato. Voglio dire che il dettato previsto dall'articolo 79

c'è stata una modifica legislativa fondamentale, l'introduzione della depenalizzazione, delle misure alternative alla detenzione, un modello carcerario che tenga conto di quelle sofferenze effettive (penso alle ragazze madri e ai tossicodipendenti), quindi un modello complessivo che cambia. È chiaro che quello è il contesto generale all'interno del quale vi è la convinta condivisione di un provvedimento come questo che raggiunge naturalmente il *quorum* dei due terzi. possiamo ragionare di un momento emergenziale, come quello che stiamo vivendo dove il dato del sovraffollamento delle carceri è l'elemento eccezionale che ci costringe, per certi versi, a varare un provvedimento che, pur non avendo in un contesto complessivo tutte le condizioni previste, merita comunque un accoglimento perché la sofferenza - come è stato detto - non dovrebbe avere diritto di cittadinanza per alcuno e rispetto a tutti. Detto questo, signor Presidente, è evidente che un'altra serie di considerazioni bisognerà farle perché il disagio del quale molti colleghi hanno parlato, probabilmente, è legato al dato temporale e cioè al poco tempo avuto a disposizione per metabolizzare un provvedimento che, comunque, coinvolge valutazioni, princìpi ideali, scelte che incidono concretamente sulla sensibilità umana e politica di ognuno di noi e dall'altra parte ci ha costretto ad una serie di considerazioni tecnico‑giuridiche sia rispetto agli effetti immediati - a volte non sempre chiari per la difficoltà di trasferire in un dato numerico, in cifre, l'effetto concreto di un provvedimento come questo - sia rispetto agli effetti differiti che dovranno essere attentamente valutati. Accanto a questo, è certamente la consapevolezza di una fortissima aspettativa che si è legittimamente materializzata in un mondo che, proprio per la sofferenza che incarna, è comunque ad altissima sensibilità. Sono convinto, signor Presidente, che l'Aula saprà ancora una volta esercitare, come sempre, la sua altissima funzione recuperando quell'equilibrio e quel senso di responsabilità che sempre, di fronte a scelte difficili e delicate, ha saputo dimostrare. Ecco perché, Presidente, sono convinto che nel prosieguo dei nostri lavori riusciremo comunque a recuperare la giusta posizione che servirà a fare in modo che si possa concorrere

ritengo insopportabile - e sottolineo insopportabile - è una strana categoria dello spirito che ha animato questo dibattito, ritenendo che vi sia una ostentata superiorità morale in chi sarebbe contro l'indulto, a fronte di una dimessa, compromessa categoria dello spirito, che comprende coloro i quali invece, partendo dal disagio, sono iscritti d'ufficio e reclutati nell'idea della immoralità.

perché ritengo che sia compito del Ministro della giustizia rendersi conto della situazione. E siccome quel che c'è viene in evidenza, si ribalta in questa evidenza, con maggiore forza e maggiore propensione,

si alzò in piedi dicendo «pena di morte». Credo che se in quella circostanza avessimo fatto un *referendum* sull'introduzione della pena di morte, tutti, tranne pochi, ci saremmo consacrati all'idea della pena di morte. Un Governo (in questo caso il Governo e il Parlamento) guida i processi, non si lega demagogicamente alle circostanze che sono mutuabili in un dato momento. Perché? Perché evidentemente il metabolismo che c'è all'interno della società determina condizioni diverse e oggi nessuno trae vantaggio da questo punto di vista, né gli uni, né gli altri. Tant'è vero che non c'è un vantaggio, e arrivo a dire che c'è, da questo punto di vista, un disagio particolare, che nessun Gruppo politico è scevro da considerazioni differenziate, finanche Italia Dei Valori:

prova questa difficoltà e questa contaminazione con una idea che non è regolatrice, che appartiene un po' a tutti. Quindi, vi sono ragioni molto più forti che propendono perché, al di là di quelle che sono le proprie convinzioni, ci sia un vettore più giusto, che è quel punto di equilibrio di cui mi pare abbia parlato Brutti ieri e Casson in questa circostanza, un punto di equilibrio sul piano di quello che è dettato dalla norma costituzionale.

ma abbiamo il dovere di tenere conto di quello che c'è e di quello che si è verificato. Questo è un atto, come qualcuno ha detto, di deflazione umanitaria. Questa è la differenza con l'amnistia che, come ha scritto brillantemente il professor Onida, è uno strumento di deflazione giudiziaria: questo è un atto di deflazione umanitaria. Siamo in grado di compierlo? Sta alla responsabilità del Parlamento nella sua interezza. Questa è anche la ragione per la quale voglio dire ai colleghi della Lega non si può accampare l'idea di essere in contraddizione rispetto a quello che fa il Governo: è il Parlamento come tale, perché ci sono divisioni nella maggioranza e nell'opposizione, divisioni e disarticolazioni all'interno dei Gruppi parlamentari, quindi non c'è una omogeneità di vedute, una *Weltanschauung* comune da questo punto di vista. Ci sono frazioni che, come dire, esprimono una qualche perplessità e rispetto a questa perplessità bisogna dare una risposta. E allora, a fronte di una serie di inesattezze che ho colto in questi giorni sui giornali da parte di illustri commentatori della vita pubblica,

che ieri ha puntualmente risposto a tutte le parole in libertà su presunte illegalità, su questa paura che chi è per l'indulto è per l'illegalità. Non mi pare: non siamo in questo caso in presenza né di illegalità diffuse né di smarrimento di legalità né di inciuci o di colpi di spugna. Il professor Onida ieri ha detto opportunamente che, nel pieno e conseguente rispetto dell'articolo 27 della Costituzione, secondo la nostra legge, le pene inferiori a tre anni non dovrebbero normalmente e per principio essere scontate in carcere, ma in esecuzione di misure alternative come l'affidamento ai servizi sociali. Non a caso, dunque, l'indulto concede uno sconto di pena di tre anni: in questo modo, onorevoli colleghi, salva l'esclusione espressamente prevista alla generalità dei detenuti, saranno condonati quei tre anni che non dovrebbero essere scontati in carcere. Dopo il turno dell'indignazione morale, che ho visto crescere, di chi pensa che lo sconto di pena si possa dare ad un rapinatore all'impiegato di sportello che si prende qualche decina di euro per sveltire una pratica, debbo dire che da questo punto di vista si è cominciato a fare anche un elenco abbastanza strano di pericolosi criminali che dovrebbero usufruire dell'indulto, paventandosi improvvise scarcerazioni di pericolosi *serial killers*. E allora, con la pazienza necessaria, mi tocca dire, evidentemente dal mio punto di vista, che l'indulto è soltanto uno sconto di pena di tre anni, che chi ha commesso un efferato delitto contro la persona, generalmente punito nel nostro ordinamento con l'ergastolo, maturerà con tre anni di anticipo la facoltà di chiedere la liberazione condizionale. A quel punto un giudice, ammesso che l'interessato durante il tempo di esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da fare ritenere sicuro il suo ravvedimento, potrà concedergli eventualmente la liberazione condizionata. Quindi, per essere chiari, a meno che non si tratti di persone in galera da almeno vent'anni, che abbiano tenuto uno specchiato comportamento, che abbiano assolto alle obbligazioni civili di reato,

e alle ragioni espresse anche dal Governo su questo provvedimento, che per quanto mi riguarda ha la mia personale approvazione. Voglio ricordare ai colleghi dell'Unione e a coloro che hanno mostrato una qualche perplessità che il programma dell'Unione ci aveva affidato la responsabilità (qui parlo con partigianeria) di associare l'obiettivo primario di un nuovo codice penale all'approvazione di un provvedimento di clemenza.

di studiare un provvedimento diretto ad alleggerire l'attuale insostenibile situazione delle carceri. E lo dovremo studiare con la profondità e la drammaticità» - sottolineava quindi la drammaticità, come faccio anche io - «che l'attuale situazione carceraria ci impone. Già da anni» ‑ aggiungeva il presidente Prodi «anche dalle sedi più elevate, questo tema è proposto alla nostra attenzione. Oggi, all'inizio di una nuova legislatura, è nostro obbligo offrire un risposta». Il che non significa, lo dico al senatore D'Ambrosio, che più si è speso da questo punto di vista, che che partendo da questo elemento si debba contraddire l'idea di riforme strutturali, che spero trovino l'ampiezza, la complementarità dell'apporto e la cospirazione tra Governo e Parlamento; significa quindi venire incontro, come ha detto il presidente Prodi, e il Governo, in realtà, ha soltanto sollecitato il Parlamento. Esso ne ha seguito le autonome e libere determinazioni e lo fa anche accettando quel che sarà il risultato. tanto più autonome e tanto più libere in quanto, come ha scritto ancora una volta il presidente Onida, l'accordo tra maggioranza e opposizione in questo caso non è frutto di una grande intesa su un nuovo Governo, né di grande inciucio, ma conseguenza diretta della norma costituzionale che richiede per l'approvazione delle leggi di amnistia e di indulto una maggioranza di due terzi. Queste sono le ragioni, onorevoli colleghi, per le quali personalmente sono a favore

Casson voglio dire che per gli incidenti sul lavoro il risarcimento del danno resta immutato, per cui non c'è ragione di avere perplessità, come ho visto anche da alcune manifestazioni di parte sindacale, in cui si è tentato, con giusta determinazione, di far riferimento a quello che era eventualmente il motivo di indulto che poteva declinare in altra direzione. Con questo ringrazio tutti i colleghi, soprattutto per la capacità che hanno avuto di ascoltare e per le parole, che a tratti ho seguito in maniera convergente,

Signor Presidente, proporrei, con il consenso degli altri presentatori, che gli ordini del giorno G115 e G116 fossero unificati. Molti dei firmatari hanno sottoscritto l'uno e l'altro, i contenuti sono convergenti, è pertanto utile che vengano unificati.

dei procedimenti, relativi al risarcimento del danno per causa di lavoro, proposti da lavoratori che hanno subito lesioni colpose gravi o gravissime. Il problema, per il quale il relatore ha parlato di un accoglimento come raccomandazione, è l'impegno del Governo «ad emanare provvedimenti normativi».

precisa orientata all'edilizia penitenziaria. Se vi è un'assunzione d'impegno di questo tipo, con questa precisione, e non un'intenzione generica, va bene, nel caso contrario chiedo sia sottoposto a voto.

Presidente, è evidente che se parliamo dell'ordine del giorno G103, l'impegno, che il senatore Mantovano propone al Governo di assumere come

così come lo stanziamento nella legge finanziaria; può essere un invito al Governo a tenerne conto e siamo sicuri che il Governo lo farà, ma non è un obbligo rispetto al quale si può materializza un impegno preciso. Ecco perché, signor

Se uno finalizza in maniera partigiana, io credo che ogni Ministro, e quindi anche il mio Ministero, abbia l'idea di potenziare, come è giusto fare, assieme ad altre misure da porre in essere, misure strutturali.

Apprezzo la prudenza del relatore e anche l'adesione, non voglio dire pedissequa, ma ulteriormente motivata, del Governo.

e non congiunturali, alle quali dobbiamo dare una risposta, e la daremo al momento giusto. Dire adesso che il Governo non può essere impegnato, come afferma il relatore, perché questo impegno graverebbe in termini potestativi, limitando quelli del Governo, è una

il senatore Castelli e non il Ministro della giustizia. Quindi, l'Aula sovrana impegna il Governo. Questo voto diventa allora importante perché è la prima occasione con la quale si può dar seguito concretamente alle tante parole che sono risuonate in quest'Aula

lo strumento indicato è stato attivato nella scorsa legislatura e consente due questioni. Certo, non ha funzionato molto bene nella scorsa legislatura perché non siamo riusciti ad alienare

di riattivazione di quei reparti che oggi sono chiusi, e di ristrutturazione dei vecchi penitenziari, senza pesare sul bilancio dello Stato e in tempi enormemente più brevi di quanto non accada oggi per fare nuovi penitenziari. dal ministro Mastella una parola definitiva su questa questione perché se dice che è contrario a questo ordine del giorno significa che non intende più avvalersi di questo strumento e credo che sia importante sapere l'orientamento del Governo in materia. PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo

Nella specie, si tratta di un'iniziativa che riguarda una società che è già stata realizzata; si cerca di utilizzare le risorse derivanti dalla vendita delle strutture carcerarie dismesse per costruirne altre. Si tratta altre. Si tratta di una scelta così specifica anche rispetto alla parte che è già stata realizzata e ai programmi obiettivamente già accolti, che il relatore non si sente di vincolare il Governo in tal senso, fermo restando che se il Ministro

e anche qualche modesta riflessione che avevo fatto personalmente, mi portano ad evitare di confondere la causa con l'effetto. L'effetto sul quale dobbiamo ora agire è l'inumana

lo accoglie, dice di voler cancellare questo strumento e che non intende avvalersene. Le due società oggi sono vive e operanti. Volevo sapere dal Ministro se intende lasciarle vive o se le ritiene una via da non praticare: questo è il punto fondamentale.

Credo che gli altri tasti siano la riforma del codice penale, già oggetto della commissione Grosso e poi della commissione Nordio nel Governo di centro-destra, esistono le misure alternative. Operiamo una discussione seria a partire da settembre. Per quanto riguarda invece l'ordine

una certa struttura che è stata predisposta dal precedente Governo, quindi legandosi le mani rispetto, perfino, alla possibilità di scelta del tipo di intervento. Non è come dice il presidente Biondi. In quest'ordine del giorno si dice al Governo: devi costruire nuove carceri attraverso quella struttura. Ma se togliamo al Governo anche la possibilità di decidere sulle strutture attuative, veramente siamo in una Repubblica dove il rapporto fra Governo e Parlamento viene completamente stravolto. Per questi motivi. noi voteremo convintamente no all'ordine del giorno

Signor Presidente, ho letto - spero con la dovuta e necessaria attenzione - l'ordine del giorno in esame: se non vi fosse un giudizio di valore così recisamente negativo sul provvedimento di cui stiamo discutendo, le considerazioni qui poste in positivo potrebbero trovarci d'accordo. È un po' difficile convergere su ordini del giorno che, in premessa, si schierano duramente contro la posizione che abbiamo assunto sul provvedimento. Se, invece, vi fosse una rinunzia alla premessa e il senatore Mantovano puntasse sul dispositivo, potremmo convergere.

chiedo che sia sottoposto al voto perché contiene un impegno di inserimento nella legge finanziaria di un'adeguata copertura per la legge sulle vittime del dovere.

vorrei ricordare che peraltro anche nel programma dell'Unione esiste un esplicito impegno della nostra maggioranza perché sia ampliata nel nostro ordinamento la platea delle vittime dei reati,

Presidente, su quest'ordine del giorno vorrei fare un'osservazione.

in linea generale e di principio, l'opportunità della revisione della normativa penale, il trovare pene alternative e così via,

si riferisce ad alcune leggi in particolare oggi vigenti, quali la normativa sull'immigrazione, il sistema sanzionatorio in materia di tossicodipendenza, all'abrogazione di norme introdotte nella legislatura precedente che riguardano mancati benefici della legge Gozzini. Capisco che questo è stato un tema di grande dibattito nella scorsa legislatura, ma mi pare impossibile prevedere in un ordine del giorno impegni di tale portata che, per giunta, chiedono espressamente di riformare, rivedere, bocciare leggi

facoltà. D'ONOFRIO *(UDC)*. Signor Presidente, mi permetto di chiedere ai sottoscrittori di quest'ordine del giorno, a cominciare dalla collega Finocchiaro, se hanno seriamente riflettuto su un fatto. Noi con l'ordine del giorno, in quanto Parlamento, possiamo vincolare il Governo a fare cose che il Governo può fare in quanto Governo. Non possiamo scrivere un ordine del giorno con il quale chiediamo di fare leggi,

"a dare compiuta attuazione al regolamento penitenziario, oggi calpestato". Oggi calpestato da chi? Dalla Polizia penitenziaria? Se si afferma una cosa del genere e il Ministro accoglie una proposizione del genere

si impegna il Governo a incaricare le prefetture di fare un monitoraggio sugli effetti dell'indulto anche in termini di sicurezza. Insomma, chiedo al Governo che si metta d'accordo con se stesso. Il Ministro dell'interno continua a non venire

non soltanto corrispondono a tre punti precisi del programma dell'Unione su questi temi... *(Commenti dal Gruppo AN).* Scusate, la Costituzione dice che il Governo ha l'iniziativa legislativa, come ogni singolo parlamentare, colleghi. Può presentare disegni di legge e tanto più è giustificato a farlo nel momento in cui lo invitiamo a presentare disegni di legge su punti precisi del programma di governo dell'Unione. Non mi pare assolutamente niente di strano, né di incostituzionale, né tanto meno questo toglie ai singoli parlamentari la possibilità di presentare provvedimenti sul tema.

è un punto non esplicitato, capisco bene: calpestato da chi, come, perché? Sarebbe complicato ragionare e può essere equivoco e quindi mi sento di accedere alla richiesta di eliminare le parole «oggi calpestato».

provvedimento e credo che lo approvò addirittura in prima lettura in Aula e non mi sento di eliminare questo riferimento, perché anch'esso è un punto del nostro programma di Governo.

gli ordini del giorno sono molto rilevanti e a volte tendiamo a trascurarli un po' in Aula. Invece vedo che, soprattutto in questa seconda parte della discussione, si dà ad essi l'importanza che meritano, perché

perché riguardano punti molto rilevanti della politica della giustizia. Ritengo che, se su alcuni di questi punti si può verificare in quest'Aula una convergenza più ampia rispetto a quella della maggioranza, sarà certamente un fatto positivo per il nostro lavoro.

il fatto che sia interesse comune avere un controllo, un monitoraggio, una verifica, visto che su questo sono state espresse opinioni diverse, in modo che in tempi molto rapidi si possa si possa conoscere e valutare se e quali effetti questo provvedimento abbia determinato. Mi auguro che sul maggior numero possibile di questi punti, posti ai

un ordine del giorno attraverso il quale il Parlamento afferma un principio grave e rilevante, quello cioè del mancato rispetto del regolamento penitenziario. Ho ascoltato con attenzione l'intervento della collega Finocchiaro quando ha ricordato che il Governo ha anche funzioni legislative, ma vorrei ricordare alla collega che il dibattito politico di questi giorni si è incentrato sulla funzione parlamentare o meno a seguito dell'eccessivo ricorso al voto di fiducia da parte del Governo e mi sembrerebbe paradossale, nel momento in cui il dibattito politico del Paese è concentrato su questo aspetto, che il Parlamento delegasse al Governo ulteriori funzioni di decretazione di urgenza. Mi troverei un attimo in imbarazzo. inoltre, la finezza del collega Salvi quando lessicalmente suggerisce una modifica del testo così com'è, quindi là dove si inviterebbe il Governo ad attivare eventuali iniziative legislative: non non è in capo al Governo la funzione legislativa piena, il Governo non legifera, il Governo può attivare iniziative legislative e quindi la decretazione d'urgenza. Ma su entrambe le riflessioni manifesto parere fortemente contrario relativamente all'approvazione dei tre capoversi, sia per una valutazione politica di fondo sia perché non è scritto nel programma della Casa delle Libertà. Ho ascoltato con interesse gli interventi dei colleghi della maggioranza che parlano di programma dell'Unione: qui siamo in un'Aula parlamentare, siamo nel Parlamento, e credo che le scelte dei singoli parlamentari si debbano attenere, su questi temi, anche alle loro singole valutazioni. Non stiamo svolgendo un'assemblea politica, stiamo legiferando; ritengo che, là dove si parla di attivare iniziative legislative e si danno valutazioni di merito in quanto si afferma che il carcere viene previsto come sanzione per la violazione di una norma in materia di espulsione

Mi trovo a disagio, perché si tratta di una serie di temi molto differenti gli uni dagli altri. Alcuni possono essere innocui: ad esempio «promuovere l'istituzione di un Garante nazionale per l'esercizio e la tutela dei diritti dei detenuti»; da quando abbiamo il Garante per la *privacy* sappiamo che la nostra *privacy* è molto più tutelata prescindo dal titolare di questa istituzione. Invece ho un dissenso specifico quando si dice di «riformare il sistema sanzionatorio in materia di tossicodipendenze, oggi particolarmente pesante, che non discrimina tra sostanze diverse e che prevede sanzioni carcerarie elevate anche per la semplice detenzione di droghe leggere»; significa allora

Vorrei solo replicare all'osservazione del collega Mantovano in ordine alla contraddittorietà dell'avere inserito in una parte dell'ordine giorno il richiamo all'attenzione da parte del Governo su quella che è la vigilanza sul territorio e il coordinamento con gli enti locali. Io non trovo affatto contraddittorio, quando il Parlamento assume un provvedimento che ha carattere legislativo, che si impegni il Governo nella sua interezza, e quindi anche il Ministero dell'interno, a fare quanto sia possibile perché tale intervento abbia il minore impatto in termini sociali sul territorio stesso. Trovo contraddittorio

il Senato impegna il Governo, in sede di attuazione del provvedimento di indulto, - ad impartire tempestivamente le opportune direttive alle prefetture, al fine di garantire il mantenimento della sicurezza sul territorio

Signor Presidente, senza voler trovare a tutti i costi una soluzione compromissoria, devo dire al senatore D'Onofrio che il Parlamento non è che possa imporre qualcosa al Governo e viceversa; quindi, c'è rispettiva autonomia dal punto di vista costituzionale. Però mi sembra che le indicazioni che venivano dalla

ovvio che questo è un fatto di legge, non un atto di natura amministrativa, quindi sarà sempre il Parlamento come tale che dovrà giudicare sul disegno di legge che proporrà il Governo.

Presidente

la normativa sull'immigrazione, specie laddove il carcere viene previsto come sanzione per la violazione delle norme in materia di espulsione, e di riformare il sistema sanzionatorio in materia di tossicodipendenze - e lì si dà un indirizzo oggi particolarmente pesante, che non discrimina tra sostanze diverse che prevede sanzioni carcerarie elevate anche per la semplice detenzione di droghe leggere, mi chiedo - e chiedo al Governo se ci si trovi dinanzi ad un'inversione dei ruoli. Evidentemente ci troviamo in un momento paradossale, in cui sembrerebbe che sia la maggioranza parlamentare a dare un programma al Ministro della giustizia.

Vorrei poi dire al senatore Schifani, che fa parte di una Commissione che certamente sarà di maggiore rilievo, che se si fosse fatto riferire o avesse avuto la bontà di scorrere alcuni piccoli fotogrammi

non ho capito il criterio per cui si vota per parti separate. In ogni caso,

bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo su tutti gli emendamenti, ad eccezione che sugli emendamenti 1.0.3, 1.0.300, 1.0.301, 1.0.302 e

Signor Presidente, dopo questa illustrazione molto partecipata, il relatore vuole ancora una volta premettere che, rispetto a provvedimenti come questi, non esistono relatori di maggioranza o di opposizione rispetto alle composizioni canoniche. canoniche. Il relatore cercherà di orientarsi nell'indicazione dei pareri sulla base del dibattito che si è svolto ieri in Commissione e del dibattito che si è svolto fin qui in Aula. Capisco che qualcuno possa provare fastidio, ma io non considero mai un adempimento lo svolgimento di una funzione delicata e importante come quella parlamentare; quindi, chi non vuole ascoltare può tranquillamente allontanarsi. Il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti, tranne su tre tipologie di emendamenti, per i quali si rimette all'Assemblea

al limite temporale di applicazione dell'indulto. Molti colleghi hanno riconosciuto, ripetendo un'affermazione che il relatore aveva fatto ieri in Commissione e stamattina in Aula, che normalmente i provvedimenti d'indulto vengono concessi per La seconda tipologia di emendamenti è relativa all'abbattimento della pena pecuniaria; il relatore ed altri colleghi hanno evidenziato come sia anomalo, nel momento in cui si interviene con un provvedimento come questo, per deflazionare le carceri,

In questo caso, signor Presidente, non c'è nessun emendamento che sopprima l'indulto per quanto riguarda le pene pecuniarie; per questo motivo, il relatore sottoporrà all'Assemblea la valutazione

dall'applicazione dell'indulto; il relatore, come altri colleghi intervenuti in Assemblea, riscontra l'anomalia dell'esclusione dell'articolo fra le figure alle quali applicare o meno l'indulto. Abbiamo già svolto questo ragionamento in maniera concreta, ricordando all'Assemblea come la previsione sottoposta al nostro esame per l'approvazione escluda già

Il problema, signor Presidente, è quello di ricomprendervi una categoria di reati nei quali sicuramente merita di essere incluso l'articolo 416-*ter* (che è il voto di scambio mafioso come rubrica semplificata,

abbiamo detto che viene utilizzato come parametro l'abbattimento da 10.000 a 1.000 perché non è prevista la soppressione, mi rimetto all'Assemblea 1.630, 1.631, 1.632 e 1.633,

1.257, 1.4003, 1.259, 1.2590,

(salto i passaggi, ma chi è esperto in materia può capire), costruiamo per i prossimi sette anni e mezzo sostanzialmente l'impunità. Questo è quanto stiamo facendo, colleghi:

consentirebbe di liberare più di 11.000 detenuti e quindi si raggiungerà esattamente lo scopo che, almeno a parole, ufficialmente, viene dichiarato in quest'Aula, che è quello di deflazionare le carceri. Non si capisce perché si debba stabilire una

il provvedimento può comunque diventare legge. Veramente, invito l'Aula a meditare su quello che stiamo facendo. Si vuole fare l'indulto, benissimo, lo si faccia, prendiamo atto che questa è la volontà del Parlamento,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono fermamente contrario a questo indulto così esteso. Sono contrario perché non riesco francamente ad afferrarne le ragioni politiche. Sarà forse perché sono entrato in politica da pochi mesi avendo esercitato per tutta la vita un'altra professione.

oltre a essere controproducente sul piano dell'educazione alla legalità, è sempre una scappatoia per evitare di risolvere o quantomeno di differire *sine die* la soluzione dei veri problemi della giustizia e dei veri problemi delle carceri. Dal 1949 al 1990 sono stati emessi ben 11 provvedimenti di amnistia e di condono, con la media di uno ogni quattro anni, sempre

Non credo che ci sia Paese civile al mondo in cui il processo penale abbia una durata media di otto anni, quant'è quella del nostro processo penale. Non credo neppure che ci sia un Paese in cui, per risolvere dei fenomeni si agisce sugli effetti e non sulle cause, come si è fatto in Italia con la cosiddetta che ha stabilito il risarcimento dei danni, mentre nessun Governo - tantomeno l'ultimo - si è mai preoccupato di prendere provvedimenti per abbreviare i tempi dei processi.

Cito solamente, in particolare, che solo il 20 per cento dei detenuti usufruisce dell' acqua calda ogni giorno. Solo il 10 per cento dei detenuti ha un lavoro:

industriale intorno alle carceri. La stessa cosa è avvenuta in Francia, che pure aveva i nostri problemi carcerari, perlomeno dal punto di vista delle strutture; non si è potuto naturalmente creare il lavoro in carcere, ma si sono creati degli istituti che consentono ai detenuti di andare a lavorare fuori dal carcere, sotto la vigilanza della polizia penitenziaria. In Italia di tutto questo non si trova traccia. Credo che la maggioranza che ha approvato alla Camera dei deputati questo provvedimento non si sia resa effettivamente conto di quale sia la portata di un indulto di queste dimensioni: è stato detto che usciranno 12.000 detenuti condannati con sentenza definitiva. Bene:

che è stato condannato a più di tre anni, che ha una pena residua di tre anni, ha commesso un reato grave. Ho consultato i colleghi di Milano e mi hanno detto che solo per rapina a mano armata usciranno 358 condannati: per rapina commessa con armi proprie. Questa è una cosa gravissima. Ma la cosa più grave...

la cosa più grave è che verranno messe nel nulla circa 100.000 sentenze di condanna, qualcuno non lo sa, ci sono ben 67.000 sentenze a condanne inferiori a tre o quattro anni, se si tratta di tossicodipendenti, che hanno il decreto di sospensione e che sono in attesa del giudizio del tribunale di sorveglianza per vedere se il condannato deve essere affidato al servizio sociale. Ma oltre a questi, ci sono quelli già affidati al servizio sociale (circa 40.000), che per ora sono sottoposti all'assistenza dei servizi sociali e alla sorveglianza della polizia, se occorre, ma che rimarranno liberi di fare quello che vogliono.

a tutti coloro che sono sotto processo. Mi metto nei panni dei miei ex colleghi che devono istruire dei procedimenti e mandarli avanti sapendo che ci sarà una condanna vana. E se dovesse esserci una condanna superiore ai tre anni, ci sarà il ricorso al rito abbreviato, con l'abbattimento di un ulteriore terzo, e se non basta, ci sarà il patteggiamento in appello. appello. Credo che non ci sia resi conto perfettamente delle dimensioni enormi di questo provvedimento, che non aiuta i poveri disgraziati. Questo è un mito. Anche questo è un mito! Non li aiuta affatto.

che sa benissimo, meglio di me, che anche l'economia è condizionata fortemente dalla criminalità, da quella che viene definita piccola criminalità, ma che non lo è. Sono delle scelte precise che si fanno. Io però, signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sono reso reso perfettamente conto di una cosa, ossia che se si dovesse respingere in questo momento *tout court* questo provvedimento, effettivamente deluderemmo delle forti aspettative che si sono create

proprio lo scopo che ci è stato detto dal relatore essere la *ratio* di questo provvedimento, cioè quello di sfollare le carceri. secondo quello che è stato riferito dallo stesso rappresentante del Ministero, i detenuti che uscirebbero per un provvedimento di indulto di un anno sono 11.346 con pene residue inferiori

di quel che è un illecito amministrativo e che, solo perché reiterato, viene considerato reato e punito con la reclusione da uno a quattro anni fa. Mi riferisco agli extracomunitari, che espulsi dall'Italia, rientrano. Secondo le indicazioni fornite dal Ministro della giustizia, solo nel 2005 sono passati per le carceri 11.500 extracomunitari puniti solo per non avere fatto niente, per essere soggetti che lavorano in nero e che vengono sfruttati da datori di lavoro senza scrupoli. Sono questi i provvedimenti strutturali che bisognava prendere! Oggi ho firmato un altro provvedimento per allargare le misure alternative al carcere. Questi sono i provvedimenti strutturali che servono ad impedire il sovraffollamento delle carceri!

derivante - come è stato ricordato - da un'approvazione in una misura così estesa, cioè quella dei tre anni di reclusione. Come è stato ricordato in termini percentuali, alla data del 22 giugno 2006 per sanzioni penali detentive fino ad un anno di reclusione risultano ristretti 11.346 detenuti. Il Ministro della giustizia ci riferirà la cifra al netto delle esclusioni che il provvedimento di indulto pone, ma immagino non si discosti molto da questa cifra. Quindi, se l'emendamento e se l'obiettivo del provvedimento fosse quello di alleggerire la popolazione carceraria, il risultato già si otterrebbe. Non riesco a comprendere le ragioni di ostilità

a rendere più dignitoso il provvedimento, dando per scontato che ormai la volontà dell'Assemblea è quella di approvarlo. Vorrei ricordare ai colleghi che magari non si sono occupati direttamente di questo provvedimento che lo stesso si applica anche ai recidivi, anche ai recidivi, ovvero quegli individui che hanno scelto di vivere dedicandosi alla delinquenza, che non sanno fare altro, che ogni volta che sono fuori dai penitenziari si dedicano a delinquere. È certo che costoro, non appena verranno messi in libertà, si dedicheranno all'unica attività che conoscono: quella di vessare i cittadini onesti. Questo è il dato fondamentale. D'altra parte - e qui mi rivolgo ai colleghi della passata maggioranza - quando abbiamo votato la cosiddetta ex Cirielli, che andava esattamente esattamente in questa direzione, si era detto che lo Stato deve essere clemente con chi sbaglia una volta e inflessibile con i recidivi e con chi dedica la vita a delinquere. bocciando questo emendamento, fate esattamente il contrario, votate in senso contrario a quello che avete votato nella scorsa legislatura. Francamente consentitemi di non capirne anche perché credo che su un provvedimento di questa natura non vi possano essere ordini di scuderia, non vi possa essere un ordine di partito, una fedeltà o una linea politica. È chiaro che stiamo votando su questioni di natura etica, in cui ognuno è libero di scegliere come

Oggi stiamo per approvare un indulto così ampio che tirerà fuori dagli istituti di pena migliaia e migliaia di criminali. Un anno fa si valorizzava in negativo la recidiva, non mettendo sullo stesso piano il delinquente occasionale e quello professionista; oggi, se si bocciasse questo emendamento questa parificazione sarebbe assoluta

CASTELLI *(LNP)*. Non più tardi di qualche ora fa ci siamo riempiti la bocca di preoccupazioni per le vittime. È stato presentato, e qualcuno ha approvato (non noi, perché lo ritenevamo ipocrita), un ordine del giorno in cui ci si preoccupava delle vittime. Nel testo che stiamo esaminando la parola «vittime» non esiste, non la troverete mai, non c'è; ci sono soltanto i reati, i colpevoli, ci si occupa soltanto di Caino,

Questo emendamento si preoccupa delle vittime e pone un principio, credo assolutamente civile: che possa essere liberato soltanto chi ha ottenuto il consenso delle vittime o dei loro parenti. Su questo emendamento chiediamo

non è vero che soltanto il 10 per cento dei detenuti lavora; la cifra è nettamente superiore: il 10 per cento si riferisce a lavori con società esterne, ai quali bisogna aggiungere tutti i detenuti che lavorano invece per attività interne al carcere.

Sappiate che in Italia vi sono detenuti che fanno causa ai loro datori di lavoro; sappiate che in Italia i detenuti lavorano con una mercede che, grazie alla legge

attività deflattiva posta in essere, ed ancora vigente, è all'interno della Bossi‑Fini. Ricordo altresì che l'articolo 15 prevede che i detenuti stranieri che abbiano meno di tre anni da scontare, possono tornare liberi a una sola condizione: che non tornino più a vessare i cittadini italiani sul loro territorio. Mi sembra un'azione di grande civiltà. Finora ne abbiamo liberati oltre 5.000;

Si afferma che l'indulto non cancella il processo civile e che, quindi, le vittime saranno risarcite. Ma scusate, voi pensate veramente che chi delinque, sia a basso livello che ad alto livello, si preoccupi di risultare nullatenente nullatenente o di non essere capiente per poter risarcire le vittime? La verità è che si liberano tutti, anche se la vittima non è stata risarcita, con la certezza che non sarà risarcita. Ancora una volta

però mi corre l'obbligo di stigmatizzare quello che ha fatto un Gruppo, semplicemente per questioni mediatiche e per poter dire che ha presentato 1.500 emendamenti.

dei reati per la verità più odiosi, perché commessi contro la pubblica amministrazione e da pubblici ufficiali.

a chi dichiara che comunque le vittime verranno risarcite, che il reato non viene cancellato, che si è pensato anche al danno che è stato fatto. La bocciatura ovviamente prevedibile di questo emendamento dimostrerà senza alcun dubbio che non interessa nulla di tutto ciò. In questo caso si parla dei corruttori, ma evidentemente la *ratio* è la stessa anche per i concussi o per i corrotti: noi liberiamo tutti, anzi voi liberate tutti. Non importa se il danno è stato in parte o in tutto riparato, non importa se le vittime sono state ristorate, non importa se il danno alla pubblica amministrazione in qualche modo è pervenuto a minori effetti, basta liberare. C'è questa *cupio* *liberandi* (lasciatemela

e per il futuro: come abbiamo prima dimostrato, le porte del penitenziario non si chiuderanno più per molti anni. Non so se avete ricevuto anche voi, colleghi, le

legati alla violazione dei marchi, verranno completamente sanati con questo provvedimento. Pensate quale immagine stiamo dando all'estero e come gli investitori stranieri potranno venire nel nostro Paese ad investire. Ricordo che

Unite. Noi andiamo a sottoscrivere patti contro la corruzione e poi diciamo al mondo intero: «Abbiamo scherzato, liberiamo tutti». Abbiamo ancora poche occasioni per avere un sussulto di dignità in quest'Aula, ma ormai l'ora è tarda, il dibattito non c'è, le decisioni sono state prese, il Senato ratifica supinamente le decisioni della Camera.

Presidente, una piccola rivincita: quando abbiamo fatto la riforma del diritto societario cui - ricordo - tutta Europa plaude, la maggioranza, incluso il senatore D'Ambrosio che dice di non aver fatto mai politica - su questo mi consenta di dissentire -, l'ha trasformata nel cosiddetto «falso in bilancio», che è una falsità perché tutti quanti possono vedere che il falso in bilancio è rimasto un reato. Per anni ci hanno letteralmente perseguitato dal punto di vista mediatico, dicendo che avevamo cancellato i reati societari

o invece andiamo avanti su una linea di rigore. Noi vogliamo e crediamo che dall'indulto vengano esclusi coloro i quali si sono macchiati di reati societari. Adesso vorrei capire cosa farà la maggioranza. Chi saranno coloro i quali diventeranno amici dei furbetti? *(Applausi dal Gruppo* *AN).* Vedete, c'è una questione che a me ha lasciato perplesso. C'è un dubbio che mi arrovella da un po' di tempo: come mai l'indulto e l'amnistia non sono mai passati nella scorsa legislatura e oggi invece passano così rapidamente, così a tamburo battente anche in quest'Aula? Cos'è cambiato

un altro motivo per il quale l'indulto passa così rapidamente perché, come abbiamo più volte denunciato, l'indulto non si applica a chi sta in carcere, quindi non è vero che si applica per deflazionare le carceri. Si applica molto di più e in maggior misura a chi in carcere rischia di andarci e, visto che siamo in tema di assicurazioni, si sono garantiti l'assicurazione contro il carcere, perché con questo provvedimento in carcere non ci vanno più e non parleranno più. Questo è il punto fondamentale.

Stiamo parlando dei reati di rapina aggravata e di estorsione aggravata, per le quali questo emendamento propone l'esclusione oggettiva dall' indulto. Sono proprio i reati che sono soggetti al maggior tasso di recidività.

La votazione dell'articolo 1 è accantonata per consentire all'Assemblea di pronunciarsi sugli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Presidente, ho rinunciato personalmente alla presentazione degli emendamenti di cui al testo appena votato, ma vorrei avere la facoltà di sottoporre ai colleghi dell'Assemblea i vari È infatti vero che noi oggi ci pronunciamo rispetto ad un indulto che dà la possibilità a decine di migliaia di persone di uscire dalle carceri, ma è anche vero che è importante che questa Assemblea si preoccupi di individuare la possibilità

propongono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, di un fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei detenuti che beneficeranno dell'indulto

Presidente, mi permetta di congratularmi con lei e di ringraziarla per la conduzione della seduta, che è stata veramente di grandissima professionalità. *(**Generali applausi).* PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Zanda. In finanziaria, quando ero espressione della maggioranza, facevo anche di meglio! Temo, quindi, che non si ripeterà!

all'indulto che oggi ci riunisce è quanto mai attuale e riguarda il provvedimento generale di clemenza richiamato dall'articolo 174 del codice penale ed ispirato a ragioni di opportunità politica e sociale che rendono quanto mai necessaria l'approvazione

Intendiamo dare una risposta al problema annoso ed insostenibile del sovraffollamento delle carceri atteso ormai da ben 15 anni, sollecitato da più parti. Mi riferisco, in particolare, all'appello - che è stato più volte richiamato da altri colleghi Santo Padre, Giovanni Paolo II, rivolto alle Camere il 14 novembre 2002, nel quale egli evidenziava come, senza compromettere la necessaria tutela della sicurezza, meriti attenzione la situazione delle carceri. La situazione insostenibile e di crescente invivibilità delle carceri giustifica l'intervento senza indugio, al fine di ripristinare la legalità nei nostri penitenziari e l'efficienza nel campo della giustizia penale. Basti pensare che nelle case circondariali sono ammassati in condizioni aberranti circa 20.000 detenuti in più rispetto ai posti disponibili. Si tratta di condizioni inconciliabili con lo spirito della nostra Carta costituzionale

di umanità». È, inoltre, regola indiscussa del buon vivere civile, peraltro spesso disattesa, che nella sanzione si dovrebbe offrire al reo un percorso espiativo indirizzato verso il pieno recupero ed il reinserimento nella società. Purtroppo, in Italia, allo stato attuale il sovraffollamento costituisce una pena aggiuntiva a quella comminata dal giudice e finisce per rendere quasi inesistente la possibilità di percorsi individuali di riabilitazione sociale. Il paradosso è alla luce del giorno: proprio laddove si lavora per il recupero, si annidano le cause di un non recupero e di recidiva. Perciò, l'indulto vuole essere, e si impone, quale vera e propria urgenza sociale. Nessuno di noi considera l'indulto panacea dei mali delle prigioni e non vi è dubbio alcuno che si deve procedere nel senso di una complessa riforma. Voglio sottolineare, però, in maniera decisa che su un piano stanno le opinioni politiche, su un altro, ben distinto, la morale. Non possiamo in alcun modo accettare che taluni, nascondendosi dietro falsi proclami demagogici, dipingano come immorali coloro che si sono fatti promotori di una misura di clemenza e si sono spesi in una celere adozione del provvedimento. Ovviamente sarebbe riduttivo ed errato intenderlo esclusivamente come un mero sconto di pena in favore dei soggetti condannati per ripagarli delle assurde condizioni carcerarie; né si può confondere un indice di voluto adeguamento ai tempi con l'ipocrita e sterile critica che vorrebbe imputare al Governo la difesa dell'illecito. Non dimentichiamo che dalla legge in esame sono esclusi quei reati che destano nella collettività un particolare allarme sociale, proprio come chiedeva il Santo Padre. Gli stessi soggetti, in maniera strumentale e menzognera, si premurano si premurano di celare all'opinione pubblica che nessuna eccezione sarà riconosciuta per i terroristi italiani e internazionali, per i mafiosi, per i nuovi schiavisti, per per gli sfruttatori della prostituzione, per gli stupratori, per i pedofili, per i rapitori, per i razzisti e per i commercianti di stupefacenti. Così come non sono a rischio i processi, né i diritti dei risparmiatori truffati, neanche gli esiti delle azioni civili incardinate aventi ad oggetto i reati indultati. Nel contempo, corre l'obbligo di sottolineare che mediante la concessione dell'indulto si salvaguardano anche i diritti di chi opera quotidianamente nelle strutture penitenziarie, riferendomi al personale amministrativo e di polizia penitenziaria, nonché a quanti si occupano del recupero sociale dei detenuti a cui va garantito un luogo di lavoro quantomeno sicuro, laddove la condizione attuale determina una vera e propria umiliazione per queste categorie. Pertanto, il provvedimento di clemenza, per il quale ci schieriamo positivamente, dev'essere inteso quale mezzo per il ripristino della legalità e del buon governo dell'amministrazione della giustizia.

di un partito di questa maggioranza di coalizione; un partito di parte. Non bisogna ergersi a censore e condannare gli altri. Questo è il messaggio che volevo dare, con rispetto, agli amici che invece stanno creando molta confusione nell'opinione pubblica. Rispetto dignitosamente il pensiero dell'opposizione che democraticamente e onestamente, secondo la sua *forma* *mentis*, ha dato

mi corre l'obbligo di precisare subito che questo non era un provvedimento di maggioranza; lo ha ribadito il Presidente del Consiglio così come il ministro della giustizia: si tratta di un provvedimento parlamentare. è stato giusto e sarà sempre giusto che quando i provvedimenti sono di natura parlamentare, vi sia il più ampio dibattito, al di là degli schieramenti e quindi al di là delle maggioranze e delle opposizioni. Per quanto riguarda l'Italia dei Valori,

Credo che il comportamento mantenuto in Commissione prima e in Aula dopo non consenta assolutamente di dare un giudizio che non sia di estrema serietà per una battaglia nella quale crediamo che abbiamo deciso di sostenere dentro e fuori dall'Aula. Si tratta di una battaglia nella quale pensiamo di non essere isolati nel Paese. Certo, gli eccessi sono fisiologici alla democrazia,

Ho apprezzato la conduzione dei lavori della Commissione giustizia e, in particolare, l'atteggiamento del relatore, che in alcuni casi si è rimesso all'Aula. Debbo constatare che la sensibilità evidentemente è stata al relatore, che da alcune parti ho sentito addirittura definire relatore di minoranza. Ricordo ai colleghi che così lo hanno definito che si tratta di un relatore di una Commissione, indipendentemente dai ruoli di maggioranza o di minoranza, perché esaminavamo un provvedimento che nasceva nel Parlamento. L'Aula non ha ritenuto di valutare le aperture offerte dal relatore rispetto ad un miglioramento del testo; non ha ritenuto di considerare fondate alcune osservazioni che per noi invece lo sono, esposte dal senatore D'Ambrosio;

Debbo apprezzare invece il relatore che ha fornito giurisprudenza all'Aula sull'utilità del mantenimento nel codice dell'articolo 416-*ter*. Probabilmente più avanti mi auguro che non sia così - capiremo perché questa esclusione sia stata così fortemente voluta da una maggioranza trasversale rispetto a quella che oggi governa il Paese. Signor Presidente,concludo fra quelli che hanno ascoltato la richiesta di Papa Giovanni Paolo II alle Camere riunite di un provvedimento di clemenza. Bene, Presidente, non credo che la clemenza che stiamo dando con questo provvedimento sia quella invocata dal Papa. Non penso che egli abbia invocato clemenza per i furbetti del quartiere o per altri che sicuramente non rientrano nella previsione che aveva in mente il Papa quando ci chiedeva di fare questo; probabilmente pensava ai poveri cristi. Penso che con questo provvedimento non salviamo - mi auguro in buona fede da parte della stragrande maggioranza dell'Aula, ma non so se è così - né i poveri,

provvedimento di oggi, si impegna a realizzare ciò che fu progettato nella scorsa legislatura. Questa è la vera soluzione dei problemi di cui tutti abbiamo parlato. Oggi approviamo un provvedimento di clemenza, dopo tanti anni di dibattito, ma insieme a questo anche l'impegno della soluzione finale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo a nome della maggioranza del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani. Devo dire che in questi giorni abbiamo ascoltato le posizioni più disparate e vorrei operare una sottolineatura. In realtà stiamo parlando di uno strumento d'eccezione: questo è l'indulto. Invece abbiamo riempito l'indulto di una serie di riflessioni che sono giuste quando si parla delle riforme strutturali che riguardano il sistema penitenziario e l'ordinamento della giustizia. Stante il collasso della giustizia penale e le condizioni di drammatica precarietà in cui versano le carceri, non vi è dubbio che un provvedimento di indulto sia, allo stato, assolutamente necessario e improrogabile. Sono passati sei anni dal Giubileo, quando un ampio «Cartello sociale» promosse la campagna per l'amnistia, l'indulto e un «piano Marshall» per le carceri e per il reinserimento sociale, vera e unica premessa per contrastare la recidiva e garantire maggior sicurezza ai cittadini. Sono passati quattro anni da quando tutto il Parlamento - ripeto: tutto - applaudì ripetutamente e calorosamente Giovanni Paolo II mentre invocava una riduzione delle pene e un provvedimento di clemenza. E sono, infine, passati sedici anni dall'emanazione dell'ultimo indulto. In questo lunghissimo lasso di tempo, in assenza di risposte, la situazione nelle carceri si è fatta drammatica, tanto che a denunciare l'insopportabilità della situazione, e spesso a chiedere l'amnistia e l'indulto, sono ormai non solo i detenuti e le associazioni ma tutti gli operatori: la polizia penitenziaria, i medici e gli infermieri, gli educatori e gli assistenti sociali, i direttori, gli avvocati, i magistrati. I numeri della crisi parlano chiaro. Non è dunque vero che aumentando le carcerazioni si riducono i reati: è vero esattamente il contrario. Una valutazione seria presuppone che sia conosciuto e riconosciuto un dato di fatto: l'attuale sistema delle pene e dei luoghi preposti alla loro esecuzione non risarcisce nessuna delle vittime del reato ma costituisce invece una gigantesca ferita al diritto e ai diritti, una simbolica e ridondante punizione che serve a nascondere il vuoto della giustizia. Come definire diversamente il fatto che - per limitarsi solo agli ultimi cinque anni, dal 2000 al 2004 ben circa 865.073 persone hanno beneficiato della prescrizione dei reati per i quali erano state inquisite? Queste linee di tendenza, che crescono in parallelo, indicano le due facce non comunicanti dell'amministrazione della giustizia. D'altro canto, va fatto un riferimento preciso anche a quello che sta accadendo negli ultimi otto anni. Se avessi una ragione per essere contrario all'indulto sarebbe l'esatto contrario di quello che ho sentito in quest'Aula: è fin troppo prescrittivo e non si può parlare di inclusione attraverso l'esclusione.

L'indulto rappresenta quindi una delle precondizioni per un ripensamento complessivo del sistema penale e della sua funzione, nella prospettiva di una riforma radicale del sistema carcerario, incardinata sulla promozione di strumenti idonei a un effettivo recupero sociale. Una percentuale alta delle persone in carcere si trova ristretta in attesa della definizione del giudizio e la popolazione carceraria è caratterizzata in gran parte da situazioni di disagio e di emarginazione, sempre più aggravate da scelte politiche e legislative che hanno esasperato la consistenza dei problemi: si pensi ai provvedimenti varati nella precedente legislatura in materia di tossicodipendenza o di immigrazione, ispirati da una logica punitiva che, incurante delle problematiche sottese a una vasta gamma di piccoli reati o alle condizioni drammatiche dei migranti, si è preoccupata soltanto dell'aspetto repressivo, nell'illusione che una sua applicazione estensiva potesse fungere da deterrente contro la reiterazione dei reati. Non è dunque un caso che più di un terzo dei detenuti sia composto da stranieri, e che il numero dei tossicodipendenti sia giunto, alla fine del 2005, a circa 16.000 unità, con una percentuale di sieropositivi che raggiunge il 2,6 per cento. Le condizioni della detenzione sono in generale lesive della dignità umana: secondo una rilevazione effettuata dall'associazione Antigone e da altri dati forniti dall'associazione Papillon, è emerso un drammatico quadro di violazioni: per cento dei detenuti non ha la doccia nella propria cella, ma credo sia inutile parlare di quelli che sono i diritti negati perché sono alla luce e tutti quelli che hanno frequentato le carceri con mandato parlamentare, per il loro lavoro, per verificare quella che è la tenuta psicofisica oltre che le condizioni dei detenuti nel nostro Paese ne è al corrente. D'altra parte, l'ultimo provvedimento, la legge n. 207 del 2003, di sospensione condizionata della pena (il cosiddetto indultino), pur avendo lo scopo condivisibile di superare le difficoltà sorte in seno allo schieramento politico circa l'approvazione di un provvedimento di amnistia e indulto, non ha sortito, e non poteva sortire, l'effetto desiderato di incidere in modo significativo sul sovraffollamento del carcere. Un provvedimento di indulto si rende dunque necessario. A beneficiarne, sarà il sistema carcere nel suo complesso: basti ricordare che agli stessi operatori penitenziari è impedito oggi di svolgere con dignità il proprio lavoro, essendo anch'essi vittime delle inadempienze dello Stato, del mancato stanziamento delle risorse necessarie, delle piante organiche rimaste inattuate, delle promesse inevase. Alcune cifre, particolarmente scandalose, possono dare l'idea della gravita della situazione: su 1.376 educatori previsti dalla pianta organica, ve ne sono attualmente in servizio circa 600, meno del 50 per cento, e lo stesso sottodimensionamento grava sugli assistenti sociali, gli psicologi, il personale amministrativo, quello infermieristico, gli agenti. Attualmente è in servizio un educatore ogni 207 detenuti, un assistente sociale ogni 48, uno psicologo ogni 148. Uno sfoltimento delle presenze in carcere sarebbe dunque propedeutico al varo di un pacchetto di provvedimenti concreti riguardanti le condizioni di vita e di lavoro e di lavoro all'interno del carcere, la formazione, la salute, gli organici, l'istituzione di un difensore civico, le misure alternative alla detenzione, l'affettività. Si tenga inoltre conto che al di là dell'indulto e la grazia, intervento rarissimo e a carattere strettamente individuale, in Italia c'è un solo strumento giuridico che consente di evitare la pena: la sospensione condizionale. Può usufruirne però, soltanto chi sia incensurato, abbia riportato condanne fino a due anni e non ricada nella reiterazione del reato per un lungo periodo di tempo, pena la revoca del provvedimento.

perché si dà per acquisito che se ne trascorrerà in carcere soltanto una parte. Ma questo ragionamento non è condivisibile per due motivi: il primo è che l'altra parte della condanna va comunque scontata, sia pure in misura alternativa; il secondo è che l'accesso alle misure alternative è molto selettivo e chi è socialmente, economicamente, culturalmente più debole rischia di non avere alcuna *chance*, finendo per scontare tutta la «doppia pena» in carcere. Questo *status* *quo* costituisce un motivo in più per approvare finalmente un vero indulto. Entrando nel merito delle tipologie di reato sulle quali l'indulto dovrebbe intervenire, so che all'interno della stessa maggioranza si è sviluppato un dibattito dai toni talvolta accesi riguardo le tipologie di reato che dovrebbero essere escluse dall'indulto, in particolare i reati finanziari, societari e quelli contro la pubblica amministrazione. Pur considerando legittima la preoccupazione di evitare che a beneficiare del provvedimento siano soggetti condannati per reati particolarmente odiosi, come ad esempio quelli che hanno portato migliaia di persone a perdere i propri risparmi, non ritengo che per questo si debba rinviare ancora una volta un provvedimento atteso con trepidazione dalla popolazione carceraria, che non può essere ricattata con lo spauracchio della questione morale. La stragrande maggioranza dei detenuti che usufruirebbero dell'indulto è composta da povera gente, che ha commesso reati che non destano allarme sociale, spesso dettati dalla necessità. È a loro che dobbiamo guardare. In ogni caso, l'indulto dovrà aprire una stagione di riforme del sistema giudiziario con cui garantire la difesa dei consumatori vittime delle speculazioni, la lotta alla grande criminalità economica, la confisca dei beni dei corrotti. Ora, intanto, dobbiamo pensare ai più deboli. Se non lo facessimo,

*(Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo di fronte a un provvedimento sostenuto da gran parte delle forze politiche. Anche noi del Gruppo per le autonomie, sensibili alle istanze di clemenza, riteniamo che i tempi per approvare un provvedimento d'indulto - vista anche la tragica situazione delle nostre carceri - siano maturi. Vogliamo, anche e soprattutto, dare seguito a una richiesta che il 14 novembre del 2002 nell'Aula di Montecitorio fu rivolta all'Italia dal sommo pontefice Giovanni Paolo II. Concedere un atto di clemenza per i detenuti, senza tuttavia compromettere la necessaria tutela della sicurezza dei cittadini: questo fu, in sintesi, l'appello di Papa Wojtyla sempre attento alla tragica situazione delle carceri italiane, nelle quali i detenuti vivono spesso in condizioni di penoso sovraffollamento. Il Papa ci chiese un segno di clemenza verso di loro. Un segno di clemenza mediante una riduzione - non abolizione! - della pena, come chiara manifestazione di sensibilità, nonché per stimolare l'impegno di personale recupero in vista di un positivo reinserimento nella società. Mi permetta, onorevole Presidente, di richiedere che a questo atto di clemenza segua anche un atto di grazia da parte del Capo dello Stato che comprenda quei reati politici compiuti in Alto Adige-Südtirol in una fase di massima tensione per la mancata attuazione delle misure a tutela delle minoranze (prevista dagli accordi internazionali) e che risalgono agli anni '60, ossia un periodo che fortunatamente ormai appartiene alla storia essendo passato quasi mezzo secolo. Tornando a parlare del provvedimento in esame, ribadisco che il Gruppo per le Autonomie è favorevole all'approvazione di questo segno di clemenza. Occorre tuttavia mettere in chiaro una cosa: con l'approvazione di questo provvedimento non si può e non si deve considerare risolto il problema dell'umanizzazione delle carceri. Il problema, infatti, va risolto alla radice. In tal senso tengo a sottolineare che purtroppo l'impronta risocializzativa dell'ordinamento giuridico e il principio di umanizzazione della pena in pratica trovano spesso delle limitazioni. comma, dell'articolo 27 della Costituzione prevede che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». condannato». Occorre pertanto aprire un serio dibattito attorno alle politiche sociali per il sistema penale e penitenziario e promuovere un progetto di integrazione dei detenuti. Entro ora nel merito del provvedimento posto all'attenzione di quest'Aula. L'indulto non si applica ai reati gravi come terrorismo, mafia, strage, pedofilia, prostituzione minorile, violenza sessuale, tratta di esseri umani, riciclaggio, sequestro di persona a scopo di estorsione e banda armata. Tuttavia, pur accogliendo con favore che il testo trasmessoci preveda l'esclusione delle pene accessorie definitive e temporanee, critichiamo fortemente che l'indulto si applichi per i reati finanziari, fiscali e contro la pubblica amministrazione. Di questo indulto potrebbero beneficiare, in caso di condanna, i responsabili dei più grandi scandali finanziari che ha conosciuto l'Italia: alludo ovviamente ai *crack* finanziari di Parmalat e Cirio. Ci trova pienamente d'accordo, invece, che non potranno usufruire dei benefici di questo provvedimento i colpevoli di reati di usura. Onorevole signor Presidente, usufruiranno di questo provvedimento soprattutto coloro che hanno commesso cosiddetti reati minori. Il ministro della giustizia, Clemente Mastella, ha affermato che l'indulto riguarderà circa 12.000 detenuti che verranno man mano rilasciati. In tal senso, richiediamo con fermezza che, con il loro rilascio, non venga messa in pericolo la sicurezza dei cittadini; esigiamo che gli scippatori, i borseggiatori, i rapinatori, colpevoli non solo del furto commesso, ma soprattutto di aver fatto passare alla propria vittima dei minuti o addirittura intere ore di puro terrore vengano, dopo il loro rilascio, rigorosamente sorvegliati.

Il cittadino ha diritto di pretendere che, in concomitanza con questo atto di clemenza, vengano rafforzate dal Ministero dell'interno le misure di sicurezza e noi intendiamo farci promotori della messa in pratica di questa richiesta. Richiediamo inoltre seri piani di reinserimento sociale, affinché chi uscirà domani dal carcere non si ritrovi a delinquere nuovamente. Con tutte le riserve espresse, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie a questo atto di clemenza, in quanto convinti che questo provvedimento sia necessario per fronteggiare l'emergenza delle carceri, ma al tempo stesso richiediamo che il Governo, ossia il Ministro dell'interno, intraprenda tutte le misure necessarie affinché la sicurezza dei cittadini non venga messa a repentaglio. *(Applausi Presidente, dopo questo intervento in cui contemporaneamente si chiede di liberare i criminali e poi di pedinarli per garantire la sicurezza dei cittadini, credo dovrei concludere subito, perché non avrei più niente da dire.*(Applausi

travaglia tutti i Governi europei, se ne è parlato spesso anche in Consiglio giustizia e affari interni. Quali le misure? Io posso citare quelle che ha messo in atto il Governo precedente, del quale mi onoro di aver fatto parte. Abbiamo cercato, da un lato, di introdurre misure deflattive e, dall'altro, di incrementare la vivibilità e la capacità ricettiva dei penitenziari. Ho citato prima, nel corso del dibattito, la legge Bossi-Fini, nella quale abbiamo introdotto una sorta diindulto permanente per i detenuti detenuti extracomunitari: coloro i quali accettano di tornarsene a casa propria possono essere liberati, se hanno ancora da scontare non più di tre anni. Con questa formula, ne abbiamo già liberati oltre 5.000. Nel frattempo, abbiamo impiegato le risorse, sicuramente scarse, che avevamo a disposizione. Abbiamo creato 6.000 nuovi posti all'interno dei penitenziari, passando da 41.000 a 47.000 posti disponibili. Abbiamo creato anche strumenti finanziari innovativi, quali il*leasing*, con il quale stiamo costruendo un nuovo padiglione a Bollate, e stiamo tentando, superati gli intralci burocratici, di costruire due nuovi penitenziari. Abbiamo ideato una nuova società di

della quale ho visto con piacere stamattina che è stato approvato un ordine del giorno, che consentirà al Governo di proseguire su questa strada. Abbiamo quindi cercato di fronteggiare il fenomeno, senza mettere a repentaglio la sicurezza e il desiderio di giustizia dei cittadini. Oggi cosa si fa? Si prende una scorciatoia - questo è del tutto evidente - e si dice che siccome lo Stato non è in grado di fronteggiare il fenomeno, anzi siccome questo Governo non ha voglia di affrontare tutti gli impegni, i rischi, le difficoltà

É stato recato un *vulnus* enorme ai cittadini. È stato creato un *vulnus* alla voglia di lavorare degli operatori di polizia, signor Presidente e colleghi. Pensate allo stato d'animo delle nostre forze dell'ordine che da domani si vedranno sbeffeggiate da quei criminali che magari pochi giorni prima avevano assicurato alla giustizia. Pensate con quale stato d'animo i nostri operatori delle forze dell'ordine avranno voglia di rischiare la vita, come fanno tutti i giorni,

Un Ministro della Repubblica ha dato dei ladri alla propria maggioranza, signor Presidente e colleghi. Questo fatto non può passare inosservato!

che cinicamente sta sfruttando un momento per lui, credo, mediaticamente ed elettoralmente favorevole, bensì una questione che riguarda i rapporti nella maggioranza e soprattutto tra Parlamento e Governo. Credo che sia chiaro che voteremo contro.

è molto difficile prendere la parola nel Senato su un tema come quello dell'approvazione di questo provvedimento che reca la concessione di indulto perché la discussione, sebbene contenuta per un insieme di ragioni in uno spazio di tempo tutto sommato breve, ha messo in evidenza le ragioni contrarie alla concessione dell'indulto con molta forza da parte di un movimento politico che fa parte della maggioranza di Governo, di singoli parlamentari, alcuni dei quali hanno ricoperto compiti di straordinario rilievo (mi riferisco al collega D'Ambrosio, procuratore capo della Repubblica di Milano). Abbiamo ascoltato i colleghi che hanno ricoperto nel Governo Berlusconi incarichi di grande rilievo come l'amico e collega Castelli, ministro della giustizia; collega Mantovano; i colleghi di Alleanza Nazionale. Quindi, è molto difficile forse spiegare perché l'UDC anche al Senato come alla Camera dà un voto convinto a favore di questo

l'ultimo indulto fu concesso in questo Paese nel 1989, diciassette anni fa; e dal 1992, in base ad una legge costituzionale approvata allora, è previsto che l'indulto come l'amnistia siano concessi a maggioranza dei due terzi dei componenti delle Assemblee. Soffermiamoci un attimo a riflettere su questi due fatti. Diciassette anni fa, nel 1989, era un periodo nel quale si concludeva una vicenda di politica internazionale di grande rilievo, com'era quella dell'Unione sovietica e del Muro di Berlino. La legge costituzionale del 1992 porta a maggioranza dei due terzi i provvedimenti di amnistia e di indulto che precedentemente erano stati approvati con molta frequenza, come abbiamo ascoltato anche in questa discussione, tra il 1947 e il 1992, appunto. Tutti ricordano altrettanto l'importanza straordinaria del primo provvedimento di amnistia dell'allora ministro della giustizia, Togliatti, che riguardava evidentemente un fenomeno di straordinario significato politico-storico per questo Paese. Ho la pretesa di ritenere che stiamo dando vita, in questo dibattito al Senato, a qualcosa di analogo rilievo, molto maggiore delle critiche che abbiamo ascoltato,

ma perché attengono alla normalità del provvedimento, cioè alla percezione che si tratta di un provvedimento normale. A mio giudizio così non è così non è per due ragioni: una di carattere molto storico ed è la ragione per la quale l'UDC ha votato a favore di questo provvedimento alla Camera e la ragione per la quale vota a favore del provvedimento al Senato. Vi è una radice fortissima di ispirazione cristiana, che non è il carattere umanitario, non è l'appello del Santo Padre soltanto perché è di tipo buonistico; la radice profonda dell'ispirazione cristiana - voleva e ha voluto per molti secoli - che le istituzioni carcerarie fossero nel centro della vita cittadina,

Vi era una radice cristiana che insegnava che visitare gli infermi ed i carcerati era un dovere dei cristiani. Questo dovere è la radice per la quale riteniamo che questo provvedimento, per la prima volta adottato dopo il 1989, ha un valore strategico di cambiamento. Occorre che noi ci riappropriamo del senso dell'appartenenza, delle sanzioni, che sono destinate a privare della libertà le persone, come fatto che ci riguarda non come fatto che riguarda solo altri. Non è solo un fatto di eccessiva sovrappopolazione delle carceri, problema anch'esso importante. Anche se non ci fosse la sovrappopolazione il problema ci riguarderebbe, perché non può essere irrilevante il fatto che questa rimozione l'abbiamo vissuta per molto tempo come psicologica, psicoanalitica e anche fisica. Con questo provvedimento tendiamo a riappropriarsi del problema carcere come problema anche nostro.

Mi riferisco soprattutto ai colleghi della sinistra di provenienza di analisi marxista della società e lo dico con cognizione di causa, perché ho cominciato a occuparmi seriamente di questo fenomeno, e forse non l'ho mai fatto a sufficienza, trent'anni fa quando insegnavo alla facoltà di scienze politiche dell'Orientale. Allora, un corso speciale di diritto costituzionale fu suggerito dagli studenti sul tema della Costituzione nelle carceri. Da loro ho imparato a capire che si trattava di un argomento molto diverso da quello con il quale abbiamo fatto i conti quando abbiamo affrontato il problema dell'amnistia e dell'indulto.

che vi è il tentativo di riappropriarsi politicamente di una funzione che impropriamente per molti decenni è stata attribuita all'ordine giurisdizionale *(Applausi dal Gruppo* *UDC)* come funzione in base alla quale si decide

a riappropriarci di una parte del potere legislativo che riguarda la sanzione delle carceri. Ovviamente se questo è l'inizio di una riflessione complessiva, questa deve partire dal codice penale, dalla gerarchia dei reati, in ordine ai quali vi è l'affollamento nelle carceri di un tipo anziché di un altro tipo. Nell'ordine del giorno che abbiamo approvato, per le parti che abbiamo approvato, vi è ovviamente l'indicazione della sollecitazione a ripartire dal codice penale. Non vi è dubbio che il problema dell'affollamento è strettamente legato al tipo di reato al tipo di reato che è una conseguenza di com'è organizzato il codice penale, che non è l'ultimo dei codici sui quali porre mano. Mi sembra del tutto significativo che per la prima volta diamo vita a un provvedimento di indulto dopo quella che noi consideriamo la fine della prima Repubblica, che è avvenuta, anche per quanto riguarda il mio partito, probabilmente perché avevamo capito fino a che punto, avendo introdotto la regola dei due terzi per la concessione dell'amnistia e in quel momento stavamo rinunciando come partito (mi riferisco a quelli che erano nella Democrazia Cristiana all'epoca) all'esercizio di un potere legislativo che ritenevamo in fondo nostro proprio dal 1948 in poi e che invece stava diventando un potere cogestito nel quale occorreva la convergenza all'epoca all'epoca del maggior partito di opposizione che era ancora il partito comunista dopo la caduta del muro di Berlino. Oggi invece si tende a mettere insieme due culture radicalmente diverse. queste riconosce una maggior libertà nel momento della commissione di reati e quindi fa parte di una generale cultura liberale anche da questo punto di vista. Sono molto

che coloro i quali saranno liberati dallo *status* di carcerati dovranno ovviamente non essere messi in condizione di dover tornare nelle carceri di lì a pochi mesi. Questo è un problema di di reinserimento nella società civile che riguarderà, lo dico ai colleghi, molto di più quanto non sia avvenuto alla Camera il problema delle pena accessorie. Il reinserimento nella vita civile, infatti, riguarda le pene accessorie molto più di quanto non si ritenga e vi è un moralismo deteriore che da questo punto di vista fa ritenere le pene accessorie come del tutto irrilevanti. Comunque, Presidente, non ho intenzione di utilizzare altro tempo. Volutamente ho chiesto che l'UDC non partecipasse alla discussione generale perché ritenevo che il lavoro fatto alla Camera fosse più che sufficiente per capire le ragioni politiche di fondo e volevo soltanto aggiungere, dal punto di vista politico, perché è stato chiesto in quest'Aula, per quale ragione gli ex democristiani sono così favorevoli a questo provvedimento. Lo ripeto ancora una volta. Le ragioni sono due: la radice cristiana della nostra ispirazione ci chiede che il carcere ci appartenga e non sia una questione estranea ed il fatto che la politica in questo modo si riapproprierà di una funzione impropriamente attribuita alla magistratura. Sono due ragioni di valore superiore alle preoccupazioni che pure in Aula ho ascoltato. Per queste ragioni il Gruppo dell'UDC voterà compattamente a favore.

verso le diverse sensibilità. È per questo che non scenderemo in polemica con un Ministro autosospeso che manifesta contro la sua maggioranza, ridotta ormai alla rango di Banda Bassotti. Il nostro orizzonte culturale spazia da Cesare Beccaria a Norberto Bobbio, passando per Mario Gozzini e Alessandro Galante Garrone, e non include certo, né Topolino né Walt Disney né tantomeno il fondamentalismo travaglista, non nel senso di un travaglio interiore, ma di un giornalista che scrive su un giornale di sinistra. Il nostro impianto costituzionale è incentrato sul principio di eguaglianza e di legalità, intimamente connessi, un'eguaglianza che deve essere, non solo formale, ma anche sostanziale, e una legalità che, proprio a causa dell'impossibilità di garantire ai cittadini l'uguaglianza, specie quella sostanziale, può essere violata per previsione costituzionale. Non c'è dubbio che la grazia, l'indulto e l'amnistia rompano il patto di legalità tra i cittadini e lo Stato, come pure non c'è dubbio che tale rottura sia permessa dalla Costituzione, che pure si pone come garanzia suprema della legalità. Non c'è una contraddizione costituzionale. L'articolo 3, comma secondo, dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. La stragrande maggioranza dei detenuti deve questa loro condizione proprio alla mancata rimozione di quegli ostacoli. È per questo che un provvedimento di clemenza non può non essere visto come una delle tante possibilità di risarcimento sociale impostaci dalla Costituzione. Certo ci vogliono riforme strutturali per svuotare le carceri, prima tra tutte un approdo al sistema penale minimo con un sostanzioso ricorso alle pene alternative al carcere, poi il depotenziamento dei meccanismi di incarcerazione che stanno aumentando in modo esponenziale in Italia, in Europa e in tutto il mondo. L'ex ministro Castelli non ha detto perché, ma questa esponenzialità della incarcerazione è data proprio dal fatto che si risponde sempre più col carcere, la più economica delle soluzioni, ai problemi dell'emarginazione sociale, dell'immigrazione, della malattia mentale (in Francia stanno rimettendo in galera i malati mentali) e della droga, tanto per indicare alcune delle più importanti autostrade che portano alla reclusione o, meglio, all'esclusione dalla vita civile. Non costruiamo più carceri. Tutti gli studi criminologici ci dicono che più ne costruiamo più le riempiamo. Cerchiamo perlomeno di non mandarci chi, potendo avere delle opportunità, non sarebbe destinato a andarci e poi di dare a chi ne esce una opportunità di ravvedimento. Non appelliamoci alla certezza della pena, perché in Italia la certezza della pena già c'è,

la validità di un sistema giudiziario o di un sistema difesa può essere testata, come si suol dire, sotto molti punti di vista (la lentezza dei processi ed altro). Uno dei *test* più importanti è il carcere. Ebbene, siamo passati dal fascismo alla democrazia con tutta la sua Costituzione, da un'Italia contadina ad un'Italia postfordista, ma la composizione

ora c'è anche un mare di extracomunitari e, quindi, si può affermare che in galera ci va chi non sa leggere, chi non sa scrivere e chi non sa neanche parlare. È a questi che noi dobbiamo guardare!

rappresenta uno stimolo a porre mano ad una seria e complessiva riforma del nostro sistema penale: l'unica riforma che potrebbe rendere inutile nel futuro il varo di un'ulteriore amnistia o di un ulteriore indulto. *(Applausi

Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare il voto finale che sarà espresso dai componenti del Gruppo di Alleanza Nazionale sul disegno di legge di concessione dell'indulto, con l'eccezione - in tutta ovvietà - di quei senatori che, a titolo personale, hanno già fatto sapere o faranno eventualmente sapere con dichiarazioni in dissenso di vederla diversamente. Per quanto riguarda Alleanza Nazionale (che è e continua a rimanere contraria rispetto alla «scorciatoia» del provvedimento di clemenza, come temporanea e quindi inidonea soluzione a problemi penitenziari e di giustizia, che hanno ben marcato carattere strutturale), marcato carattere strutturale), «vederla diversamente» vuol dire, signor Presidente, considerare la concessione dell'indulto cosa giusta e opportuna in sé, oltre che cosa giusta ed opportuna per come è stata congegnata dalla maggioranza di parlamentari, che si è formata alla Camera dei deputati e che si formerà qui in Senato. Alleanza Nazionale ritiene invece che vi siano forti e fondati argomenti che militano nella direzione del considerare il disegno di legge incongruo e mal concepito, per le sue contraddittorietà, per le sue palesi incongruenza ed inopportunità

un Paese che, malgrado taluni cattivi maestri e taluni non autorevoli portatori di diversa opinione, crede nel diritto e non nel «diritto ad orologeria», come inevitabilmente è quando un Paese che, non riuscendo a garantire giustizia, fa finta di risolvere il problema assumendo che non vi sia (in un certo momento) alcuna ragione per aver "bisogno di giustizia". Il disegno di legge è inaccettabile in sé anche perché è contrario a princìpi di giustizia; perché è rappresentativo di una giustizia con la logica dello sconto; perché è rappresentativo di un Paese che non è in grado di esprimere una direzione di marcia seria ed univoca, in una decisiva area del confronto sociale e delle esigenze sociali, qual è quella della tutela dei diritti e della necessità di sicurezza, cioè - in uno - della determinata aspirazione dei suoi cittadini ad una buona qualità di vita, che sia legittimo compenso delle fatiche, delle rinunce e degli sforzi che sono da essi quotidianamente affrontati; ancora, perché (ahimè) contribuisce a dipingere il nostro Stato, soprattutto agli occhi degli interlocutori internazionali, come il Paese del "tutto che finisce in burletta", in burletta", del "solleone", assai bravo nell'enunciare i grandi princìpi e assai rapido nel trovare le più rapide soluzioni per non rispettarli. Ho ricevuto in questi giorni, colleghi di Forza Italia, come tutti voi, le perorazioni dell'industria dell'informatica, della musica, del cinema, della letteratura, di quell'industria che abbiamo ascoltato con attenzione quando si è trattato di stabilire leggi, anche severe, a protezione dei loro saperi, che sono i nostri attuali e futuri saperi, dall'indebita appropriazione degli stessi ad opera di scaltre organizzazioni criminali, maestre del doppio reato, del furto di beni di altri e dello sfruttamento di poveracci per la relativa rivendita. Quell'industria oggi ci chiede di escludere dal novero dei reati che beneficiano dell'indulto quelli che li riguardano. Vi chiedo scusa, colleghi, e chiedo scusa a chi ha fatto la richiesta, ma non ho potuto trattenere il sorriso per la doppia ingenuità: come è possibile chiedere a chi è determinato a concedere indulto, senza pensare di escludervi, per esempio, coloro i quali hanno compiuto omicidi, con le sevizie successive di cui ancora in questi giorni siamo stati costretti a leggere, e di escludervi invece coloro che, meno sanguinosamente, trafficano con i beni della proprietà intellettuale? E come è possibile - posto che in carcere di costoro non ve ne è uno - chiedere a chi vuole l'indulto di platealmente smentire il grande alibi, che è quello della norma svuota carceri? In ogni caso ad Alleanza Nazionale, formazione politica come è, che ha quale proprio fondante valore quello di essere composta da gente, fra la gente, non può appartenere un provvedimento che è testimonianza, invece, di incolmabile distanza tra lo Stato e chi Governa lo Stato, tra il comune sentire delle persone e chi governa le persone. Ci ha ripetuto il ministro Mastella, ci ripetono i colleghi della maggioranza, che quella dell'indulto è una misura indispensabile prima dell'estate, prima del momento di maggiore sofferenza per chi si deve misurare con le ristrettezze del carcere, e che tale è la ragione per cui è stato necessario imprimere al provvedimento l'irragionevole accelerazione che ne ha di fatto impedito anche il più banale miglioramento. Mi vengono in mente, signor Ministro, un bel po' di anziani e di nostri concittadini senza condizionatori d'aria e tuttavia altro non posso che dirle si tratta di una bugia, questa sua e della sua maggioranza, che è bugia fra le tante di questi giorni, che non ci è sfuggita, e che non sfuggirà alla gente. Si tratta di una bugia che fa il paio con quella che è rappresentata dalle ispirate parole con cui il ministro Bersani e il vice ministro Visco hanno cercato di giustificare le loro recenti iniziative. Si tratta di una bugia, perché ben sappiamo, signor Presidente, che è banale tattica politica (della politichetta con la «p» minuscola) quella di assestare all'inizio della legislatura i colpi più duri e meno graditi agli elettori - tasse e amnistie, fra questi con la convinzione che gli elettori poi dimenticheranno, in quell'attitudine tutta italiana all'assuefazione, nel tempo che intercorrerà rispetto alle successive elezioni. Non sarà così questa volta, perché le successive elezioni non si faranno attendere, non solo perché siete una maggioranza composta da pochi, ma soprattutto perché siete una maggioranza composta da arroganti, fedeli servitori non di chi vi ha fornito il voto per governare, in tutta buona fede, ma solo di quei poteri forti, vecchi e nuovi, di quelle cupole e di quelle nomenclature che non vi hanno lesinato il loro appoggio, e che vi hanno fornito i loro strumenti (scrutatori e presidenti di seggio compresi), perché poteste vincere il confronto elettorale, nella ridicola misura con cui l'avete peraltro vinto. Non sarà così questa volta, perché non dimenticheranno i professionisti, non dimenticheranno gli ingegneri, i dottori commercialisti, gli avvocati, i farmacisti, i tassisti, i panettieri, tutti coloro che pagheranno il conto della vista lunga del ministro Bersani, e del braccio corto del vice ministro Visco. Non sarà così questa volta, perché non dimenticherà la gente che ha subito le conseguenze dei reati che sono oggi da voi perdonati e dalla gente che subirà le conseguenze dei nuovi reati che saranno compiuti a partire da domani. Ho detto prima delle bugie, tra le bugie. E devo aggiungere, le omertosità, tra le omertosità. Devo dare atto, in relazione a queste ultime, che il presidente della 2a Commissione, senatore Cesare Salvi, non ha avuto esitazione alcuna ad accogliere con intelligenza politica - e con intelligenza, e basta la mia richiesta che fosse ascoltato il Ministro dell'Interno o chiunque del suo Dicastero, a qualsiasi livello, fosse dallo stesso ritenuto, perché il Ministro dell'Interno ci dicesse quali sono le sue previsioni, le sue valutazioni e le iniziative preventive, soprattutto, con riferimento all'aumento dei reati atteso nei prossimi mesi, in conseguenza della ritrovata libertà - in alcuni casi della completa libertà - da parte di decine di migliaia di persone la cui stragrande maggioranza è costituita da delinquenti professionali e abituali nella sostanza. Mi spiace per il senatore. Manzione, che si è un po' lamentato della reiterazione dell'argomento, ma il fatto è - e resta - che il Ministro dell'Interno non è venuto, il Ministro dell'Interno non ha risposto. Non ha ritenuto che fosse ragionevole che il Parlamento fosse informato, prima di decidere di quali saranno, per i cittadini, per il Paese, per la sua economia, le conseguenze del provvedimento che sarà deliberato. Forse la verità è che il Ministro non ha avuto il tempo per pensarci; forse il Ministro non sa quali conseguenze possono attendersi e forse le vorrà apprendere dopo, a cose fatte, così come il senatore Brutti ha ieri cercato di convincere che è intelligente che sia. sia. Forse, è meglio il silente ed assente Ministro dell'interno, rispetto a chi, dalle parti della giustizia, non ha viceversa avuto il minimo riguardo, non solo istituzionale, ma finanche personale, nel rappresentare in maniera falsa ed omertosa la situazione per come si assume che sia. Ci è stato detto che il provvedimento di indulto riguarderà circa 12.750 detenuti e che il Ministro ha stimato tale numero tenendo conto - in anticipo rispetto a quando questo è poi accaduto che la Camera avrebbe da una parte aumentato il relativo numero, portando dal 31 dicembre 2005 (come era nella prospettazione iniziale) al 2 maggio 2006 la data entro cui potevano essere impunemente compiuti reati dai soggetti interessati. In secondo luogo, ci è stato altresì detto che la Camera avrebbe da altra parte diminuito il relativo numero, escludendo chi ha compiuto taluni reati. Ci fa piacere apprendere che ai cento sottosegretari che il presidente Prodi ha voluto intorno a sé ora si sia anche aggiunto, nell'ombra come gli è caratteristico, anche il mai sufficientemente lodato Otelma, mago e divinatore, perché solo a questi sarebbe riuscito un esercizio come quello che ci è stato propinato; che è stato propinato a me, signor Presidente, ma anche a colleghi senatori come Castelli e D'Ambrosio, che - non tra le stelle, ma assai più semplicemente sul sito Internet del DAP (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) hanno letto il vero numero dei detenuti che saranno resi liberi senza aver espiato pena, o avendola espiata solo

Il provvedimento di indulto non riguarda i soli detenuti ed è quindi una bugia quella di chi sostiene che si tratta di un provvedimento di clemenza verso chi è in carcere. Il provvedimento di indulto riguarda infatti un numero almeno dieci volte superiore a quello dei detenuti indicati dal ministro Mastella, perché riguarda infatti anche le circa 50.000-60.000 persone affidate, con libertà limitata e controllata, agli Uffici dell'esecuzione penale esterna, perché riguarda anche le ulteriori 60.000 persone che, condannate in via definitiva, sono in attesa che i tribunali di sorveglianza si pronuncino proprio sul fatto se esse devono essere destinati al carcere o, viceversa, all'Esecuzione penale esterna. Circa 140.000-150.000 persone che hanno commesso reati saranno da domani

Non perché si sente migliore di qualcun altro - come lei ha poco fa sussurrato - ma perché ha sempre creduto in una giustizia che non fosse mai esemplare, ma semplicemente proporzionata ed effettiva e non ha cambiato ora idea.

eccezione, che deriva dall'entità di tempo che ha diviso un precedente provvedimento rispetto anche a quello che nel 1992 ha deciso il Parlamento, con legge costituzionale, indicando che occorrevano due terzi

non è un'eccezionalità politica, non crea degli archi rampanti tra chi è all'opposizione o chi alla maggioranza attuale. No, non è questo e mi spiace che non sia stato colto da molti. Questa è una valutazione che che la Costituzione chiede al di là delle differenze politiche, che restano e dividono gli schieramenti, quando il problema investe questioni molto diverse, che sono etico-politico-giuridiche e insieme rappresentano la politica nel senso più greco del termine, intendendo cioè quello che è necessario in un determinato momento storico. eviterò le polemiche con chi va a mezzo servizio tra il Governo e l'opposizione: capisco la tentazione propagandistica, l'ho praticata tante volte anche io. Questo, tuttavia, è un tema che non lo consente. Ho avuto piacere che il collega Formisano abbia fatto un discorso molto misurato, gliel'ho detto di persona, perché è così che si manifestano le diversità. Tuttavia desidero dire che Forza Italia nel prendere questa posizione è convinta, non da motivi d'interesse politico e nemmeno propagandistico,

come vuole la Costituzione, senza vincolo di mandato, ognuno a seconda delle proprie convinzioni e dei propri sentimenti.

molte volte si va in galera anni dopo il reato commesso. La durezza della carcerazione significa anche l'abbandono di un recupero che la vita civile aveva consentito. Certo, si è commesso un delitto. I delitti e le pene sono certamente gemelli nella necessità che siano gli uni prevenuti e gli altri repressi, quando è necessario.

Non credo che chi decida in un modo possa appartenere alla Banda Bassotti e qualcun'altro alle pie vergini, che assumono atteggiamenti sempre all'insegna di una castità che è tutta da dimostrare. Credo, invece, che in un caso come questo, la nostra scelta debba essere estremamente e rigorosamente razionale. Nel carcere - chi ci è andato lo sa convive una realtà vergognosa. Ho difeso recentemente un pentito che poi si è pentito e ha militato dalla parte ritenuta sbagliata da qualche parte della magistratura. Ha scritto tante lettere di sofferenza, poi ho saputo che a Busto Arsizio è morto suicidato o suicidatosi: è ancora in corso l'inchiesta. Mi chiedo quanti non resistano a una vita carceraria dove la compressione della comunità le stesse opportunità che il carcere offre - la stessa televisione e la radio - sono motivi di tortura nella convivenza compressa della gente che sta insieme. Perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, quando discutiamo di queste cose dobbiamo immaginare che da una parte ci siano i giustizialisti e dall'altra i garantisti? Non è così; è nel processo che devono esservi le garanzie. Quando si riceve una pena, questa deve essere scontata, ma lo Stato, nella Costituzione, ha previsto l'indulto: a chi è stato affidato il compito di decidere sull'indulto? Non è più il sovrano che, qualche volta, gratificava con il condono i peggiori dei suoi sudditi per assicurarsene i favori, ma è il popolo, oggi, rappresentato in Parlamento, che decide, con una maggioranza

ho avuto, nella mia lunga vita anche istituzionale, occasione di misurarmi sulle questioni che possono, in un determinato momento storico, far scegliere le vie più rigorose e dure e quelle che sono state considerate indulgenziali,

possano avere la speranza di uscire. Si esprime una specie di prognosi negativa: si trasforma la presunzione di innocenza in presunzione di recidiva: è una visione pessimistica della vita.

Ci sono delle persone che, recuperata la propria libertà, la mettono a capitale di una speranza di vita. Ci saranno anche quelli che sbaglieranno ancora e allora la legge prevede che scontino la doppia pena. motivo non vi è, tra di noi, una differenza di valutazione che obbedisca a motivazioni di carattere politico o di carattere partitico. Si tratta

per dismettere questa impostazione cuore contro cuore, cervello contro cervello, perché vi è la necessità di rimuovere le cause che rendono eccezionale oggi la nostra decisione, in modo che i processi siano più rapidi, i rapporti con la magistratura e con l'avvocatura siano più chiari e che si possa svolgere finalmente un grande discorso nuovo su come affrontare, eliminare, elidere i problemi difficili della giustizia. Va bene: il tempo è passato ed è anche il momento che io dica che Forza Italia voterà convintamente a favore di questo provvedimento.

la discussione e lo schieramento che si è delineato in materia di indulto nella giornata che abbiamo trascorso, rivelano una consapevolezza largamente diffusa nel Senato e nel Parlamento italiano. L'articolo 27 della Costituzione prescrive che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Ebbene la nostra consapevolezza larga, che va la di là delle divisioni politiche, è che i fatti, le condizioni concrete di vita nelle carceri si discostano drammaticamente da questa norma costituzionale: essa non trova applicazione ed è per questo che, da più parti, ci si interroga su quel che si deve fare per intervenire qui ed ora, subito, senza rinvii, sulla condizione di sovraffollamento, di disagio, di disperazione che è propria dei penitenziari italiani. l'onorevole Bossi, nei giorni scorsi, in un'intervista alla «Repubblica», ha dichiarato la sua disponibilità ad un provvedimento di clemenza; disponibilità teorica che prescindeva dalla proposta che poi sarebbe stata avanzata, eppure è il segno di una sensibilità che va al di là delle opinioni politiche, al di là degli schieramenti e che si muove di fronte ad un dramma:

privati di qualsiasi prospettiva di recupero e gli stranieri, gli stranieri poveri. Nel 2005, cento degli stranieri che sono entrati nelle carceri italiane vi sono entrati per la violazione delle norme in materia di espulsione. dobbiamo distogliere lo sguardo dalle condizioni drammatiche della popolazione carceraria, dobbiamo intervenire. Tutto questo pone alla collettività e allo Stato democratico un problema ineludibile. Ho ascoltato le argomentazioni serie e convinte del collega D'Ambrosio e ho riflettuto in questi giorni sulle parole che egli ha più volte pronunziato nelle nostre riunioni. È vero, occorre intervenire sulle ragioni di fondo che determinano il sovraffollamento, il disagio e la disperazione nelle carceri. per intervenire su queste condizioni di fondo è necessario varare leggi, procedere ad una razionalizzazione delle leggi penali che in questi anni si sono sovrapposte le une alle altre, quasi con un inseguimento delle pene, come se ogni problema della società italiana dovesse essere affrontato attraverso lo strumento della reclusione. Abbiamo bisogno di leggi e di leggi che non possono essere varate senza il confronto, il dibattito e anche la convergenza tra forze politiche diverse, tra maggioranza ed opposizione. Per questa ragione c'è bisogno di tempo, non si varano immediatamente leggi capaci di intervenire sull'emergenza delle carceri italiane. Proprio per questo siamo convinti che se l'obiettivo, la prospettiva è quella che è stata lucidamente indicata dal collega D'Ambrosio, come da altri, sia necessario, per aprire una nuova stagione di riforme, adottare un provvedimento eccezionale, con una riduzione delle pene detentive, che attenui la tensione e il disagio delle carceri italiane. Pensiamo alle persone, alle donne e agli uomini, alla povera gente, a quelli che stanno in carcere per reati minori e pensiamo ai bambini e alle bambine che oggi sono nelle carceri italiane assieme alle loro madri e che si trovano là soltanto perché le loro madri sono state incarcerate, magari per reati lievi.

È un provvedimento eccezionale, sono 16 anni che non si ricorre all'indulto nell'ordinamento italiano. Sono 16 anni: l'ultima volta fu nel 1990 e vi fu anche un'amnistia per reati puniti con pene non superiori ai tre anni. Oggi si propone qui esclusivamente un indulto, una riduzione del carcere, della pena detentiva. Dovrebbero comunque uscire questi detenuti; usciranno prima: questo è il senso della riduzione della misura della pena detentiva. In questa legge vi è l'elenco più lungo che mai vi sia stato nei provvedimenti d'indulto, durante la storia della Repubblica, di reati che vengono esclusi dal provvedimento di clemenza. Abbiamo infatti escluso i reati più gravi, i reati che colpiscono le persone, come la tratta degli esseri umani, la violenza sessuale, i reati che contengono in sé una violenza intollerabile, come il sequestro di persona, i reati che feriscono l'ordinamento democratico, come i delitti di mafia, i delitti di terrorismo e poi altri come l'usura e come tutti i reati che si commettono avvalendosi dei mezzi dell'associazione mafiosa. Vi è insomma una lista assai Non è un'amnistia. L'amnistia cancella i reati, l'indulto riduce le pene e ciò significa che per i reati contro la pubblica amministrazione, per i reati finanziari e per i fatti di corruzione, le responsabilità verranno accertate, le complicità verranno individuate, la verità verrà scoperta,

che saranno messi al bando, che usciranno dalla vita pubblica. Essa non toccherà le pene accessorie temporanee: chi ha commesso reati in qualità di professionista o come membro di un consiglio di amministrazione uscirà dall'attività professionale, verrà messo fuori da quel consiglio di amministrazione. E allora le parole pronunciate in questi giorni dal ministro Di Pietro, le sue argomentazioni non hanno fondamento, questo non è un colpo di spugna! Ed io mi rifiuto di accettare lezioni che si fondano su argomentazioni prive di fondamento, su argomenti che non hanno consistenza. E mi rifiuto tanto più di accettare queste lezioni, poiché esse poiché esse vengono proposte e formulate con parole insultanti. È grave ed è penoso per noi che parole insultanti nei nostri confronti, nei confronti del lavoro parlamentare che abbiamo svolto in questi giorni, vengano rivolte da un Ministro della Repubblica che noi sosteniamo lealmente come membro del nostro Governo. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, colleghi, il Gruppo dell'Ulivo si schiera, prende una posizione, assume una responsabilità. Non siamo di fronte ad una decisione che abbiamo preso in queste settimane a cuor leggero. Essa è il risultato di un incontro tra forze politiche, sensibilità e punti di vista diversi tra loro, perché era necessaria la maggioranza dei due terzi per varare una legge come questa. Tuttavia, questo incontro ha un suo significato: vuol dire che nel Parlamento italiano, quando sono in gioco valori e decisioni che riguardano la vita della nostra società e che toccano la coscienza di ciascuno di noi, è possibile non trattarsi da avversari che non parlano tra loro, da persone che non si conoscono, da

dannosi per tutti - del sovraffollamento, della inadeguatezza delle strutture, della mancata attuazione delle leggi, a cominciare dalla riforma dell'assistenza sanitaria in carcere. Noi voteremo convintamente a favore di questo testo di legge.

la legge che il Senato si avvia a votare è giustificata, o meglio imposta dall'urgenza di sfoltire le carceri per ridurre i disagi e le umiliazioni che aggiungono un aggravio iniquo alla più terribile delle pene, la restrizione della libertà personale. È scritto, lo ha appena ricordato il senatore Brutti, che il trattamento dei detenuti non può essere contrario al senso di umanità. Ma la questione è se per provvedervi occorra e convenga ricorrere ancora una volta, all'ultima ora della canicola, allo strumento dell'indulto. Ritengo che più che un atto di clemenza, l'indulto sia per tradizione un residuo dell'indulgenza dell'antico regime ed in realtà anche una resa dello Stato di fronte alla propria inefficienza. Non credo davvero che nella tradizione dell'indulto vi sia alcunché di liberale, perché quel potere che concede clemenza può anche negarla a suo piacere, mentre le garanzie di giustizia, comprese quella dei carcerati, sono diritti del cittadino e non concessioni saltuarie del potere. Dunque, l'umanità della condizione carceraria va garantita nelle premesse che la determinano e non negli effetti che la offendono. Non c'erano dunque altre strade, le abbiamo sentite anche qui, si potevano e si possono disporre pene alternative alla carcerazione e non è difficile individuarle, almeno per le due categorie più numerose: i clandestini stranieri e i tossicodipendenti. Si poteva e si può, per i condannati alla detenzione, attrezzare carceri adeguate, a cominciare da quelle che, a quanto si sente dire, sarebbero già pronte o quasi pronte, ma restano chiuse per mancanza di fondi. L'obiezione è quella di sempre: gli interventi strutturali hanno bisogno di un tempo che non c'è, ma io frequento, salvo un consistente intervallo, il Parlamento dal 1976, e per trent'anni ho sentito ripetere quella obiezione, devo per ciò ammettere *pro quota* anche a mio carico che il tempo c'era. Temo che il ricorso all'indulto varrà soltanto a spostare ancora una volta il tempo degli interventi strutturali. Non credo che la soluzione sia giusta se si paragonano i suoi suoi benefici presunti con i costi più che probabili. Per questi motivi, signor Presidente, che non hanno nulla a che vedere con i tatticismi politici e credo non deroghino al senso della giustizia, dichiaro che voterò contro il disegno di legge.

Noi non voteremo a favore di questo pessimo indulto, daremo un voto d'astensione, consapevoli che al Senato equivale ad un voto contrario. Condividiamo quanto detto dall'onorevole Bulgarelli, perché a Bulgarelli ci unisce un rapporto profondo di stima e di amicizia, ma per una di quelle contraddizioni non così rare nei rapporti e nelle relazioni, che a volte si determinano, le sue stesse considerazioni ci inducono a trarre conseguenze diverse. Noi conosciamo bene le condizioni in cui versa la popolazione carceraria. L'attività politica mi ha portato qualche anno fa a conoscerla bene, a studiarne le tremende condizioni, a tentare di individuare possibili rimedi, che non sono quelli di un indulto in cui si ravvisano con chiarezza scambi intervenuti tra forze politiche anche avversarie. Il sovraffollamento carcerario deriva dal fatto che nelle galere vengono rinchiusi i problemi sociali che non si sanno o non si vogliono affrontare, perché difficili, certo, complicati, a volte persino disperanti, ma ineludibili, se vogliamo che le nostre carceri abbiano una parvenza di civiltà. Nelle carceri vengono rinchiusi problemi sociali come la tossicodipendenza e l'immigrazione. Dico per inciso che gli immigrati in Italia hanno il privilegio di godere di due tipi addirittura di detenzione: le galere e i CPT, più che dell'indulto hanno bisogno dell'abrogazione urgente della Bossi-Fini. Il sovraffollamento è dovuto al fatto che non si ha il coraggio di depenalizzare radicalmente il codice penale. Troppe sono le resistenze miopi, egoiste, anche autoritarie; il sovraffollamento deriva dal fatto che non esistono gli strumenti di recupero previsti, che il carcere non viene inteso come misura finale, estrema, ma come prima, e anche impotente socialmente, misura. Ci sono tutte le ragioni, più di quelle che ho elencato, che rendono necessario l'indulto, ma se la ragione prima è davvero quella del sovraffollamento, perché comprendete reati che in realtà non affollano affatto le nostre galere? Voto di scambio mafioso, colletti bianchi, truffe contro i risparmiatori, delitti contro l'integrità dei lavoratori, reati fiscali, sì, cari colleghi, reati fiscali. Quanta gente c'è in galera che si è macchiata di questi delitti? Che messaggio manda un indulto per i delitti contro i lavoratori ad un Paese, dove i morti sul lavoro, gli omicidi cosiddetti bianchi, sono in media - sono dati dell'INAIL - quattro al giorno. Che messaggio manda l'indulto per i reati fiscali ad un Paese dove l'evasione ha una unica eccezione, quella dei lavoratori dipendenti, perché a loro si applica direttamente il prelievo sulla busta paga?

Onorevoli colleghi, la votazione finale del disegno di legge al nostro esame, per la cui approvazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato, avrà luogo mediante procedimento elettronico. ***Votazione nominale

*Il Senato approva.*

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per un comprensibile contrattempo, giustificabile in giornate complesse come quella di oggi, non ho potuto rendere la mia dichiarazione di voto quando sarebbe stato forse più ragionevole farla. Mi preme dire *a posteriori,* comunque, che esprimermi positivamente

Non infierite su una persona che ha commesso un errore, per favore. Sono anch'io quasi un novizio dell'ambiente...

Per rispetto ai colleghi che altrimenti avrebbero il dubbio sul momento della conclusione della seconda parte per potersi recare a votare, chiedo che si voti prima sulle dimissioni dei parlamentari

Voglio precisare che per quanto riguarda la decisione dell'ordine del giorno, avendolo fissato questo con il parere

nel ricordare come il nostro Gruppo abbia apprezzato la coerenza del Presidente del Senato, allorquando stamattina era stata prospettata un'inversione dell'ordine dei lavori che andava a contraddire la lunga la lunga mediazione attraverso la quale si era arrivati a un calendario approvato all'unanimità, mi permetto, prendendo atto che il richiamo al Regolamento e la sua applicazione non sono che una garanzia per tutti - quindi, se viene

Per la verità non ero a conoscenza del fatto che il problema fosse stato già posto questa mattina, perché in quel momento non ero in Aula, quindi ritiro la proposta avanzata. La Commissione mi ha autorizzato a riferire oralmente: normalmente non mi piace depositare il

prenderà atto. Voglio solo ricordare però che nella passata legislatura, molto spesso, decine di volte, si è modificato il calendario deciso dalla Conferenza dei Capigruppo

con il disegno di legge in esame il Governo propone la sospensione di alcuni dei decreti attuativi della riforma dell'ordinamento giudiziario approvati nella precedente legislatura. Le ragioni di sintesi, richieste dalla breve discussione appena svoltasi mi portano ad indicare soprattutto i punti politici di questa scelta del Governo e delle intenzioni del Governo e della maggioranza.

D'altra parte, occorre considerare le materie affrontate dai tre decreti in questione, concernenti la formazione e la professionalità dei magistrati, la distinzione di funzioni tra pubblico ministero e giudice, l'esigenza di una tipizzazione dell'illecito disciplinare e le maggiori garanzie per il cittadino circa il fatto che di fronte agli illeciti dei magistrati ci sia giustizia, un sistema e un'organizzazione delle procure della Repubblica che - pur senza avere la rigida gerarchizzazione del sistema previsto dalla riforma - non comporti tuttavia un ritorno alla situazione pre-esistente perché la diffusività della funzione del giudice non può essere riproposta negli stessi termini per quanto riguarda la funzione della pubblica accusa. Tutte queste ragioni hanno indotto a proporre, non già l'abrogazione, bensì la sospensione dell'efficacia di questi provvedimenti onde consentire al Parlamento, non di lasciare che nulla sia fatto, ma di intervenire nel periodo di tempo che il Governo ha chiesto in Commissione (fino al luglio del prossimo anno) per introdurre una nuova normativa per ciascuno di questi punti. Una normativa che tenti di porre il tema della magistratura non sul versante del contrasto tra politica e giustizia, ovvero all'interno del sistema giustizia tra avvocatura e magistratura, ma dal punto di vista dei diritti del cittadino. Quindi diritto ad avere una giustizia in tempi rapidi, una giustizia che abbia la sua efficacia e la sua prontezza, soprattutto per i cittadini più deboli dal punto di vista economico e finanziario. Ciò non vuol dire che quello dei tempi e dei costi della giustizia sia l'unico tema da affrontare, anche se è certamente centrale. Sono da affrontare anche Sono da affrontare anche i temi che la legge sull'ordinamento giudiziario ci offre. Noi proveremo a farlo in una prospettiva nuova, guardando la questione, anche in questo caso, dal punto di vista del diritto del cittadino. Quindi diritto ad avere una difesa forte ed efficiente

Nel fare questo vogliamo operare alla ricerca del più ampio confronto parlamentare. Il Governo non ha presentato suoi disegni di legge sostitutivi rispetto ai decreti delegati per la scelta di affidare al confronto parlamentare la soluzione di questi problemi.

la dialettica e perfino lo scontro, ma solo su quelle che il Governo ritiene decisive ed essenziali per la propria funzione di indirizzo politico. Credo che il Governo abbia quindi fatto bene ad affidare al Parlamento la soluzione di questi problemi, perché mi auguro che sarà possibile, superando le contrapposizioni del passato, trovare i più ampi consensi per affrontare questi temi. Una giustizia nella quale il cittadino non ha fiducia non è una giustizia rispondente ai nostri principi costituzionali. Questa è la ragione, signor Presidente, onorevoli colleghi, della proposta del Governo, di cui raccomando l'approvazione. In Commissione abbiamo avuto un confronto molto serrato, perché l'opposizione ha legittimamente difeso - sarebbe stato che aveva sostenuto nella passata legislatura. Mi auguro che alla ripresa dei lavori a settembre, nel tener fermo questo punto di vista, ci sia la stessa disponibilità al confronto e alla discussione che c'è stata in Commissione, in modo che si possa operare tutti insieme

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sulle dimissioni presentate dalla senatrice Turco. I senatori favorevoli ad accogliere le dimissioni premeranno il tasto verde al centro della postazione di voto; i senatori contrari il rosso; i senatori che intendono astenersi il bianco a sinistra.

degli sgambetti parlamentari e del filo di goliardia che ha guidato molte votazioni, desidero dichiarare pubblicamente che voterò contro le dimissioni di questi colleghi senatori,

è null'altro che un *assist* all'azione antiparlamentare che sale dal Paese e che fa di questo nostro mandato uno strumento sempre più derelitto.

Già si afferma che noi siamo senatori nominati perché eletti in liste bloccate; pensate cosa si dirà quando sarà evidente che i partiti che ci hanno nominato hanno anche il potere di revocarci come, se invece di eletti del popolo, fossimo banalmente personale di partito in posizione di comando presso la Camera e il Senato. Allora, se a questa Camera rimane la consapevolezza del suo mandato, della sua dignità e e della rilevanza che si sa dare *(DC-Ind-MA)*. Invito tutti i colleghi a difendere la dignità, la libertà e la sovranità del popolo votando contro l'accettazione di queste dimissioni. Siamo senatori, non siamo impiegati in posizione di comando presso il Senato!

dal legittimo desiderio della maggioranza - che io ho appoggiato, ma della quale non faccio parte - di mantenere la possibilità di controllare, com'è suo diritto, questo sistema. In tutti i regimi parlamentari del mondo, per essere Ministri bisogna far parte di una Camera. Poiché noi non sappiamo in quale regime siamo, possiamo tollerare anche questo, ma non chiamiamola divisione dei poteri. Tipico del regime parlamentare è che non si può essere membri del Governo se non si fa parte di una Camera, salvo la Francia che non è un regime parlamentare, ma è il regime che la Commissione presieduta dall'attuale ministro D'Alema aveva auspicato, cioè il regime semipresidenziale il Presidente della Repubblica eletto dal popolo. Purtroppo, il centro-destra non ha accettato la riforma proposta dall'allora presidente D'Alema. La seconda questione è che non basta che uno dissenta dal Gruppo che lo ha eletto, argomenti anche delicati come possono essere la pace e la guerra. Scusate! Ho usato un termine improprio; dare la caccia ai talebani, fare i rastrellamenti, usare le bombe al napalm,

Indíco la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sulle dimissioni presentate dal senatore Pinza. Dichiaro aperta la votazione. *(Segue la votazione).*

Indíco la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sulle dimissioni presentate dal senatore Bubbico.

scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sulle dimissioni presentate dal senatore Vernetti. Dichiaro aperta la votazione.